con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. Signor Presidente, colleghi, è con profondo dispiacere e commozione che desidero oggi ricordare in quest'Aula il senatore Maurizio Pieroni, che ci ha lasciato nella notte tra lunedì e martedì, colpito da una malattia grave e inaspettata. Maurizio Pieroni è stato consigliere comunale nella sua città, Senigallia, negli anni Ottanta in cui diede vita ad una delle primissime liste Verdi. È stato eletto deputato sempre per i Verdi nel 1992, e poi senatore nel 1994, confermato nel 1996, nella XIII legislatura, in cui per cinque anni è stato Capogruppo dei Verdi in quest'Aula. Lo voglio ricordare proprio qui, tra questi banchi, che lo videro protagonista di tante iniziative, proposte e battaglie. Il suo impegno ambientalista e sui diritti civili ha ispirato tutta la sua iniziativa parlamentare. Cito qui alcune delle proposte su cui lavorò moltissimo per far comprendere quanto la sua cultura ecologista fosse molto ampia e come marcasse un po' tutto il suo lavoro. Penso, per esempio, alla proposta dell'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla corruzione; norme contro la discriminazione motivata dall'orientamento sessuale; al riordino delle fondazioni bancarie; all'istituzione di un sistema di certificazione contro il lavoro minorile; all'istituzione del garante dei diritti animali. Norme

per la sicurezza ambientale; la messa in sicurezza della città di Falconara Marittima. Molte sono le iniziative che lo hanno visto protagonista in quest'Aula. Anche il suo impegno sulle riforme costituzionali fu sempre all'insegna di quella cultura ecologista che è stata la cifra del suo pensiero politico e della sua vita, perché Maurizio Pieroni è stato innanzi tutto un ecologista.

negli anni Ottanta e grazie anche alla sua intuizione e alla sua capacità organizzativa, l'arcipelago verde che nasceva allora - fatto di tante liste e comitati che lottavano per la difesa del proprio territorio, contro le discariche abusive, contro la violenza nei confronti del territorio e del paesaggio - grazie, appunto, alla sua intuizione, insieme a molti altri diede vita alla federazione delle liste a Finale Ligure nel 1986. Quindi, è stato uno dei fondatori dei Verdi e questa è stata la caratteristica di tutta la sua militanza: militante ecologista e dirigente politico. un uomo politico colto, ironico. Il suo ecologismo non è mai stato banale o dogmatico. Oggi, per tutti noi che discutiamo spesso in quest'Aula, la lotta ai cambiamenti climatici, il surriscaldamento globale, l'economia verde, la transizione energetica

quasi una rarità. Avere l'intuizione dell'ecologia era di pochi, di coloro che avevano iniziato a combattere sul proprio territorio per difendere la propria città e le proprie Regioni dall'assalto del cemento, di coloro che pensavano che la chiave ecologista fosse la possibilità di trasformare questo Paese. Abbiamo avuto vittorie insieme e abbiamo avuto anche tante sconfitte. So che lui ha guardato anche all'evoluzione della cultura ecologista, sempre con interesse in questi anni, dando il supporto come meglio poteva. È stato, quindi, importante, per la federazione e per il partito dei Verdi, il suo lavoro e il suo impegno in tanti anni.

perché era ossessionato dall'idea di una partecipazione dal basso, di liste dal basso, di un'idea anche federata della soggettività politica verde. La sua scomparsa ci ha lasciato veramente sgomenti e noi vogliamo essere essere vicini ai suoi cari, alle persone che gli sono state più vicine in questi anni, che non sono stati né facili e né semplici. Gli otto Gli otto anni che ha passato in quest'Aula, nelle Commissioni, hanno lasciato un segno, perché era un politico colto, intelligente e ironico. Egli ha saputo, in tutti questi anni, costruire ponti e trasversalità, perché il suo ecologismo ha sempre puntato a ottenere degli obiettivi immediati, per il bene di questo Paese e per gli obiettivi che ci eravamo posti in tutti questi anni. Lo ricordiamo, quindi, con rimpianto e lo ricordiamo con dolore. Voglio soltanto dire, ancora una volta: grazie, Maurizio, per tutti gli anni che ci hai dato. Addio, e che la terra ti sia lieve. *(Applausi)*.

le ho chiesto la parola avendo ascoltato adesso le parole della senatrice De Petris in ricordo di Maurizio Pieroni. Io ho saputo, in realtà, solamente poche ore fa della sua scomparsa e voglio unirmi alle parole della senatrice De Petris nel suo ricordo, che penso doveroso, in quest'Aula. Voglio farlo da marchigiano, come egli fu, e da democratico, come in qualche modo egli fu, da precursore delle battaglie ecologiste e ambientaliste, che oggi sono tanta parte costitutiva della della coscienza civile e politica dei democratici in Italia, in Europa e in tutto il mondo. Pieroni fu un precursore, negli anni Ottanta, questo impegno civile legato ai temi dell'ambientalismo stava crescendo impetuosamente, intanto, nelle coscienze e, poi, prendendo forma politica in tante parti d'Europa e anche in Italia, con la costituzione della Federazione dei Verdi. Prese poi forma politica nell'Ulivo - lo voglio ricordare - di cui Pieroni fu parlamentare.

innovativa e capace di portare alla nostra cultura politica un valore aggiunto. Se ci sono oggi migliaia di ragazzi in tutto il mondo che reclamano un futuro diverso, un mondo diverso, a partire da uno sostenibile e dal rispetto della compatibilità ambientale, che reclamano di poter consegnare alle nuove generazioni il mondo, il nostro patrimonio ambientale e paesaggistico, così come stato a noi consegnato, lo dobbiamo anche a figure e a personalità come quella di Maurizio Pieroni, che anch'io voglio ricordare.

straordinaria, intelligente e competente attività nel momento in cui è nata una delle esperienze politiche più significative di questi ultimi anni, l'Ulivo. La sua intelligenza, la sua ironia, la sua capacità di trasformare le idee in fatti politici ci mancheranno molto.

Mi unisco al cordoglio espresso dalla senatrice De Petris e dai senatori Verducci e Bressa per la scomparsa del senatore Pieroni e invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri, ha approvato il calendario dei lavori fino a giovedì 30 luglio. Nella giornata di oggi si svolgerà la discussione delle mozioni sull'occupazione giovanile e sulla tutela del patrimonio artistico nazionale. Alle ore 12 il Presidente del Consiglio dei ministri renderà un'informativa sugli esiti del Consiglio europeo. I Gruppi potranno intervenire per quindici minuti, divisibili per due interventi. È prevista la trasmissione diretta televisiva. Al termine dell'informativa, la seduta sarà sospesa e riprenderà alle ore 16,30 per concludere la discussione delle mozioni. Domani, alle ore 15, avrà luogo il *question time*, con la presenza dei Ministri degli affari esteri, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'innovazione tecnologica. Il calendario della prossima settimana prevede, nella giornata di mercoledì 29 luglio, la discussione congiunta del programma nazionale di riforma 2020 e della relazione sullo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale. I tempi di discussione sono stati ripartiti per un totale di sette ore, escluse le dichiarazioni di voto. Si ricorda che per l'approvazione della risoluzione sul cosiddetto scostamento è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Giovedì 30 luglio sarà discussa la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di non concedere l'autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei confronti del ministro *pro tempore* Salvini. Per l'approvazione della proposta, è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Dopo l'effettuazione della votazione nominale con scrutinio simultaneo, non si procederà alla proclamazione immediata del risultato. I senatori che non hanno partecipato allo scrutinio potranno comunicare il proprio voto ai senatori Segretari, che ne terranno nota in appositi verbali fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle ore 18. Sempre giovedì 30 luglio, alle ore 15, avrà luogo il *question time*. Le Commissioni permanenti sono convocate per il rinnovo, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del Regolamento, mercoledì 29 luglio nei seguenti orari:

poi stiamo qua a dire che non c'è lo spazio d'iniziativa legislativa e si fanno solo i decreti, perché c'è l'emergenza.

1686, che riguarda l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari, anch'esso licenziato dalla Commissione.

Ricordiamo, come abbiamo detto in Conferenza dei Capigruppo su stimolo arrivato dai colleghi di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, che, visto che la settimana prossima andremo a votare lo

quantomeno si può ragionare; invece si dice - sempre a parole - che si vuole la collaborazione dell'opposizione, ma poi, nei fatti, purtroppo notiamo, come abbiamo visto anche ieri dalla Conferenza dei Capigruppo,

ricordo di avere proposto formalmente nella Conferenza dei Capigruppo di ieri che, prima dell'esame dello scostamento di bilancio, ci fosse una sessione in cui

che, prima dell'esame della proposta di scostamento dal pareggio di bilancio, si svolgano le comunicazioni del Presidente del Consiglio, durante le quali naturalmente si potranno presentare delle proposte di risoluzione, a proposito degli indirizzi della politica economica

intervengo giusto per lasciare anche una voce da parte della maggioranza rispetto alle dichiarazioni dei senatori Romeo e Malan che mi hanno preceduto. Il calendario dei lavori della prossima settimana (abbiamo stabilito anche quello di questa settimana) è abbastanza denso.

chiesto di avere un tempo sufficiente per poter affrontare la questione del senatore Salvini. Un'accelerazione dei tempi - secondo noi - era inopportuna oltre che sconveniente dal punto di vista politico, perché si tratta comunque di discutere di di una questione molto delicata che riguarda l'attività politica e la libertà di espressione, di pensiero e di azione di un Ministro della Repubblica, che richiede più tempo non per essere rinviata all'infinito, ma per essere esaminata. Ribadisco anche qui in Aula quello che ho detto nella Conferenza dei Capigruppo riguardo allo scostamento di bilancio. Il ministro D'Incà ieri ha riferito - cosa che peraltro avevamo anche letto sui giornali - che il Governo ha intenzione di proporre uno scostamento quantificabile

abbiamo votato a scatola chiusa, affidando poi al Governo il compito di distribuire le risorse. Il bilancio di questo atto di fiducia è per noi estremamente negativo. Quindi, questa volta chiediamo semplicemente al Governo e alla maggioranza di dirci prima come intenda utilizzare i 15-20 miliardi di scostamento che il Senato e la Camera dei Deputati dovranno votare da qui a pochi giorni. Non ci pare una richiesta strana, stravagante o lunare. Ci pare una richiesta di responsabilità, di condivisione delle responsabilità in un momento drammatico per la vita del Paese. Spesso il Presidente del Consiglio ci ha accusati di non voler dialogare con lui. Noi ribaltiamo questa logica: gli offriamo la possibilità di dialogare sullo scostamento, sulle cifre ipotizzate. Vogliamo semplicemente conoscere almeno le macrovoci su cui il Governo intende agire per spendere i 20 miliardi o quanti saranno, che faranno ballare alla fine lo scostamento complessivo rispetto ai piani al Governo per circa 100 miliardi di euro. quindi, è un atto politico. Le risposte non possono essere di ordine regolamentare, come abbiamo sentito ieri dal Ministro, e ci aspettiamo una risposta politica. Poiché *intelligenti pauca*, attendiamo dal Governo, della maggioranza, da un Ministro, una risposta su questa richiesta semplice, chiara e trasparente.

per l'Europa intera. In un momento di grave crisi sanitaria ed economica, l'Europa dimostra, pur nelle differenze che abbiamo seguito negli ultimi giorni, il suo volto solidaristico di sostegno e di aiuto alla crisi più nera dal Dopoguerra ad oggi, lasciando anche intravedere un embrione di bilancio federale dell'Unione.

concentriamoci sulle opportunità che le risorse portano con sé. Il nostro sistema Paese tutto deve dimostrare, *in primis* a se stesso, ai suoi concittadini e poi alla Comunità europea, che intende risollevarsi, ponendo al centro crescita, istruzione, sanità e lavoro. Eh già, il lavoro: è nel quadro del *post* Accordo di Bruxelles che vanno ricentrate le nostre politiche, per prendere linfa in un rinnovato percorso europeo. europeo. La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Sostegno all'occupazione giovanile - Un ponte verso il lavoro per la prossima generazione» del 1° luglio 2020 è stata anticipatrice dell'Accordo di questi giorni. Ma per stabilire le nostre politiche bene, presto e senza contraddizioni, il lavoro dei giovani va inserito in un orizzonte di senso. Se il lavoro è una parte preponderante della vita umana, un nostro tratto identitario che ci definisce come persone, questa condizione antropologica è ancora più veritiera per i giovani, che devono costruire il proprio futuro nella consapevolezza che il lavoro cambia la realtà, crea nuove idee, produce e trasforma le persone. Il lavoro è relazione degli altri con gli altri, è servizio, ha un impatto sociale, cambia il mondo, lo cambia da dentro e, se viene fatto bene, lo cambia in meglio. Per questo noi diciamo: lavoro e meno sussidi. Per l'amore dell'Italia e dei nostri figli, proponiamo di impegnarci su dodici priorità.

verde. Accanto a questo piano dobbiamo mettere un piano per la formazione, l'orientamento e la valorizzazione delle competenze dei giovani e l'occupazione giovanile.

più di quello che stiamo facendo - sul diritto allo studio e la riduzione delle tasse universitarie. Dobbiamo incrementare gli istituti tecnici superiori (ITS), ma non basta; basta; allo stesso tempo dobbiamo prevedere anche piani per la formazione, con esperienza di enti formativi che realizzano percorsi professionalizzanti brevi (*vocational master*). Ci sono delle

con la cassa integrazione così come l'abbiamo conosciuta. Gli ammortizzatori sociali devono avere in sé tre questioni: accompagnamento alla pensione, piano di formazione e ricambio generazionale.

da predisporre un progetto per l'imprenditorialità giovanile, compresa l'imprenditorialità sociale: ci sono in giro tantissime esperienze e la politica deve sostenerle.

Chiudo dicendo che ieri sera rileggevo alcune parole di Tina Anselmi, la quale affermava che nei momenti particolari il Parlamento, negli anni precedenti ai nostri, ha avuto il coraggio di fermare gli orologi per addivenire a soluzioni, come nel caso della legge sulla maternità. Noi pensiamo sulla maternità. Noi pensiamo che con queste mozioni prossimamente noi dovremo fermare gli orologi delle istituzioni per il bene del Paese, per un sistema economico e sociale giusto, che metta al centro il lavoro dei giovani.

Signor Presidente, la Carta costituzionale riconosce il lavoro come principio fondamentale della Repubblica italiana; particolare, attraverso la promozione del lavoro, diritto e dovere, si realizza la democrazia sostanziale, fondata su un'idea di eguaglianza e di libertà. libertà. Nella visione dei Padri costituenti, una persona che non ha lavoro non solo non può aspirare a una vita degna

ha creato un enorme buco nell'economia italiana. Secondo le previsioni che conosciamo tutti, abbiamo un calo complessivo previsto del 9,5 per cento nel corrente anno, e questo è il peggior risultato dalla Seconda guerra mondiale. Un primo effetto della pandemia - come abbiamo visto - si ripercuote sui numeri del lavoro, che hanno cominciato a peggiorare in maniera forte già da marzo, in una spirale che non vediamo accennare ad arrestarsi.

Anche se pensiamo al futuro, le previsioni non sono certo confortanti se si pensa, una volta finito il blocco dei licenziamenti,

a proseguire la propria attività produttiva, mantenendo intatta la forza lavoro impiegata. Dobbiamo premiare in particolare tutte quelle aziende virtuose

prevedendo iniziative normative volte alla riduzione del carico fiscale sui datori di lavoro che abbiano scelto o scelgano di non ricorrere alla cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali; sociali; 2) a prevedere proposte di sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, mantengono almeno l'80 per cento dei livelli occupazionali dei giovani lavoratori in forza alla data del 1° febbraio febbraio 2020, un incentivo, sotto forma di esonero dal 40 per cento del versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi.

parlare - permettetemi un piccolo pensiero - degli invisibili del mondo del lavoro, dimenticati anche nei decreti del Governo in carica, ossia gli stagionali e i precari, la parte fragile del lavoro; persone che si sono trovate in difficoltà economica, sociale e culturale. Gli stagionali

Anche il fallimento del *turnover* nella pubblica amministrazione ha dimostrato quanto questo Governo sia frenato. E ciò comporta anche un invecchiamento del mondo del lavoro nella pubblica amministrazione. Non ci sono più i *know-how* competitivi

Tutti sono lasciati a loro stessi: lavorano H24, ma non lavorano per nulla con questo metodo. Bisogna avere il coraggio di riscrivere le regole. Non mi voglio dilungare, perché tutti conosciamo la situazione dell'occupazione giovanile o, meglio, della disoccupazione giovanile e dell'immigrazione. Noi stiamo sostituendo con un'immigrazione incontrollata e non qualificata i giovani italiani, ma questo non è possibile e non è più

La grave crisi socio-economica che stiamo vivendo ha aggravato ulteriormente quella che è da anni una piaga del nostro Paese e per la quale, già prima dell'emergenza Covid, eravamo agli ultimi posti in Europa: la disoccupazione. Il dato Il dato più amaro riguarda la disoccupazione giovanile, che una recente indagine della Commissione europea rileva essere il più alto rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea, tra l'altro con una disparità di genere notevole. In Europa siamo agli ultimi posti per l'occupazione giovanile, ma siamo primi per il numero di Neet, con il 29,7 per cento a fronte di una media europea del 16,6 È molto alto e preoccupante il *gap* tra l'Italia e l'Europa riguardo all'abbandono scolastico: tre punti sopra la media. Nel 2018 sono stati 598.000 i ragazzi che hanno abbandonato precocemente la scuola. numeri che fanno paura per la grave perdita di risorse umane ed economiche, ma soprattutto per il disagio sociale che le centinaia di migliaia di ragazzi che abbandonano la scuola si trovano a vivere. Ora non c'è più tempo da perdere. Il Covid-19 ha accelerato un processo avviato verso la deflagrazione. Il problema della disoccupazione tra i giovani non può più essere rimandato e va affrontato in tutti i suoi molteplici aspetti, a partire dalla scuola, che deve saper coinvolgere tutti i ragazzi e seguirli in un percorso formativo adeguato non solo alle loro predisposizioni, ma anche alle richieste del mercato del lavoro. La scuola deve saper intercettare le esigenze contemporanee, ma soprattutto le professionalità future. Il Governo deve investire efficacemente per eliminare il degrado di molte zone del nostro Paese e permettere ai ragazzi di affrancarsi da quelle situazioni socio-culturali che impediscono e impoveriscono il loro percorso scolastico; utilizzare in modo proficuo i fondi europei (l'esistente Fondo sociale europeo e ora anche il *recovery fund*), perché le risorse messe a disposizione dall'Europa ci sono, ma bisogna essere in grado di intercettarle - purtroppo non è sempre stato così - con progetti e riforme per utilizzarle. A tal proposito, ci chiediamo che fine ha fatto SURE. È pur vero che si tratta di prestito, ma metterebbe a disposizione 20 miliardi per gli ammortizzatori sociali, con l'obbligo, però, ai lavoratori in cassa integrazione di fare formazione, che è importantissima. (*Applausi*). Infatti, pure a fronte di una disoccupazione giovanile del 25 per cento, le imprese faticano a reperire personale con competenze specializzate. Occorre prevedere, quindi, a livello scolastico orientamenti e informazioni atti a soddisfare richieste di imprese che ricercano specializzazioni altamente tecnologiche e digitali.

È assurdo: oggi non si riesce a soddisfare circa il 40 per cento delle domande per professioni specializzate, nonostante l'enorme disoccupazione giovanile. La vera riforma del lavoro passa attraverso la formazione: la scuola deve diventare vera preparazione alle professioni, incrementando i percorsi con le competenze trasversali e per l'orientamento e, quindi, la valutazione dei fabbisogni. Dall'altro lato, occorre impedire la cosiddetta fuga dei cervelli, dettata da molteplici motivi, tra cui la non valorizzazione delle professionalità, la bassa retribuzione, l'alta fiscalità, la difficile ascesa nei livelli professionali. Il percorso universitario deve essere competitivo rispetto agli altri Paesi europei, permettendo anche agli studenti di seguire con una tempistica più snella i praticantati, laddove durante i corsi di studio; di ottenere agevolazioni a chi frequenta specializzazioni fuori Regione, soprattutto per alcune materie. Anche Anche se nel decreto rilancio è previsto un ulteriore incremento delle risorse destinate a finanziare l'aumento del numero dei contratti di formazione medico-specialistica, questo, però, costituisce un incentivo non sufficiente per trattenere i giovani in Italia, ma solo per cercare di colmare le lacune del Sistema sanitario nazionale. Resta, tuttavia, da risolvere il cosiddetto imbuto formativo, che comporta la permanenza di tanti giovani laureati in situazioni di precariato, inoccupazione o disoccupazione. Il Governo deve anche intervenire con misure più a breve termine, con provvedimenti che rendano snelle e flessibili le assunzioni. In un momento storico, in cui purtroppo ai datori di lavoro manca la possibilità di eseguire una qualsiasi programmazione,

Le politiche attuate per incrementare il lavoro giovanile devono assumere una veste strutturale e organica. Non basta prevedere una decontribuzione per l'assunzione dei giovani *under* 35 di anno in anno. I provvedimenti devono potersi rinnovare automaticamente ogni anno e devono poter essere applicati anche ai contratti a tempo determinato. Non siamo solo noi a chiederlo; ce l'ha chiesto anche il Consiglio del nazionale dei giovani perché poi, magari, possono essere convertiti

delle imposte per l'avvio di nuove imprese da parte degli *under* 30 e la stipula con appositi provvedimenti di convenzione con gli ordini professionali. Norme certe e continuative: si devono dare le certezze sia alle imprese sia ai lavoratori dipendenti. Non si possono dare regole che vengono continuamente cambiate, pena la perdita di fiducia da parte degli imprenditori italiani e la fuga da parte degli investitori esteri. I giovani più che mai hanno bisogno di certezze per il loro futuro, e, se non le trovano qui, sempre più le cercheranno altrove. È un fenomeno, questo, che deve essere limitato al più presto. Viceversa, il calo della natalità e l'emigrazione all'estero di tantissimi giovani determineranno un gravissimo vuoto professionale e previdenziale. Il reddito di cittadinanza ha fallito. Le misure assistenzialistiche devono essere sostituite subito con investimenti per il lavoro e a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici che si trovano spesso - troppo spesso - in difficoltà per la conciliazione vita-lavoro. In un momento storico in cui l'ascensore sociale viene meno, il Governo ha il dovere di impegnarsi in maniera efficace per permettere ai giovani italiani di crearsi un futuro qui e non altrove, con le competenze adeguate, ma anche con una valorizzazione adeguata: sogno che viene, però, stroncato quando si sentono frasi demolitorie del sistema imprenditoriale da parte di alcuni Sottosegretari, e - peggio - un sogno che si infrange sul nascere con un Ministro dell'istruzione che sta distruggendo il nostro sistema scolastico, perno della crescita non solo personale ma di tutto il Paese.

il lavoro dei giovani va messo in un orizzonte di senso. Se il lavoro è una parte preponderante della vita umana, un tratto identitario che ci definisce come persone, questa condizione antropologica è ancora più veritiera per i giovani che devono costruire il proprio futuro, nella consapevolezza che il lavoro cambia la realtà, crea nuove idee, produce, trasforma la natura e le persone. Il lavoro è relazione con gli altri, è servizio, ha un impatto sociale; cambia il mondo, lo cambia dal di dentro e, se viene fatto bene, lo cambia in meglio. Il lavoro impronta l'esistenza e, dunque, al centro delle politiche deve esserci il lavoro e non i sussidi e l'assistenzialismo, soprattutto per le giovani generazioni. L'emergenza sanitaria si è immediatamente trasformata in emergenza economica. Tutti gli indicatori e le previsioni degli osservatori istituzionali dicono che, nonostante la ripresa graduale delle attività economiche, l'Italia e il mondo intero si stanno addentrando in un periodo di recessione economica davvero molto grave e senza precedenti. La pandemia in Europa provocherà un aumento dei disoccupati e, secondo una nota dell'Organizzazione internazionale del lavoro, i giovani sono stati già colpiti in proporzione estremamente più marcata. Dall'inizio della crisi, uno su sei ha smesso di lavorare. Molti giovani, infatti, lavorano in settori particolarmente colpiti, come quelli del turismo, della ristorazione, delle arti, dell'intrattenimento, del commercio all'ingrosso e del commercio al dettaglio, mentre altri stanno cercando di entrare nel mercato del lavoro proprio ora; ora che tali settori non sono più in grado di assumere, in un momento in cui, in generale, le prospettive economiche negative impediscono nuove assunzioni. I giovani avranno quella che già viene definita quest'anno come un'estate del nulla, in cui non potranno più approfittare della pausa estiva per accumulare esperienza extra universitaria, e non avranno la possibilità di migliorare i *curricula* per l'ingresso nel mercato del lavoro. L'emergenza Covid-19 ha spazzato via il tempo della semina e ha portato alla sospensione o alla completa cancellazione di tirocini, eventi e scambi internazionali. Particolarmente colpiti sono stati l'apprendimento basato sul lavoro e gli apprendistati, che sono incentrati sulla formazione e pratica e direttamente collegati al luogo di lavoro. Con la chiusura delle scuole e dei centri di formazione e l'apprendimento a distanza, l'istruzione e la formazione, che solitamente contribuiscono a correggere le distorsioni della nostra società, hanno potuto fare ben poco per combattere la povertà giovanile e l'esclusione sociale. Già prima della pandemia l'Italia soffriva particolarmente per fenomeni quali un elevato tasso di disoccupati giovanili e un alto numero di NEET (cioè quei giovani che non sono impegnati né nello studio, né nel lavoro, né nella formazione) e di ragazze e di ragazzi sottopagati, al primo impiego

non si possono guardare i giovani come categoria debole ma è necessario mettere nelle loro mani il futuro con politiche adeguate; per farlo, si devono anzitutto considerare le differenze tra i giovani per politiche mirate,

e le giovani lavoratrici con l'esigenza di costruire i propri percorsi lavorativi in rapporto alla famiglia e alle scelte di genitorialità; valutato che: la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni recante "Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione", del 1° luglio 2020, afferma che è il momento che gli Stati membri e le istituzioni europee rivolgono la loro attenzione verso la prossima generazione; le azioni che si immaginano sono: rafforzare la garanzia per i giovani e quella relativa all'istruzione e formazione professionale per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza insieme a un nuovo impulso agli apprendistati e che contribuiranno a creare occupazione giovanile. La comunicazione presenta inoltre ulteriori misure per il conseguimento di tale obiettivo; le proposte della Commissione per la Next Generation Eu e il futuro del bilancio UE consentiranno finanziamenti significativi a favore dell'occupazione giovanile; spetta ora agli Stati membri stabilire le priorità di investimento, dato che l'occupazione giovanile è principalmente di loro competenza; Da anni l'organizzazione internazionale del lavoro si batte per garantire che tutti gli uomini e tutte le donne abbiano accesso ad un lavoro produttivo e ad un lavoro dignitoso. Per questi motivi, Italia Viva ha deciso di presentare questa mozione, per chiedere al Governo: di definire e approvare un grande piano industriale di investimenti in digitale e di transizione in economia verde, al quale sia connesso, quale parte essenziale ed integrante, un piano per la formazione e la valorizzazione delle competenze dei giovani e l'occupazione giovanile; di rafforzare l'azione di Governo già in corso al fine di provvedere al riassetto dei vari istituti connessi alla formazione e riqualificazione professionale, con una disciplina di sistema per un vero sistema duale formazione-lavoro, che abbia, nelle principali esperienze europee comparabili, significativi riferimenti culturali e legislativi; di istituire un piano per l'integrazione della cultura digitale quale insegnamento fondamentale presso tutti i cicli di istruzione superiore secondaria, per l'acquisizione, da parte dei giovanissimi, di una *forma mentis* e di una capacità di discernimento utili per un mondo nuovo; di adottare misure di sostegno per gli studenti universitari e le loro famiglie, promuovendo il diritto allo studio e la riduzione delle tasse, a cominciare dall'immatricolazione. di incrementare e rafforzare gli istituti tecnici superiori e di effettuare il contestuale coordinamento dei piani per la formazione, con l'esperienza degli enti formativi, che realizzano nei territori percorsi professionalizzanti brevi, che nascono dal continuo dialogo con le aziende e che consentono di rispondere in tempi rapidi all'esigenza di competenze delle aziende. E, ancora,

a predisporre uno specifico investimento sui giovani professionisti che scelgono di restare in Italia, con un accesso alle professioni che sia semplice e a predisporre le misure affinché tale lavoro sia congruamente retribuito, evitando forme di sfruttamento; a rafforzare l'azione di governo già in atto al fine di continuare il confronto con le parti sociali per definire una normativa unitaria a partire dalla tutela del lavoro sulle piattaforme digitali; a predisporre un grande progetto per l'imprenditorialità giovanile, compresa l'imprenditorialità sociale, concentrandosi, tra l'altro, su istruzione e formazione all'imprenditorialità, servizi di consulenza, *mentoring* o *coaching* per i giovani;

che in questi giorni, fino alla fine del mese, i contribuenti italiani dovranno affrontare l'ingorgo fiscale più grande della storia, che conta 246 scadenze fiscali a carico dei lavoratori autonomi e 115 a carico di commercianti, artigiani e anche degli imprenditori più piccoli. Italia Viva ha chiesto più volte al Governo, anche con l'intervento del presidente del Gruppo Davide Faraone, di prorogare le scadenze fiscali di luglio; senza questo intervento le nostre imprese non saranno in grado di progettare il proprio futuro, né tantomeno quello dei giovani. Più soldi liquidi, più investimenti si traducono in assunzioni. Non credo Non credo sia difficile capirlo: è un'equazione facile. Speriamo che il Governo si ravveda e faciliti la creazione di posti di lavoro, rinunciando a soldi che potrebbe incassare ugualmente a fine anno. *(Applausi)*.

guardano al futuro, vorrebbero impegnare il Governo a evitare gli errori del passato (e anche quelli del presente), per garantire alle nuove generazioni quanto necessario per poter mettere le proprie radici nel nostro Paese. Le cause del divario generazionale, sappiamo, sono molteplici; tra queste va sicuramente annoverata la persistente difficoltà tra gli *under* 35 di trovare un lavoro, come testimonia il loro basso tasso di occupazione. Inoltre, quando i giovani lavorano sono spesso sottooccupati o lo fanno *part-time* anche quando vorrebbero farlo a tempo pieno. A questo si aggiunge la forte precarizzazione del mercato del lavoro italiano, che non si è affatto risolta con il decreto dignità, anzi, direi che si è complicata, e i bassi salari, che penalizzano soprattutto i giovani. Non si tratta comunque solo di disoccupazione, ma proprio di una mancanza strutturale di opportunità di una grave carenza nella formazione, come segnalano imprenditori che vorrebbero assumere giovani, ma che non ne trovano formati per il compito che li dovrebbe attendere. Non oso pensare, certamente con il caos del prossimo anno scolastico, come si potrà pensare alla formazione organizzata da un Ministro totalmente incompetente. In altri Paesi la politica si è già resa conto di questo problema e tende a improntare le politiche economiche e sociali sulle reali necessità dei giovani, visti come una risorsa del loro Paese. Questo comporta maggiore attenzione e risorse per educazione, formazione, ricerca, inserimento nel mercato del lavoro e per le famiglie giovani con bambini. Quali sono le politiche economiche e sociali che l'Italia potrebbe adottare per far fronte a questo problema? La prima cosa è far ripartire l'economia: senza una maggiore crescita, i redditi delle giovani generazioni e di quelle future sono destinati a stagnare e il presente divario generazionale non potrà essere colmato o tenderà ad aumentare ancora. Le politiche economiche e sociali devono tenere maggiormente maggiormente presenti le esigenze dei giovani. L'ultimo rapporto OCSE sull'Italia fornisce dati agghiaccianti e vediamo raccomandazioni molto forti a tale riguardo: in primo luogo, taglio dei contributi sociali a carico delle imprese per i salari medi e bassi, che favorirà occupazione e crescita economica; in secondo luogo, una vera riforma delle politiche attive del lavoro unita a una riforma dell'apprendistato e corsi professionali che facilitino l'inserimento nel mondo del lavoro o in percorsi educativi per i giovani che attualmente sono esclusi dalla società, in quanto non studiano e non lavorano.

dal momento che oltre l'80 per cento dei diplomati troverebbe occupazione al termine degli studi, se ci fossero percorsi formativi professionalizzanti. Penso alle tradizioni tipiche dell'Italia (la falegnameria, la moda e la lavorazione del vetro, del ferro battuto e del cuoio), tutte realtà che meritano di ritrovare la loro valorizzazione anche in virtù del fatto che il nostro Paese non può più permettersi di perdere queste eccellenze, invidiate nel mondo e purtroppo tante volte copiate e vendute in maniera contraffatta. Riscoprire la bellezza del lavoro manuale non vuol dire abbandonare la tecnologia, ma anzi, rendere più attrattivo il nostro Paese, che ha sempre avuto una vocazione per i settori dell'agricoltura e della manifattura. Occorre dunque investire nella formazione attraverso riforme che puntino sui programmi scolastici (ahimè, non finiremo mai di ricordarvelo). L'Italia su questo, ma in generale nella scuola investe ancora poco se paragonata agli altri Paesi sviluppati. Non intendiamo certo la formazione in stile *navigator* assunti per assistere i percettori di reddito di cittadinanza, una follia:

i *navigator* hanno pure percepito l'indennità da 600 euro per marzo e aprile prevista dall'emergenza coronavirus, anche se hanno continuato a prendere regolarmente lo stipendio, nonostante i centri per l'impiego siano stati chiusi. *(Applausi).* Vergogna! C'è gente che aspetta ancora integrazione! Ma voi li sentite? Nella ristorazione non hanno ancora preso la cassa integrazione e a giugno hanno ricevuto quella di marzo; ovunque si sente, anche nelle aziende:

Nella nostra mozione chiediamo tra l'altro al Governo di risolvere in via strutturare il problema del cosiddetto imbuto formativo, affinché a ciascun laureato in medicina corrisponda un percorso formativo post laurea, per assicurare ai cittadini un'assistenza di qualità e immettere nel sistema un congruo numero di specialisti e medici di medicina generale. Sappiamo infatti che le borse di studio per le scuole di specializzazione, seppur incrementate, non permettono a tutti i laureati in medicina di avere un futuro da specialisti nel nostro Paese.

perché, dopo il decreto ministeriale che permette l'abilitazione, i medici saranno molti di più, quindi i posti non bastano per questi primi due anni. Bisogna dare un aiuto concreto alle mamme e alle donne attraverso l'incremento del *welfare* aziendale, come fanno ad esempio tante aziende private dalle quali il pubblico potrebbe prendere esempio. Parliamo tanto di carenza di natalità nel nostro Paese, ma non facciamo niente di concreto: qualche parola c'è stata. i campanelli d'allarme sono ormai campane che non smettono di suonare e il tempo di fare cose serie è già scaduto, come scadono anche le scatolette di tonno, nonostante purtroppo abbiano una lunga conservazione. È come la voglia degli italiani di sentirsi ripetere ogni giorno che presto tutto cambierà e che questo Governo andrà a casa. Il lavoro e i nostri giovani hanno la priorità. Non sprecate anche questa grande occasione in cui Forza Italia vi concede

come saranno utilizzati questi soldi, perché è vero che si dovranno comprare i banchi ergonomici - o forse faremo anche i banchi monopattino, non lo so - ma magari non sarebbe male presentare un piano d'investimento, visto che passerà solo se lo votiamo noi Noi abbiamo a cuore l'Italia. Non accogliendo queste proposte, voi andrete ancora una volta contro la volontà di questo Paese e della maggioranza dei cittadini che vogliono, prima di tutto, lavorare e vivere serenamente. *(Applausi)*.

Nonostante tutti i Governi si impegnino (ma a parole) per risolvere il grave problema degli alti tassi di disoccupazione che caratterizzano il mercato del lavoro soprattutto per i più giovani, all'atto pratico si fa veramente poco. Come ha avuto modo di evidenziare il collega De Vecchis, l'Istat ci segnala che tra il 2009 e il 2018 circa 320.000 giovani giovani di età compresa tra i venti e i trentaquattro anni hanno lasciato il nostro Paese, non per una scelta di vita magari legata a fattori familiari o affettivi, ma proprio perché questi ragazzi non hanno la possibilità di trovare un impiego che valorizzi gli studi fatti, che gratifichi l'impegno che mettono nella loro attività professionale, che consenta di avere un reddito sufficiente per vivere in modo dignitoso senza dipendere dai genitori. I giovani fuggono e l'Italia non perde solo delle persone, ma anche delle risorse che potrebbe valorizzare. Si parla in proposito di un costo di circa 16 miliardi di euro, oltre un punto percentuale di PIL, un tesoro che i nostri giovani finiscono di riversare su altri Paesi più lungimiranti del nostro. Cosa fa il nostro Paese per i giovani? Si limita purtroppo all'assistenzialismo, umiliando i nostri ragazzi ricchi di risorse, che hanno conseguito titoli di studio importanti, con grandi sacrifici da parte delle famiglie, e non chiedono un sussidio: vogliono lavorare, produrre, far crescere il Paese, migliorarlo, arricchirlo. Sappiamo che il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, ha istituito il reddito di cittadinanza quale misura di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza, all'esclusione sociale. L'obiettivo del legislatore era nobile: garantire un reddito ai non abbienti, ma creando al contempo i presupposti affinché questo reddito fosse impiegato per consentire agli interessati di trovare un lavoro. di trovare un lavoro. Il MoVimento 5 Stelle, il principale sostenitore di questo istituto, dichiarava a gran voce che doveva figurare non tanto come strumento di politica assistenziale, quanto piuttosto come strumento di politica attiva del lavoro.

che il reddito di cittadinanza era una misura proattiva collegata all'inserimento nel contesto sociale e lavorativo del cittadino. Infatti, l'erogazione del reddito è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che prevede attività di servizio della comunità. Tutti obiettivi condivisibili. Coloro che beneficiano del reddito sono quindi tenuti a sottoscrivere presso i centri per l'impiego un patto per il lavoro o, qualora ricorrano i presupposti, un patto per l'inclusione sociale, in ragione dei quali devono assicurare la propria disponibilità alla partecipazione a progetti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo o di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo Comune di residenza, mettendo a disposizione non meno di otto ore settimanali, aumentabili fino a un massimo di sedici. Quali sono stati i risultati conseguiti dopo un anno e mezzo di sperimentazione? i dati dell'osservatorio sul reddito di cittadinanza e di ANPAL testimoniano il fallimento completo di tale politica. L'osservatorio riferisce che nel 2019 la misura ha coinvolto 968.645 nuclei familiari e 2.540.575 persone, per un importo medio mensile pari a 527 euro, mentre nel 2020 ha coinvolto rispettivamente 1.057.319 nuclei e 2.721.036 persone, per un importo medio mensile di 568 euro. La nota mensile del 29 maggio 2020 pubblicata da ANPAL ci riferisce che alla data del 1° aprile 2020 il numero complessivo di beneficiari del reddito di cittadinanza presenti nel *data base* ANPAL è appena superiore a 990.000 individui, dei quali solo 800.000 sono soggetti a patto per il lavoro e appena 365.000 sono presi in carico dai servizi per l'impiego. La stessa ANPAL riferisce che, alla data del 10 febbraio 2019, i beneficiari che hanno iniziato un rapporto di lavoro dopo l'approvazione della domanda sono

In pratica, l'Agenzia nazionale che si occupa di politiche attive del lavoro, che dovrebbe quindi operare per favorire l'occupazione, l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, ci dice che meno del 2 per cento di coloro che hanno percepito il reddito di cittadinanza ha poi ottenuto un impiego quasi tutti quelli che hanno avuto un contratto di lavoro hanno ottenuto il tempo determinato. Persino la Corte dei conti, nella relazione sul rendiconto generale del 2019, ha bocciato il reddito di cittadinanza, rilevando che a fronte di un costo di quasi quattro miliardi di euro, solo il 2 per cento dei beneficiari ha poi ottenuto un lavoro attraverso l'intermediazione dei centri per l'impiego. Colleghi, ne valeva davvero la pena? A conti fatti, l'Italia ha investito moltissime risorse, ma non è stata in grado di andare oltre le mere politiche assistenziali. Ha erogato sussidi, ma non ha dato lavoro e quando il lavoro c'è è a tempo determinato. Non sarebbe quindi opportuno rivedere queste politiche del lavoro, adottare iniziative affinché l'erogazione del reddito di cittadinanza non si traduca in una mera attività di assistenzialismo, ma sia funzionale a consentire la partecipazione dei cittadini al mercato del lavoro? Ecco perché, come Gruppo della Lega, abbiamo deciso di presentare una mozione che impegni il Governo ad adottare un piano strutturato ed organico che non si limiti a dare sussidi, ma valorizzi i giovani attraverso serie politiche attive del lavoro, incrementando l'offerta di lavoro in modo particolare per i giovani aumentando il tasso di occupazione giovanile per fare in modo che i nostri ragazzi siano sempre più incentivati a restare in Italia, a far crescere e migliorare il nostro Paese, anziché andare a cercare fortuna altrove.

sul punto 5 con la seguente riformulazione: «ad assumere iniziative di competenza al fine di effettuare il contestuale coordinamento dei piani per la formazione con l'esperienza degli enti formativi che realizzano nei territori percorsi professionalizzanti brevi, *vocational master*, che nascono dal continuo dialogo con le aziende e che consentono di rispondere in tempi rapidi all'esigenza di competenze delle aziende». Il parere è favorevole sul punto 6. Sul punto 7 il parere è favorevole con la seguente riformulazione: «ad incrementare il Fondo nazionale del servizio civile per dare sostanza all'universalità prevista dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e consentire a tutti i giovani che volessero fare questa esperienza (circa 85.000 nel 2019) di poterla realizzare». Il parere

punto 12 con la seguente riformulazione: «a promuovere nuove specifiche misure per il sostegno e l'incentivazione del lavoro dei giovani nell'ambito della ricerca accademica e applicata».

che, dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, mantengono almeno l'80 per cento dei livelli occupazionali dei giovani lavoratori in forza alla data del 1° febbraio 2020, un incentivo, sotto forma di esonero dal 40 per cento del versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi.

Sull'unico impegno il parere è favorevole con la seguente riformulazione: «ad intraprendere iniziative volte al rafforzamento delle politiche attive per il lavoro con il fine di incrementare l'offerta di lavoro, in modo particolare per i giovani, aumentare il tasso di occupazione giovanile, le entrate dell'erario in termini di contributi previdenziali e puntando verso la valorizzazione delle risorse umane prodotte dal nostro Paese». Quindi, a parte la riformulazione iniziale («ad intraprendere iniziative volte al rafforzamento»), c'è l'eliminazione delle parole: «tralasciando misure

Sull'impegno n. 2 il parere è favorevole con la seguente riformulazione: «a sostenere l'introduzione di forme di detassazione in favore delle *start up* innovative, anche mediante istituzione di un apposito fondo». n. 3 il parere è favorevole con la seguente riformulazione: «a sostenere l'adozione di provvedimenti» (il resto rimane identico). n. 4 il parere è favorevole con la seguente riformulazione: «a valutare la possibilità di adottare i necessari provvedimenti normativi affinché, d'intesa con gli ordini professionali, si possano rendere abilitanti i titoli universitari dei relativi corsi di laurea, anticipando all'interno di questi, se del caso, il tirocinio propedeutico all'abilitazione professionale». Peraltro assicuro che stiamo lavorando in questa direzione. Sull'impegno n. 5 il parere è favorevole. Sull'impegno n. 6 il parere è favorevole con la seguente riformulazione: «a valutare la possibilità di prevedere iniziative normative per l'erogazione di contributi a giovani italiani di età inferiore a 25 o 28 anni per la frequentazione, in un istituto ubicato in una Regione differente rispetto a quella di residenza, di corsi altamente qualificanti nelle materie ambientali, dell'agroalimentare, delle biotecnologie, dell'economia,

le riformulazioni proposte dal Sottosegretario sono abbastanza copiose, se c'è un atteggiamento concorde da parte di tutti i Gruppi propongo che alla ripresa, se qualcuno di noi ha delle osservazioni da fare o un chiarimento da chiedere, possa farlo in continuazione con l'intervento del Governo,

abbiamo mezz'ora di tempo, onde evitare che alle 16,30 si ricominci con una nuova interruzione.

una condivisione. Per me non ci sono problemi, però io in questo momento sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 12 con l'informativa del presidente Conte.

una nuova finestra"). L'ordine del giorno reca: «Informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sugli esiti del Consiglio europeo». Ricordo che è in corso la diretta televisiva con la RAI. Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio dei ministri, professor Conte.

ho ritenuto mio dovere essere qui oggi davanti a voi per riferire sugli esiti di un Consiglio europeo che ha assunto decisioni di portata storica e che, per il rilievo delle questioni trattate, si è prolungato ben oltre le aspettative iniziali. Si è trattato di un vertice straordinario anche in termini di complessità, in linea con l'elevata posta in gioco. Quello che nelle comunicazioni rese qui al Parlamento lo scorso 15 luglio consideravo un auspicio oggi è certezza. L'intesa raggiunta rappresenta senza dubbio un passaggio fondamentale, che ci spinge ad affermare, senza enfasi, che l'Europa è stata all'altezza della sua storia, della sua missione e del suo destino. L'Unione europea sta affrontando una crisi sanitaria, economica e sociale che si è manifestata sin dal suo più tragico esordio simmetrica e sistemica. Ha coinvolto tutti i Paesi; ha profondamente scosso la vita dei cittadini europei; ha inciso in misura significativa sulla società, sulle economie,

tramite l'emissione di titoli di debito autenticamente europei. In questo modo, si è realizzato ieri un un radicale mutamento di prospettiva: in passato si tendeva - non lo dimentichiamo - a intervenire nel segno del rigore, affidandosi a logiche di *austerity*,

che peraltro completa il quadro di molti altri interventi già assunti e adottati, è interamente orientato alla crescita economica e allo sviluppo sostenibile, nel segno in particolare della digitalizzazione e della transizione ecologica. Con la decisione di ieri il Consiglio ha abbracciato, quindi, una diversa prospettiva in favore di un'Europa più coesa, più inclusiva, più solidale, più vicina ai cittadini in definitiva, più politica e certamente più coerente con lo spirito originario del sogno europeo, quello di coloro che, dopo la tragedia della Seconda guerra mondiale, prefiguravano l'idea di un'unità fondata su una comunione di valori, di storia e di destino. È l'unico percorso possibile per preservare l'integrità dello stesso mercato unico e la stabilità stessa dell'Unione monetaria. Questo risultato positivo non era affatto scontato a marzo - lo ricordiamo tutti -quando l'Italia, insieme ad altri otto Stati membri, propose che il *recovery fund* affiancasse, con pari dignità politica ed economica, gli altri strumenti di risposta che erano già sul Come è noto, sin dall'inizio dell'emergenza del Covid-19, l'Italia ha subito messo in evidenza che la crisi nella quale l'intero continente era precipitato presentava caratteri di straordinaria gravità, assumendo i tratti di una recessione senza precedenti, peraltro sopraggiunta in un contesto macroeconomico già caratterizzato da elementi di profonda fragilità, acuito dall'inasprimento di persistenti squilibri sociali e territoriali. Già la proposta franco-tedesca del 18 maggio e la proposta della Commissione europea del 27 maggio per la creazione del pacchetto *next generation* EU e per l'elaborazione del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 erano animati da questa visione. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, nell'elaborare la proposta che ha fornito poi la base negoziale su cui si è avviato il confronto fra i Paesi membri, non si discostava nella sostanza da quei presupposti. Si è trattato di un'interlocuzione serrata, complessa, nel corso della quale si sono confrontate una pluralità di posizioni e di interessi. Un intenso impegno politico e diplomatico, nei giorni e nelle notti di negoziato in particolare - ma ovviamente il lavoro è iniziato ben prima

e *loan* (prestiti), passati da 250 a 360 miliardi di euro, a causa della visione anacronistica di pochi Stati membri.

È stata in tal modo confermata una risposta ambiziosa, adeguata alla posta in gioco, il funzionamento del mercato unico e il rilancio delle economie europee interdipendenti, in questa prospettiva abbiamo lavorato non soltanto - vedete - per tutelare la dignità del nostro Paese, per promuoverne il ruolo di primo piano in Europa, ma anche per salvaguardare le prerogative stesse delle istituzioni europee da alcuni tentativi ben insidiosi, emersi durante il negoziato, di snaturare l'essenza autenticamente comunitaria del programma *next generation* EU, contribuendo alla piena affermazione del principio di solidarietà. Devo confessare che ci sono stati dei momenti, durante la lunga fase dei negoziati, nei quali la rigidità delle differenti posizioni sembrava addirittura insuperabile. Anche in quei momenti più critici, tuttavia, continuava a maturare la sempre maggiore consapevolezza di un profondo senso di responsabilità verso i nostri popoli; non potevamo fallire, né accedere a un mediocre compromesso o addirittura rinviare la decisione. Per questo, con tenacia, con determinazione, abbiamo proseguito il confronto a oltranza fino all'alba di ieri. Possiamo dirci soddisfatti di un risultato positivo, che non appartiene ai singoli; non appartiene neanche a chi vi parla e al Governo e - se mi permettete - neppure alle forze di maggioranza: è un risultato che appartiene all'Italia intera.

Presidente. Non si possono fare foto in Aula; devo ripeterlo a ogni seduta. Senatrici Botto e Leone, vi prego di non usare la macchina fotografica, d'accordo? Non si può fare. Ormai dovremmo averlo imparato tutti. Mi scusi ancora, Presidente, ma non è possibile che ogni volta devo ricordare le regole.

tutti i Ministri, i quali non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno nel corso dell'intera durata del negoziato. Permettetemi di riservare una particolare menzione al ministro Amendola perché era con me a Bruxelles e ha condiviso le difficoltà che materialmente abbiamo incontrato. Mi sento davvero di ringraziare tutte le forze di maggioranza: avete sostenuto in modo compatto il Governo, l'azione del Governo, sulla base di una convinta condivisione di questo progetto. Grazie! Permettetemi di ringraziare anche quelle forze di opposizione che, pur nella diversità di posizioni, hanno compreso l'importanza di questo passaggio storico e i beni in gioco, nella prospettiva dell'interesse nazionale. Anche a voi, grazie! Possiamo riassumerlo: la classe politica italiana, nel suo complesso, ha dato una grande prova di maturità in quest'occasione. Infine, voglio ringraziare anche tutti i cittadini italiani, perché il loro comportamento, il loro sostegno, che ha portato a questo risultato, è iniziato già nei primi giorni della pandemia. di cui, primi fra tutti in Europa, i nostri cittadini hanno dato testimonianza, con il senso di comunità che hanno saputo esprimere in quei giorni, durante i quali ho avvertito forte il loro sostegno, essi hanno rafforzato oggettivamente la posizione, l'autorevolezza e la credibilità del Governo italiano al tavolo delle grandi decisioni. è anche grazie a loro che l'Italia è stata all'altezza della sfida e ha portato a casa questo importante risultato. Tutti dobbiamo esserne orgogliosi. L'Italia ottiene un risultato all'altezza delle aspettative, un esito - lo avete constatato - persino migliore rispetto all'iniziale proposta avanzata dalla Commissione europea per quanto concerne l'ammontare complessivo dei fondi destinati al nostro Paese. Nello schema attuale, l'Italia riceverà 209 miliardi di euro: il 28 per cento delle risorse totali previste dal *next generation* EU - è pari a 750 miliardi di euro. In particolare, resta fissato a 81 miliardi l'ammontare dei trasferimenti, i famosi *grant* destinati all'Italia, così come previsto dalla proposta della Commissione. Aumenta, invece, davvero in modo significativo, di circa 36 miliardi di euro, la componente dei prestiti disponibili, che arriva così alla ragguardevole cifra di 127 miliardi di euro. Tali risorse potranno essere impegnate fino al 31 dicembre 2023. Il 70 per cento di queste risorse sarà disponibile tra il 2021 e il 2022 e i relativi pagamenti legati allo svolgimento dei progetti definiti all'interno dei piani nazionali per la ripresa saranno disponibili fino alla fine del 2026, quando l'Unione interromperà l'emissione di titoli e inizierà il periodo di restituzione da parte degli Stati membri. Oltre alla componente principale di *next generation* EU, cioè la *recovery and resilience facility,* potenziata a 672,5 miliardi di euro dai 560 miliardi proposti proposti dalla Commissione europea, giocheranno un ruolo importante altri due strumenti: *invest* EU, con una dotazione complessiva di 8,4 miliardi di euro, che sosterrà gli investimenti privati - è un po' l'erede del piano Juncker per gli investimenti di cui, peraltro, l'Italia si è rivelata uno dei principali destinatari - e l'iniziativa *react* EU, con una dotazione complessiva di 47,5 miliardi di euro, grazie alla quale potranno essere proseguiti gli investimenti anti Covid a favore del sistema sanitario e a sostegno del reddito dei lavoratori e della liquidità delle imprese. Un altro risultato politicamente rilevante dell'intensa azione politica e diplomatica condotta, prima e durante il Consiglio europeo, insieme ad altri Stati membri e dal Presidente della Commissione europea e del Consiglio europeo, è che il meccanismo di *governance* di *next generation* EU preserva le competenze della Commissione europea sull'attuazione dei piani nazionali di ripresa e di resilienza. I piani saranno approvati dal Consiglio dell'Unione europea a maggioranza qualificata, come peraltro già avviene ordinariamente per i programmi nazionali di riforma del semestre europeo, mentre i singoli esborsi verranno decisi dalla Commissione, sentito il Consiglio. Anche il freno di emergenza eventualmente attivabile presso il Consiglio europeo avrà una durata massima di tre mesi e non potrà prevedere un diritto di veto. Sono stati, dunque, evitati i passaggi all'unanimità che avrebbero innescato derive pericolose sul piano sia giuridico, finendo per ledere le competenze della Commissione in materia di bilancio europeo, sia politico, perché avrebbero imprigionato lo strumento chiave della ripresa economica europea in veti incrociati tra Stati membri. Su questo punto l'Italia da subito ha definito la sua linea rossa.

su questo, poi, abbiamo agito con la massima determinazione, ottenendo che l'ultima formulazione - peraltro ben migliorata rispetto alle precedenti - fosse ulteriormente rinnovata.

in via del tutto eccezionale - con specifiche e motivate richieste che debbono addurre dei significativi inadempimenti

che richiamano la competenza della Commissione. Da ultimo, non paghi, abbiamo voluto che fosse rilasciata una *legal opinion*, un parere legale, da parte dell'ufficio legale della Presidenza del Consiglio europeo, da allegare agli atti. agli atti. Abbiamo evitato, in questo modo, che fossero compromessi i consolidati meccanismi decisionali delle istituzioni europee e, nello specifico, l'efficacia del programma *n**ext generation* EU. Il Consiglio europeo ha adottato una decisione adeguata alla posta in gioco anche per quanto riguarda i tempi. Era, infatti, fondamentale e indispensabile dare un segnale chiaro ai cittadini, alle imprese e agli stessi mercati finanziari: l'Europa risponde in modo tempestivo, ben determinato rispetto alla crisi. Al riguardo, segnalo che il 10 per cento delle risorse, sotto forma di trasferimenti del *recovery and resilience facility*, potrà essere anticipato come prefinanziamento del 2021. In secondo luogo, anche i progetti di investimento già avviati a partire dal 1° febbraio 2020 potranno beneficiare dei finanziamenti del pacchetto europeo, purché siano coerenti con gli obiettivi del programma. Nell'ambito di questo Consiglio europeo è stato anche approvato il bilancio settennale, il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che abitualmente, come sapete, richiede più sessioni. Il saldo italiano sul quadro finanziario pluriennale, pur restando negativo, migliora rispetto a quello attuale, 2014-2020, passando da meno 0,24 a meno 0,17 per cento del PIL (in termini assoluti, da meno 4,11 miliardi di euro a meno 2,9 miliardi di euro in media all'anno) ed è più che compensato dai rientri attesi dal *next generation* EU. Siamo inoltre uno dei pochi Stati membri che vede aumentare, rispetto al quadro finanziario pluriennale attuale, da 36,2 a 38 miliardi di euro le proprie dotazioni sulla politica di coesione, che invece è stata ridotta, per un totale di 37 miliardi, nei vari Stati membri. Si tratta - se mi permettete di sottolinearlo - di un risultato decisivo, perché la politica di coesione, tanto più in questa particolare congiuntura socio-economica, svolge un ruolo fondamentale a beneficio dei territori. Sempre in materia di coesione, è stata ottenuta maggiore flessibilità nell'uso dei fondi strutturali, grazie a obblighi di concentrazione tematica meno stringenti e disimpegni più lunghi, il che consente di orientare in modo più proficuo la spesa verso le esigenze specifiche delle diverse aree territoriali, anche in chiave di sostegno ai settori più colpiti dalla crisi da Covid-19. Quanto all'altrettanto fondamentale politica agricola comune, il rafforzamento delle dotazioni per lo sviluppo rurale (77,1 miliardi a valere sul quadro finanziario pluriennale e 7,5 miliardi su *next generation* EU) avvantaggia l'Italia, che ne ha ritorni elevati, oltre l'11 per cento del totale. Le conclusioni del Consiglio europeo straordinario in materia di quadro finanziario pluriennale hanno inoltre confermato l'impegno a introdurre nuove risorse proprie già a partire dal 2021, mentre - come aveva

Dal lato delle entrate, alcuni Paesi potranno beneficiare di un aumento degli sconti - lo avete anche sentito, è stato anticipato - rispetto alla quota di contribuzione del bilancio comunitario, di cui già potevano avvalersi nell'attuale quadro finanziario pluriennale. Sono i famosi *rebate*: è un elemento che abbiamo sempre dichiarato anacronistico, che ci è servito anche per contrastare ulteriori pretese ed esercitare un potere negoziale, su cui ogni nostra parziale flessibilità è stata comunque condizionata dall'esigenza prioritaria di garantire l'esito positivo del negoziato su *next generation* EU. Il Consiglio europeo ha trovato un punto di sintesi anche in materia di stato di diritto e di lotta al cambiamento climatico. Con riguardo allo stato di diritto, le conclusioni collegano il suo rispetto alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, in coerenza con quanto già contenuto nella proposta negoziale portata al tavolo dal presidente Michel. Quanto alla lotta al cambiamento climatico, è stato confermato che il 30 per cento della spesa europea sarà collegato al raggiungimento di quest'ambizioso obiettivo e la riduzione rispetto alla proposta iniziale della dotazione complessiva del *just transition fund*, che comunque ammonta a 10 miliardi di euro, non ha uno specifico impatto negativo sull'Italia. In via generale, occorre riconoscere che il fondo soffre purtroppo di un'impostazione disfunzionale, perché premia i Paesi che sin qui non si sono impegnati abbastanza nella transizione ecologica, trascurando la necessità di riconoscere gli sforzi di quegli Stati che, come l'Italia, hanno già intrapreso l'ineludibile percorso del *green deal.* Concludo, gentile Presidente, onorevoli senatrici e onorevoli senatori: all'esito del Consiglio conclusosi all'alba di ieri, siamo chiamati a profondere un forte e intenso impegno per far sì che il percorso riformatore avviato nelle scorse settimane trovi concreta e puntuale attuazione, innanzitutto con la predisposizione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza propedeutico all'accesso ai fondi europei di *next generation* EU. Di questo piano abbiamo già posto le basi, individuando gli obiettivi da perseguire nel corso della consultazione nazionale e progettiamo il rilancio. Dovremo impiegare in maniera efficiente le nuove risorse, indirizzandole a finanziare gli investimenti necessari per affrontare con successo le sfide del futuro. La crisi da Covid-19 ha reso evidenti alcune storiche criticità del nostro Paese. Questo Governo si assume la responsabilità di predisporre e realizzare tale piano con impegno, determinazione e lungimiranza, avendo consapevolezza che un futuro migliore per i cittadini, nonché - dobbiamo esserne consapevoli - la credibilità dell'Italia in Europa passeranno anche da qui, dal saper dimostrare di cogliere quest'opportunità storica, manifestando una capacità propositiva, decisionale e attuativa che non ceda a particolarismi. Sarebbe un errore epocale di cui non potremmo certo accusare l'Europa. Questi giorni di negoziato ci rafforzano nella convinzione che l'interesse nazionale oggi più che mai va perseguito all'interno del perimetro europeo. Visioni egoistiche, spesso ancorate alla difesa di anacronistici interessi, non offrono alcuna risposta efficace, se non quella di alimentare le paure dei cittadini e il distacco dalle istituzioni. Il piano per la ripresa sarà un lavoro collettivo, ci confronteremo con il Parlamento dobbiamo impegnarci assolutamente in questa direzione. Dobbiamo impegnarci anche per alimentare la fiducia nelle istituzioni italiane e nell'Europa. Con l'accordo raggiunto ieri al Consiglio europeo sembra realizzarsi l'auspicio espresso da Jacques Delors, da molti invocato lunedì 20, il giorno del suo compleanno, per un esito positivo del Consiglio europeo, quando ventisette il 10 febbraio 1993 dinanzi al Parlamento europeo affermò che era veramente giunto il momento di ricollocare il fiore della speranza al centro del giardino europeo.

(poi dirò qualcosa sui momenti di giubilo) per dire che siamo a valutare l'esito di un vertice europeo. Colleghi, vi confesso che questa mattina venendo in Senato mi è venuto in mente quello che mi diceva sempre Carlo Azeglio Ciampi, che è stato un grande Presidente della Repubblica, e con lui quanto dicevano sempre i grandi protagonisti della tradizione democratica cristiana di questo Paese,

che noi abbiamo avuto vicini e abbiamo avuto bisogno - e l'Europa ha avuto bisogno - della cancelliera Merkel e di Macron Ritengo pertanto che dobbiamo riconoscere, al di là dei Gruppi politici di appartenenza, che il ruolo dell'Italia è lavorare con Germania e Francia perché l'Europa possa andare avanti. La posta in palio in questo vertice non era solo la condizione con cui il Presidente del Consiglio sarebbe venuto qui dopo il mandato ricevuto dal Parlamento la scorsa settimana; era qualcosa di più.

si è affermato qualcosa di molto importante, cioè l'idea che l'Europa va avanti sullo spirito e l'idea di un'Europa comunitaria.

per come spenderemo i soldi non è un problema, perché questo controllo lo dovremmo rivendicare noi per i nostri figli. *(Applausi)*. Il tema non sono i controlli che vengono imposti agli Stati, ma

della visione comunitaria: gli Stati non prevarranno. Questo è l'elemento di fondo importante di questo vertice. Colleghi, ho apprezzato che il Presidente del Consiglio sia venuto qui e abbia detto che è un successo degli italiani. Sì, Presidente, ha ragione, è un successo degli italiani che noi dobbiamo anche alle migliaia di morti per il Covid-19, ai quali ci inchiniamo perché è giusto che sia così. bene i trionfalismi, colleghi, ma non abbiamo vinto la schedina del Totocalcio, non abbiamo vinto al Bingo, qui non c'è uno "zio d'America" che ci porta dei soldi: qui ci sono degli impegni che lo Stato andrà ad assumere e dei debiti che andrà a contrarre in sede europea e pertanto la nostra necessità non è quella oggi di fare dei trionfalismi,

di capire che oggi questa vicenda è stata condotta bene dal Governo italiano e io non ho alcuna difficoltà a dire che il Presidente del Consiglio ha dato una prova di resistenza, che è stata anche fisica. Quando vengono dei giovani e chiedono consigli su come fare politica, io dico sempre che bisogna avere resistenza fisica e lei ha dimostrato resistenza e tenacia; tenacia; l'avevamo già capito nel passaggio dal primo al secondo Governo Conte che lei aveva un po' di tenacia, ma in questo caso è stato anche più tenace del solito. *(Applausi).* Ha fatto bene, perché ha negoziato bene in nome e per conto del nostro Paese. Colleghi, qui siamo arrivati al punto: il richiamo che il Presidente del Consiglio ha fatto alle opposizioni - lo voglio dire con chiarezza - per me non è un richiamo formale. Per me non può essere un richiamo di comodo. So benissimo che le opposizioni la pensano diversamente sui temi europei e nessuno qui è Alice nel paese delle meraviglie: Forza Italia ha una posizione, un'altra ce l'ha Fratelli d'Italia e un'altra ancora Mi viene da dire che è un po' come per noi della maggioranza, perché anche noi sul MES la pensiamo in un modo gli uni e in un modo gli altri, ma qui non si tratta di evocare l'opposizione per dividerla,

sia una condivisione degli obiettivi tra maggioranza e opposizione. Questo rafforzerà il Governo, ma rafforzerà anche l'Italia, perché abbiamo bisogno di procedere insieme su scelte che diventano esistenziali per il nostro Paese. Paese. Per la prima volta si è mutualizzato il debito europeo, per la prima volta l'Italia ha la possibilità di avere, come Paese, l'attenzione che ha meritato anche per la gestione del Covid. Bisogna presentare piani credibili, non disperdersi in rivoli assistenziali, bisogna coinvolgere tutte le componenti della società civile, perché sappiamo che questo è il nostro grande obiettivo. Infine, un punto è stato omesso dal Presidente del Consiglio: il tema del MES. Colleghi, io farei un lodo sul MES; credo che ci siano partiti della maggioranza, come il MoVimento 5 Stelle, che si fidano del Presidente del Consiglio; molti altri ancora si fidano del Presidente del Consiglio e altri si fidano meno, come è naturale in politica. Il tema del MES vai deideologizzato e visto in concreto. Lo guardi lei, in concreto, con i suoi collaboratori, con i ministri Amendola, Gualtieri e Di Maio, con tutti coloro che sono in cabina di regia. Guardate voi le condizioni, le condizionalità, i tempi e vedete voi se il Paese avrà questa necessità. Evitiamo di continuare a dividerci, maggioranza e opposizione, sul tema del MES *(Applausi)* come se questo fosse un macigno ideologico che grava su questo Parlamento. Dobbiamo andare avanti con più serietà rispetto al passato e più serietà significa anche che affidiamo a lei la responsabilità di capire se le modalità del MES siano convenienti o no per il nostro Paese, magari per ristrutturare il sistema sanitario; poi chiaramente ci sarà il Parlamento. Credo che il Gruppo per le Autonomie, che ho l'onore di rappresentare, e per il quale parlerà poi anche la Capogruppo, sia pienamente convinto che l'esito sia stato positivo e che il Governo abbia eseguito bene il mandato ricevuto dal Parlamento. Le auguro buon lavoro perché il più deve ancora essere fatto.

ci siamo comportati da patrioti perché questo noi siamo. Lo dico con chiarezza, Presidente: noi abbiamo tifato per l'Italia, perché quando si va in Europa la nostra maglia è quella della nazionale. Devo dirle però con la stessa chiarezza che, a parti inverse, molto probabilmente - anzi, io ne avrei la certezza - avrebbero tifato per Rutte, Presidente, e lei di questo ne deve essere consapevole.

Noi crediamo che non siate stati capaci, che non siate capaci e che non sarete capaci, Presidente, a portare fuori l'Italia da questa crisi e tanti sono gli elementi che danno ragione al nostro pensiero.

il Governo e l'Italia sono usciti da questa trattativa con meno soldi a fondo perduto e più prestiti, quindi con un maggior debito, e non devo spiegarlo a lei. *(Commenti)*. È così, presidente Conte e sono contenta che la pensiamo diversamente. È uscita sicuramente con più debito e, come lei sa, noi abbiamo già un'enormità come debito pubblico e devo sottolineare che anche il suo Governo lo ha fatto crescere. Un altro elemento che però ci preoccupa moltissimo sono i tempi. I soldi arriveranno, sì, ma nel 2021, e forse nel secondo semestre del 2021. Quei soldi dovevano servire a salvare molte delle nostre aziende che il Covid-19 e questa crisi hanno messo in ginocchio. La nostra preoccupazione è che questi soldi arriveranno troppo tardi, quando le imprese avranno già chiuso, con un ulteriore problema che aumenterà moltissimo il tasso di disoccupazione. Conte, forse lei oggi non ci ha ascoltato, ma noi l'avevamo messa in guardia di quello che sarebbe potuto accadere in questo vertice europeo e le parlo delle condizionalità sul *recovery fund*. sono i soldi, è vero, e le abbiamo dato merito che lei, Presidente, si è battuto. Si poteva fare meglio, ma noi le riconosciamo di essersi sicuramente battuto per l'Italia. Adesso abbiamo però il problema di capire se quei soldi li potremo spendere; noi vediamo un rischio molto concreto che, forse, per spendere quei soldi dovremo passare troppo tempo a convincere gli olandesi ed i tedeschi e magari anche a farci dire cosa dovremo fare sulle nostre pensioni; o magari un domani capire che i clandestini ce li dobbiamo tenere tutti in Italia, nella nostra Nazione. Su questo non abbiamo nessuna chiarezza.

Abbiamo anche altre preoccupazioni, perché adesso ci sono festeggiamenti, applausi e dichiarazioni pazzesche ma noi abbiamo anche paura del cosiddetto freno di emergenza e non vorremmo che si realizzasse il sogno, coltivato da molti Paesi europei in questi anni, di perdere la nostra sovranità. Ci dovrebbe allora anche spiegare una cosa che non abbiamo capito: perché i famosi Paesi frugali, come l'Olanda (le cito un esempio per tutti), sono usciti da questi vertici con ancora più privilegi?

ossia uno sconto sui soldi che deve dare all'Europa, privilegio che - come lei sa molto bene - all'Italia non è mai stato concesso (chissà perché). Avremmo bisogno di qualche parola di chiarezza su questo punto. punto. Tanti sono i motivi di preoccupazione. Le chiederei allora, presidente Conte, di consigliare a Casalino e ai suoi uomini della comunicazione di essere più cauti e di evitare di parlare di questa montagna di miliardi, di questa pioggia di miliardi che sono arrivati,

queste categorie che sono state messe in ginocchio più di tante altre, stavano pagando le tasse. Ecco, credo che questo non si possa fare; per noi è assolutamente inaccettabile.

chiediamo che questi soldi vengano spesi per le infrastrutture, per le autostrade, per l'alta velocità, per il digitale, per la banda larga, per la scuola. Presidente Conte, sin quando lei non sarà in grado di far riaprire le scuole, l'Italia non potrà ripartire; se lo deve mettere ben chiaro in testa. Noi siamo patrioti, ma concludo dicendo che il nostro giudizio su questo Governo è pessimo, perché in tutto quello che avete fatto fino adesso non ne avete indovinata una. *(Applausi)*.

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio dei ministri, signor Ministro degli affari europei, onorevoli colleghi, l'Europa ha fatto bene, a differenza del 2012. L'Europa ha ottenuto un risultato straordinario, a differenza del 2012. E l'Italia, presidente Conte, è stata dalla parte giusta. Lei è stato bravo e noi gliene diamo atto, perché ha fatto l'interesse del Paese in un quadro di ideale europeo. Noi la apprezziamo per questo e le diciamo che, se questa sarà la strada su cui il Governo dovrà proseguire, saremo sempre più convintamente al fianco suo e di chi sceglie l'Europa contro il nazionalismo e il sovranismo. Glielo diciamo con un «bravo» che, dal nostro punto di vista, vale doppio: vale doppio perché, se potessimo tornare indietro all'improvviso, a un anno fa, vedremmo un Governo diverso. Quanto è cambiato da un Governo nella cui maggioranza stavano quelli che organizzavano le conferenze e le campagne elettorali con Alternative für Deutschland. Oggi il nostro riferimento in Germania è Angela Merkel, cui va la gratitudine alla quale faceva riferimento il senatore Casini. *(Applausi)*. In maggioranza stava chi evocava i gilet gialli in Italia:

ai miei colleghi - vorrei dire ai miei amici - del Partito Democratico. Forse, cari amici, adesso è chiaro perché, anche perché, anche contro le resistenze del nostro Gruppo dirigente di allora, un anno fa abbiamo scelto di prolungare la legislatura. Non era, come qualcuno ha detto, semplicemente il desiderio di allungare la vita di uno scranno parlamentare. Era qualcosa in più: l'idea che la politica potesse convertire il populismo era l'idea che un Governo sovranista potesse diventare europeista, e mi rivolgo a voi, perché la partita inizia adesso. Il bello o il brutto, il difficile inizia adesso. Saremo capaci di assumere la *leadership* per cui l'assistenzialismo diventa crescita, il giustizialismo diventa garantismo, la capacità di scommettere sul populismo diventa voglia di scommettere sulla politica? Questa è la sfida, signor Presidente, che ci vede su due campi di gioco diversi. Il senatore Salvini ha detto che questo accordo è una fregatura grossa come una casa

Oggi l'Europa batte un colpo, altro che fregatura. Però, questa scelta ci riempie di responsabilità. Il presidente Conte ha fatto l'elenco dei punti

perché adesso nessuno potrà evocare il nemico come causa del fallimento. Adesso la partita sta nelle nostre mani, nel bene e nel male, e adesso non è facile, perché la situazione esterna è complicata, perché la crisi morde severamente e perché, o facciamo scelte coraggiose, o saremo anche noi portati via dall'onda, che non è la seconda ondata del Coronavirus, ma è l'onda di ritorno delle aspettative che abbiamo creato. Signor Presidente, quando si vince una partita, c'è un sacco di gente che viene ad adularti: diciamo che io potrei parlare da cultore della materia per invitarla ad avere fiducia in chi la guarda negli occhi, come ha sempre fatto, in chi le dice qui in Parlamento - utilizzando il Parlamento come il luogo della discussione, non un luogo dove si mettono *like* - che su alcune cose siamo d'accordo e su altre abbiamo qualche resistenza. Glielo abbiamo detto sulle scuole e sui DPCM e lei, devo dargliene atto, ad esempio sul *family act* - approvato ieri dalla Camera in prima lettura - o sul piano infrastrutture - ci accingiamo a discutere il decreto semplificazioni - ha dato delle risposte. Ebbene, guardandola in faccia, le dico che non c'è mai stato negli ultimi trent'anni un Governo con queste risorse. Mettete il compasso sul 2020, utilizzate il raggio di apertura di trent'anni e arrivate al 1990: non c'è stato alcun Governo che abbia avuto queste risorse, evidentemente perché c'è una crisi che morde severamente. Penso - spero di sbagliarmi - che non ci sarà alcun Governo che nei prossimi trent'anni, girando il compasso da qui al 2050, avrà le stesse risorse. È un fatto epocale per la storia repubblicana. Di fronte a questo evidente elemento di novità, hanno ragione il Presidente del Consiglio dei ministri e il senatore Casini a chiedere un coinvolgimento delle opposizioni, che non sia formale, pur nelle differenze tra noi e loro, ma anche nelle differenze tra di loro (tra chi sta con la Merkel e chi con e chi con Wilders, tra chi sta con Rutte e chi con Le Pen). Noi abbiamo oggi uno spazio politico pazzesco e difficilissimo: è lo spazio della politica, non del populismo. Ecco perché, signor Presidente,

questo vuol dire fare della nuvola (non vivere con la testa tra le nuvole), del *cloud*, dei *big data* e dell'intelligenza artificiale la straordinaria occasione per valorizzare i talenti italiani

la moda. So che può sembrare una barzelletta, perché tutte le volte che si parla di moda in ambiti politici c'è sempre qualcuno che storce il naso. Voglio parlare di moda per dire che sta rischiando di saltare, per tessuto di ricchezza fatto di sarte, modellisti e piccoli artigiani (non sono semplicemente le modelle e i modelli). È un mondo in cui il *made in Italy* ha fatto la storia. Sono stato orgoglioso, quando era al Governo, di partecipare a una sfilata di moda (pur non avendone il *physique du rôle*) per dare una dimostrazione di vicinanza a quel mondo. È un mondo che sta "saltando in aria": si interviene attraverso la Cassa depositi e prestiti e strumenti *ad hoc* (un soggetto che magari riesce finalmente a creare il grande campione italiano nel settore della moda che piccole e grandi ambizioni personali ed egoismi non hanno permesso in passato), oppure un pezzo di economia salterà. Infine, vi è la sanità. Abbiamo il coraggio di dirlo? Nei prossimi dieci anni nella sanità cambierà tutto; mi riferisco alla medicina personalizzata e alle analisi che stanno cambiando profondamente il volto e le modalità della farmaceutica, dell'ospedalizzazione e della medicina di base. Per questo, signor Presidente, la invitiamo a riflettere attentamente sulla questione del MES. I 37 miliardi di euro del MES - sia chiaro a quest'Assemblea - hanno una condizionalità inferiore ai prestiti del *recovery fund*. Se non si ha il coraggio di dirlo, si sta mentendo. I 37 miliardi di euro del MES arrivano in autunno e io sfido l'intero arco parlamentare

che dica no al MES, perché si tratta di soldi che vanno ai cittadini. Presidente Conte, sorprenda il Parlamento e il Paese. Anziché una *task force*, ci regali ad agosto un dibattito parlamentare in cui la forza della maggioranza dovrà essere quella di sfidare le opposizioni non sulla base di un generico programma di riforme ma di un concreto *business plan* per il futuro del Paese. Andiamo in Aula ad agosto, sfidiamo le opposizioni e diciamo come vogliamo spendere questi soldi. Se lo faremo, signor Presidente, avremo dimostrato due cose: la prima è che la maggioranza c'è (lei l'ha citata) la seconda, ancora più importante, è che il Parlamento non abdica di fronte alle questioni del sondaggismo esasperato. Il Parlamento non è il luogo in cui si fanno le *standing ovation* o si mettono *like* su Facebook: il Parlamento è il luogo in cui si discute e la politica ha un senso. Nel mese di agosto 2019 abbiamo dimostrato che la politica aveva un senso; a noi il compito di dare un futuro al nostro Paese.

In questa mia opposizione costruttiva penso oggi di dover riconoscere, per onestà politica e intellettuale,

Penso che la vostra squadra abbia operato in modo costruttivo da mesi (ripeto, da mesi), il che nel merito dimostra anche che i pugni sul tavolo improvvisi non servono a molto.

sarebbe stato più forte se avesse già messo nero su bianco, anche per evitare critiche interessate e strumentali, progetti di riforma definiti e se la maggioranza non avesse mantenuto in piedi l'equivoco sul MES. Collega Casini, togliamo qualunque dato ideologico. E non è, signor Presidente, un problema di attenzione morbosa da parte mia; non è neanche una questione di pregiudizio: è una questione di giudizio netto e motivato sull'utilizzo e l'utilità di quei fondi, alle condizioni che voi stessi fortunatamente avete negoziato, giusto? Vi siete impegnati a togliere le condizionalità e ci siete riusciti. Alla fine di questo esito positivo, però, ancora non va bene. Io vorrei sfidare chiunque ad una assemblea di pazienti, familiari, medici, infermieri ed altri a dire: «Ne avevamo bisogno ma, sapete com'è, abbiamo fatto i signori chissà perché». Questo non si può fare, tant'è vero che abbiamo una fame di liquidità enorme, tant'è che state già pensando a un nuovo scostamento di bilancio. quindi su questo tema come cartina di tornasole non di ideologie ma di impostazioni economico-politiche e di necessità di questo Paese. C'è qualcuno che mi dice che non c'è bisogno di interventi nella sanità? Lo devo ancora vedere. O nelle scuole, di cui ancora non si sa neppure quando come e dove aprono?

2021, e avanti di questo passo. Anche le finalità sono diverse, perché il MES consente anche spese correnti sul tema sanitario e sull'istruzione, ad esempio, il *recovery fund* riguarda le riforme strutturali, giusto? Quindi abbiamo tempi diversi e scopi diversi di intervento. Io non so se questo sia un accordo storico appunto la storia), ma certamente è un accordo importante per consentire all'Europa di fare un passo in avanti. Ovviamente siamo lontani ancora da una costruzione federale, questo è evidente, ma adesso la palla torna a noi. Noi, da contributori netti, per necessità siamo oggi divenuti ricevitori netti. Questo, insomma, non è proprio brillante, ma facciamone almeno buon uso, in modo da riprendere a correre in qualche modo; e se non a correre, almeno a camminare. Io sono convinta che l'Europa abbia fatto il suo lavoro e il suo mestiere in tempi in cui non speravo neppure. Adesso tocca a noi, perché dopo la solidarietà europea è il momento della responsabilità italiana. E non dobbiamo avere paura se c'è una specie di controllo orizzontale di tutti su tutti. infatti dicendo che faremo le riforme, ma invece non le faremo? Credo invece che la correttezza e la lealtà siano parte integrante della credibilità di un Paese e del suo Governo.

straordinaria: la capacità di fare di una crisi drammatica un'opportunità per togliere questo Paese da tanti anni di blocco. anni di blocco. Lei deve dare a nome di tutti noi coraggio, fiducia e speranza a questo Paese in modo che tutti possiamo riprendere a camminare. Auguro davvero che, anche sul piano italiano, lei possa dimostrare la persistenza

*(PD)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, membri del Governo, autorevoli oggi è una giornata importante e io, magari con un po' di leggerezza, la vorrei definire una giornata di festa per il nostro Paese. È una bella giornata in cui sarebbe naturale, che tutti gli italiani si unissero intorno al proprio Governo, al proprio Presidente del Consiglio e al proprio Parlamento per viverla come si deve, come una grande vittoria. Gli italiani sono sempre stati descritti - forse, ci siamo anche sempre descritti - come quelli che si uniscono solo quando vincono i mondiali di calcio.

sulla capacità di tenuta del nostro Paese rispetto alle proposte che ci sarebbero state fatte e sulla capacità di gestire una trattativa complessa dal nostro Governo.

che l'Italia a testa alta in Europa, sapendo di aver fatto per decenni il proprio dovere, oggi era nelle condizioni di riscuotere, in un momento di difficoltà successiva all'emergenza sanitaria e in una fase di gravissima emergenza economica. E lo avete fatto fino in fondo, con il Parlamento al vostro fianco in tutti i passaggi, inclusi quelli recenti che ci sono stati anche in quest'Aula. Dopodiché, questo non può e non deve permetterci di allentare l'attenzione. Anzi, come è stato detto anche in interventi precedenti, l'attenzione vera inizia proprio oggi.

dall'Europa, si debba avere la forza, il coraggio, l'intenzione precisa di fare quelle riforme che ci sono state chieste; di farle semplicemente perché quelle riforme vanno nell'interesse del nostro Paese, della nostra comunità nazionale. fare quelle riforme e dare una spinta e un supporto ai nostri concittadini, alle nostre imprese, ai nostri lavoratori, ai nostri imprenditori, che oggi hanno bisogno più che mai che questa occasione non solo non sia persa ma sia sfruttata fino in fondo per garantire un futuro migliore alle nostre generazioni, signor Presidente. *(Applausi).* Come hanno detto in molti, confidiamo nel supporto costruttivo e anche dialettico, di confronto e qualche volta di scontro, da parte di tutte le forze politiche, che giustamente pretendono il coinvolgimento e il dialogo. Credo che il Parlamento sia il luogo dove questo confronto possa avvenire, ma partendo da una considerazione oggettiva del quadro nel quale ci troviamo. valutazione oggettiva non può che partire dal grande risultato ottenuto, dalla grande opportunità che abbiamo e dal dovere che abbiamo oggi nei confronti dei nostri cittadini di fare un piano di riforme, di farlo bene, e di ottemperare ai nostri doveri fino in fondo. Neanch'io mi esimo dal toccare il tema del MES. Signor Presidente del Consiglio, ho avuto più volte modo di dire cosa penso, e lo confermo oggi. Finalmente il quadro è chiaro, e invito lei e i suoi Ministri a valutare oggi le tante, grandi opportunità che ci sono state date dalla nostra Europa: Europa: dalla capacità della Banca centrale di comprare in maniera copiosa i nostri titoli fino ai provvedimenti previsti dal Sure in particolare sul lavoro, financo ovviamente al MES sugli interventi, sapendo che è un fondo disponibile in tempi più rapidi e con una chiara condizionalità. Chi dice che non ci sono condizionalità ma la chiara condizionalità è l'indirizzo di spesa, ovvero investimenti in ambito sanitario. Una sanità che ha tenuto in una fase d'emergenza ma che - lo sappiamo - ha davanti a sé la grande scommessa di un cambiamento per il futuro. Facciamola questa valutazione, senza pregiudizi e a favore di un fondo o dell'altro, senza schemi, anche da parte del Partito Democratico, signor Presidente del Consiglio e autorevoli Ministri. Verifichiamo semplicemente qual qual è l'interesse del nostro Paese e facciamo insieme le scelte che vanno esattamente in quella direzione. Facciamo tutti insieme il piano di riforme; aiutiamo noi oggi la nostra economia, i cittadini italiani, i nostri lavoratori, i nostri imprenditori e facciamo le scelte che la storia ci chiama a fare con urgenza. Facciamole in tempi rapidi. È il momento di agire, di saper prendere decisioni, di creare il consenso nel Parlamento e nel Paese. Non possiamo sottovalutare la fase. La festa di oggi per il miglior risultato ottenuto da parte di questo Governo non ci può far dimenticare i problemi che abbiamo quotidianamente nella nostra Italia: il fatto che il turismo sia in crisi, che il commercio si trovi in uno stato difficilissimo, che le imprese abbiano difficoltà a continuare l'attività, che la cassa integrazione verrà prorogata ma ma che i licenziamenti non possono essere bloccati per sempre (si può prorogare lo stop ai licenziamenti, ma non per sempre). Quindi, noi abbiamo il dovere di capire cosa fare, partendo, signor Presidente, dai fondi che il Governo negli anni non è riuscito a spendere in ogni Ministero; partendo dai fondi europei delle precedenti misure, che non sono ancora esauriti; partendo da tutte le opportunità. Ci sono le condizioni per tirare fuori il nostro Paese da questa situazione, per uscire più forti di prima, con maggiore autorevolezza, grazie a questo Governo, a questa maggioranza e a questo Parlamento tutto.

un buon lavoro nelle prossime settimane. Saranno settimane intense, dove dovranno esserci, insieme, capacità, senso di responsabilità e senso del dovere nei confronti degli italiani da parte di tutti. *(Applausi)*. PRESIDENTE.

Signor Presidente, signori membri del Governo, colleghe e colleghi, come Forza Italia, noi apprezziamo il risultato complessivo raggiunto con l'accordo dei 27 Paesi europei. È un risultato per l'Europa, è un risultato per l'Italia e lei, presidente Conte, ha fatto il suo dovere nella trattativa e nel rappresentare il nostro Paese. Rispetto all'intervento che mi ha preceduto, però, io penso che la festa dovranno farla gli italiani a fine operazione *recovery* e fondi strutturali, perché, in questo momento, mancano ancora tutte le azioni, che questo Governo non ha ancora fatto, nei confronti dell'economia e della società italiana, a partire da quelli che sono i principi dell'accordo dell'Unione europea. Parliamo di semplificazioni: il decreto attualmente in discussione semplifica molto poco. Apprezziamo, però, l'accordo per l'entità economica, che permette di raggiungere, tra

si avrà una mutualizzazione comunitaria, a livello europeo, dei 27 Paesi. È un grande fatto politico. Ci si è concentrati molto sulla parte ma questo è un grande fatto politico, che il nostro presidente, Silvio Berlusconi, ha voluto rimarcare nelle sue dichiarazioni. Tutto ciò permette all'Italia di godere di tassi sui finanziamenti molto convenienti di vantaggi per l'ingente quota di fondo perduto. Gli 81 miliardi del *recovery*, aggiunti naturalmente al quadro di finanza pluriennale, permettono di fare una valutazione molto seria sugli interventi, sugli interventi, che, in questo caso, devono essere le grandi infrastrutture: ferrovie, strade, scuole e intervento a fianco delle imprese che, in questo momento, soffrono ancora moltissimo, anche per È una sfida che, come Paese, dobbiamo saper cogliere e non sprecare. Il nostro essere favorevoli, certamente, non ci esime dal fare proprie ed essere attenti anche a tutte le critiche o riserve che vengono espresse sulle doppie condizionalità: condizioni di gestione sull'economia nazionale che, in linea con quanto anche nel programma del Partito popolare europeo, cui noi aderiamo, prevedono liberalizzazioni. Il Governo, in questo momento, va in senso esattamente opposto.

Finora tutti gli indirizzi del Governo non sono andati in queste direzioni, che sono direzioni normative e costituiscono anche il programma di Forza Italia.

Purtroppo è nota, prima di tutto a noi italiani, la nostra difficoltà ad attuare e a spendere in tempi certi e con investimenti efficaci i fondi strutturali: basta scorrere negli anni

ma anche dei programmi minori (Interreg e Leader non sono da meno), per renderci conto della nostra difficoltà nella capacità di spesa. Non deve più succedere. Stato e Regioni, i veri gestori, devono essere responsabili di quello che dovranno fare, dei programmi da mandare avanti. Permettete, colleghi,

ragionare nell'interesse dell'Italia e degli italiani. Colleghi, potremmo anche poi dividerci nelle scelte, che sono scelte politiche,

azione odierna a parte. È una grande occasione, ma il rischio è che la litigiosità che il vostro Governo finora ha manifestato la vanifichi e ci renda incapaci di coglierla. il centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia) ha anche posizioni diverse su alcuni settori e su alcuni particolari, ma ha posizioni univoche sull'obiettivo che deve avere il nostro Paese. comunque è all'opposizione, non si è ancora seduto a discutere per provare l'univocità su alcuni temi, che naturalmente non ci vedono sulla stessa posizione, il MES. Questa è la differenza: voi governate, quindi avete il dovere di trovare una posizione univoca, nell'interesse degli italiani. Forza Italia, come da indirizzo del presidente Berlusconi, ha sempre dato dimostrazione di responsabilità, ma chiediamo che il Governo ascolti le opposizioni (apprezzo che anche esponenti della maggioranza

Sappiate, noi saremo vigili e determinati affinché anche queste risorse non siano sprecate verso obiettivi elettoralistici o di propaganda. Noi non vogliamo questo tipo di obiettivi; noi ci impegneremo davvero per contribuire a cambiare l'Italia e a modernizzare il nostro Paese.

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, membri del Governo, innanzitutto, se c'è qualcosa di buono per l'Italia, siamo tutti contenti e su questo non ci piove. Valuteremo nei prossimi mesi se e quanto di buono ci sarà. Ho due obiezioni di metodo sul grande successo e sul giorno di festa. Questo è il primo caso in cui - rapportandolo alla vita reale del nostro Paese - un imprenditore (in questo caso, il Governo italiano o il Paese Italia) va in banca a chiedere un prestito, che dovrà restituire nell'arco di qualche anno, gli concedono, dopo quattro giorni di trattative, di insulti, di tira e molla, questo prestito, però gli dicono: «Amico mio, i soldi del prestito - che sono peraltro tuoi soldi, perché me li hai pagati tu negli anni - li spendi come ti dico io». Senza l'*okay* della Commissione europea, il prestito non viene erogato: chiamatelo freno di emergenza o voto a maggioranza. È un prestito un po' strano, signor Presidente del Consiglio: se da imprenditore andassi in banca a chiedere un prestito e mi dicessero che con quei soldi ci potrei... Tutti hanno parlato senza essere disturbati, colleghi, per cortesia. Abbiamo ascoltato in religioso silenzio il vostro trionfalismo: lasciate parlare anche l'opposizione, che è maggioranza nel Paese, o vi dà fastidio? *(Applausi).* Possiamo parlare a nome della maggioranza degli italiani o ci è vietato farlo?

se qualcuno - non in Aula, ma a casa - volesse approfondire, sono le parole del professor Alessandro Mangia, ordinario di diritto costituzionale della sovversiva università Cattolica di Milano, che sostanzialmente definisce questo prestito un super-MES. Veniamo però a quello che faremmo, se questi soldi arriveranno. Innanzi tutto, ricompenseremmo uno dei settori massacrati da questa trattativa (e mi spiace che il Ministro di competenza si sia allontanato): avete massacrato gli agricoltori, gli allevatori e i pescatori italiani. Ministro, ma non lo voglio distogliere dal dialogo con il senatore Faraone. Vengono tagliati 9 miliardi di euro alla Politica agricola comune, dei quali, stando alle associazioni degli agricoltori italiani, almeno 2 miliardi a un settore già in difficoltà:

il latte, l'olio, la carne, i salumi, la frutta, la verdura e il pesce italiani stanno soffrendo; e siccome l'uomo è ciò che mangia, se mangiamo male, veniamo su male. *In primis* quindi occorre difendere l'agricoltura e i prodotti italiani. Non è abbastanza nobile per i frequentatori di Capalbio parlare di agricoltura? C'è gente che si spacca la schiena per dar da mangiare ai nostri figli, quindi vi chiedo di portare rispetto a chi si alza alle 4 della mattina, che è stato dimenticato da questa trattativa. Questo è il luogo del confronto e del dibattito, per cui vorrei che ci fosse silenzio. *(Proteste).* Abbiamo ascoltato tutti e nessuno è stato interrotto: prego, senatore Salvini, Attenzione: faccio una precisazione, visto che ci sono cento parlamentari del PD e dei 5 Stelle che ritengono che per rilanciare l'agricoltura italiana occorra legalizzare e spacciare droga a nome e per conto dello Stato. *(Proteste).* Questo no: no: parlo di grano, frutta, verdura, olio, latte e formaggio, non di canne, per intenderci. Non ritengo la coltivazione e lo spaccio della canapa fondamentali per il futuro del nostro Paese, anzi ritengo che la droga sia morte da combattere paese per paese, città per città, scuola per scuola.

Non intendo che ci siano interruzioni di sorta. Ognuno dice quello che vuole. utilizzare una parte di questi millemila miliardi per sostenere l'agricoltura e la pesca italiane, utilizzare una parte di questi soldi per tagliare le tasse, ma lo faccia sul serio, signor Presidente del Consiglio. Se lei la settimana prossima porta in quest'Aula la proposta di taglio dell'IVA, i voti della Lega ci sono tutti, dal primo all'ultimo, ma porti una proposta di taglio delle tasse in quest'Aula, non sui giornali! *(Applausi)*. C'è depositata la proposta della Lega sulla *flat tax* per famiglie e imprese con redditi fino a 70.000 euro, al costo di 13 miliardi. Avete portato a casa 209 miliardi, 13 miliardi di questi 209 li usiamo per tagliare le tasse agli italiani o stiamo chiedendo troppo? A proposito, ricordo a qualche Sottosegretario che invitare i ristoratori che non ce la fanno a cambiare mestiere è un insulto alla gente che lavora.

Il 3 agosto verrà inaugurato il ponte di Genova e penso, a nome di tutta l'Assemblea del Senato, di ringraziare Genova, la Liguria, gli operai, i tecnici, gli architetti, gli ingegneri per il miracolo che hanno fatto. Ringrazio il sindaco di Genova e tutta la comunità di Genova per il miracolo che hanno fatto in quella città e vi chiedo di applicare il modello Genova a tutte le opere pubbliche ferme, come la Gronda di Genova.

dire che le code in autostrada i liguri se le inventano, di evitare di prendere in giro un'intera Regione e una popolazione che vorrebbe lavorare. *(Applausi. Commenti)*. Usiamo una parte di questi soldi per fare strade, autostrade, porti, aeroporti: la Gronda di Genova, la TAV, la dorsale adriatica, il ponte sullo Stretto di Messina, che sarebbe un bellissimo messaggio di cambiamento, di inventiva.

e lo chiedo da genitore - per la scuola italiana, non per prendere dei banchi con le rotelle che serviranno ai bambini durante la ricreazione, ma per digitalizzare, per sistemare aule magne, *(Applausi)*. Oggi leggiamo sul «Corriere della Sera» che il tempo pieno è a rischio per le scuole elementari: usate una parte di queste risorse per dare speranza e lavoro certo almeno a una parte dei 200.000 insegnanti precari che

in questo momento 373.000 pensionati italiani che hanno preso la residenza all'estero, ad esempio in Portogallo, dove per i primi dieci anni non si tassa la pensione di chi si trasferisce lì. proposta della Lega è di usare una parte di questi millemila miliardi per copiare il Portogallo e rendere esentasse la vita dei pensionati nelle Regioni del Sud del nostro Paese: la Calabria, la Puglia, la Sicilia, la Campania, la Sardegna, che sono anche più belle,

Se volete dire che Giuseppe Conte è migliore di Papa Francesco, ditelo voi, ma se noi abbiamo qualcosa da criticare, potremo farlo in quest'Aula, visto che la cassa integrazione ancora non l'avete pagata e i soldi in banca ancora non li avete dati? Possiamo farlo, sottovoce? Scuola, taglio delle tasse, taglio della burocrazia, giustizia, digitalizzazione dei tribunali, processo veloce e possibilmente separazione delle carriere per evitare nuovi casi Palamara. Separazione delle carriere: chi giudica, giudica; chi indaga, indaga. Sulle pensioni, vi prego di non tornare alla legge Fornero, non occorre uno scienziato per intuire che in base a questo accordo c'è la cancellazione di quota 100 e il ritorno alla legge Fornero. Quota 100 ha restituito vita, speranza e futuro a 300.000 donne e uomini in questo Paese, ha permesso a tanti giovani di cominciare a lavorare in questo Paese, se qualcuno pensa di cancellare quota 100 e tornare a quella gabbia che è la legge Fornero, la Lega farà le barricate dentro e fuori il Parlamento, perché alla legge Fornero, per quello che ci riguarda, non è possibile tornare, sarebbe un'ingiustizia sociale assolutamente

è al centro di questi fondi, per aumentare il numero delle borse di studio per i ragazzi e le ragazze laureati in medicina, che ad oggi devono andare all'estero per poter diventare medici.

perché per la prima volta nella storia è stata sequestrata e sigillata una caserma dei Carabinieri, a Piacenza, dove ci sono stati indagati ed arrestati. Da ex Ministro dell'interno, ribadisco che chi sbaglia, paga e chi sbaglia in divisa, paga come e più degli altri, ma questo non serva a nessuno per attaccare, disarmare o infangare le nostre Forze dell'ordine, le nostre donne e i nostri uomini in divisa. Le dico questo perché, per evitare morti e feriti sia fra le Forze dell'ordine, sia fra i catturandi, avevamo introdotto la sperimentazione del *taser*, la pistola a impulsi elettrici. Era tutto pronto, la sperimentazione era finita, poi, una circolare del Ministero dell'interno di queste ore non solo blocca l'ampliamento dell'utilizzo della pistola elettrica che funziona in tutto il mondo, ma chiede anche la restituzione dei dispositivi che erano stati dati in via sperimentale alle Forze dell'ordine. Non vorrei che dietro ci fosse un pregiudizio che vuole disarmare le nostre Forze dell'ordine, che invece vanno aiutate, incentivate e accompagnate. Mi sembra di aver dato più di uno spunto di utilizzo di questi soldi. Vi auguro buon lavoro, perché se fate un buon lavoro è una buona notizia per tutti gli italiani. L'unico problema, signor Presidente del Consiglio, è che è che gran parte di questi soldi arriveranno nei prossimi anni, ce lo avete detto voi. I primi prestiti, se tutto va bene, arriveranno a 2021 inoltrato. Le dico una cosa che chiunque giri l'Italia in questo momento tocca con mano: per molte imprese, per molte partite IVA, per molti artigiani, per molte famiglie e per molte mamme e papà, il problema economico è adesso, non è nel 2021. I soldi che arriveranno domani potrebbero non servire a niente perché rischiamo di perdere un milione di posti di lavoro nei prossimi mesi. In attesa dell'aiuto benefico di mamma Europa, l'Italia faccia tutto quello che stanno facendo gli altri Governi europei, aiutiamo le famiglie e le imprese adesso, perché domani potrebbe essere troppo tardi e rischiamo di non avere niente da festeggiare. In bocca al lupo a lei, ma soprattutto in bocca al lupo all'Italia, perché di promesse, in questi mesi, ne abbiamo sentite anche troppe. *(Applausi)*.

torniamo a noi dopo aver visto che il collega Salvini ha parlato di tutto tranne che dell'argomento per cui siamo qui in questo momento. Il percorso non può certo dirsi concluso, ma oggi quell'ideale di Europa che venne coltivato a Ventotene, in un periodo altrettanto difficile della storia, è più vicino. Questo grandissimo risultato, presidente Conte, è stato raggiunto grazie alle sue capacità e alla sponda, alla spinta, al sostegno che il MoVimento 5 Stelle le ha costantemente garantito. Il MoVimento 5 Stelle - voglio ribadire con nettezza - da anni conduce una battaglia che ha contribuito a rendere più fertile il terreno dal quale il cambiamento finalmente comincia a germogliare. L'accordo raggiunto in sede europea, dopo giorni di faticosissimo negoziato, introduce per la prima volta una condivisione del debito futuro per finanziare il *recovery fund*. Questa idea, nata a metà degli anni Novanta, da Jacques Delors, oggetto nei decenni di dibattiti infiniti e finora sempre naufragata contro gli egoismi di alcuni Paesi membri, oggi diventa realtà. Una realtà, certo, che dovrà ancora essere sviluppata, ma l'affermazione del principio e la sua prima applicazione rappresentano un passaggio fondamentale. L'Italia risulta beneficiaria della fetta più grande del *recovery fund*, 209 miliardi di euro, che sono il 28 per cento dei 750 miliardi, come ha ben precisato prima lei, complessivamente coinvolti nel piano. Non solo, all'interno di questa cifra, gli 82 miliardi di contributo a fondo perduto, che sono confermati per l'Italia, rappresentano la più alta dotazione rispetto agli altri *partner* europei. All'interno dei 209 miliardi è vero che la componente di prestiti è la più rilevante; una componente che, sappiamo bene, per un Paese che ha un debito pubblico che viaggia verso il 160 per cento del rapporto con il PIL non rappresenta certo lo strumento più maneggevole. però tutta l'impostazione del *recovery fund* che deve valutata. L'emissione di titoli da tripla A da parte della Commissione, cioè con il massimo del *rating*, è di per sé in grado di far scendere la temperatura sui nostri titoli e sul loro costo. In più i fondi *recovery* possono sostituire una quota di spese in conto capitale, cioè investimenti, che altrimenti sarebbero state finanziate con titoli di debito pubblico italiano ben più costosi. inoltre, che le risorse che derivano dal *recovery* dovranno essere restituite, ma a condizioni di favore e con una durata lunghissima. Presidente, abbiamo incassato un risultato davvero importante, viste le condizioni di partenza e soprattutto visto l'atteggiamento che hanno avuto alcuni Paesi frugali fino alla fine. A lei il merito di aver posto l'accento su una certa ipocrisia dei Paesi del Nord, in capo l'Olanda, che, da una parte, sbandierano la loro cultura calvinista di frugali formichine e, dall'altra, hanno dentro casa paradisi fiscali e normativi che ogni anno sottraggono ingenti risorse ai *partner* dell'Unione europea. Presidente, che il risultato raggiunto al vertice europeo ha cominciato a creare qualche incrinatura anche nelle reazioni delle opposizioni. Accanto a Fratelli d'Italia, che non ha potuto fare a meno di notare che lei è uscito in piedi dal negoziato, c'è la sempre più scomposta propaganda della Lega, che parla di fregatura grossa come una casa. Eppure un grande amico e alleato europeo della Lega, quel Geert Wilders che prima del vertice andava in giro con un cartello con sopra scritto «Non un centesimo all'Italia», ha commentato l'accordo dicendo che l'Unione europea ha fatto un regalo all'Italia, destinandole 82 miliardi a fondo perduto. La posizione dell'amico alleato olandese della Lega è tra le prove più evidenti del successo ottenuto dal Governo e della convulsa propaganda del principale partito di opposizione. nell'ultima settimana, con lo smantellamento del sistema affaristico cresciuto intorno ad Autostrade e con l'ottenimento del *recovery fund*, il Governo e il MoVimento 5 Stelle hanno ottenuto due risultati fondamentali per l'interesse di tutti gli italiani. Presidente, andiamo avanti senza curarci troppo dei rumori di sottofondo, andiamo avanti con l'accresciuta credibilità del Governo e dell'Italia, con il riconoscimento del ruolo di interlocutore fondamentale in tutte le principali decisioni europee. L'Unione europea, con l'accordo sul *recovery fund*, ci ha aperto una strada molto importante per effettuare investimenti in settori che rappresentano obiettivi storici del MoVimento 5 Stelle, come l'ambiente, il digitale e la transizione energetica. Sta a noi adesso mettere i soldi a terra in tempi rapidi. Ci stiamo lavorando con un ambizioso piano all'interno del decreto semplificazioni, che ha il merito di sveltire tutta una serie di procedure e di introdurre un innovativo sistema di monitoraggio delle opere pubbliche. Allo stesso tempo, signor Presidente, crediamo anche che l'Italia debba alimentare un suo canale autonomo di reperimento delle risorse, un piano di autofinanziamento che permetta al Paese di allentare una certa dipendenza dai mercati finanziari. Abbiamo un Paese da rimettere in carreggiata dopo la crisi economica globale più drammatica dal 1929. Questo è il momento della responsabilità, non delle chiacchiere, non della disinformazione né della propaganda; queste cose lasciamole fare ad altri.

UV))*. Signor Presidente, signor presidente Conte, per circa novanta ore i cittadini e i mercati hanno avuto gli occhi puntati sul Consiglio europeo nel quale era in gioco il futuro dell'Unione. Nonostante posizioni inizialmente molto distanti, si è trovato un compromesso che ha permesso a tutti gli attori di dirsi soddisfatti. Insomma, è un momento storico per l'Europa, ma anche per l'Italia, che adesso ha l'opportunità e i mezzi per sviluppare tutto il suo potenziale. Penso di non esagerare attestandole grande abilità nelle trattative, come le è stato riconosciuto anche dalla stampa estera e addirittura da parte dell'opposizione. Non vorrei paragonarla con Papa Francesco, ma direi che ha fatto un ottimo lavoro. Sono rimasti veramente in pochi a dire che un accordo che porta all'Italia 81 miliardi di euro a fondo perduto e 127 miliardi di prestito con un basso tasso di interesse sia una fregatura. Forse per i sovranisti si è rivelata una fregatura il fatto che i grandi nemici della loro narrazione, i Merkel e i Macron, si sono spesi per l'Italia. Tra l'altro, signor Presidente, i suoi colleghi,

che hanno detto che è stato fatto un grandissimo regalo all'Italia; Wilders ha contestualmente detto «a un popolo di evasori fiscali». Penso allora che i sovranisti si debbano chiarire le idee. Il *recovery fund* o è una grande fregatura oppure è un regalo per l'Italia e una fregatura per i Paesi frugali; tutti e due è un po' difficile.

In realtà è anche colpa del sovranismo se questa trattativa è stata così lunga e difficile. Non dimentichiamo che Kurz e Rutte, ma anche i Paesi scandinavi, hanno una forte opposizione antieuropea. In Olanda presto ci saranno le elezioni e quindi dovevano difendersi anche dalla propaganda di casa propria. è vero che in tutti questi anni l'Italia non ha certo brillato per l'utilizzo delle risorse europee, per attenzione ai conti pubblici o per riforme in grado di modernizzare il sistema e questo non dipende solo dai mezzi finanziari, perché semplificare non costa nulla. Pertanto, mi sembra logico e anche giusto che ci siano delle forme di supervisione sul modo con cui ciascun Paese spenderà queste risorse: ciò tutela tutti i cittadini europei, che hanno il diritto di avere il massimo beneficio dai soldi di questo debito comune, perché il punto più importante è che l'Europa, per la prima volta nella sua storia, ha accettato una mutualizzazione del debito. Presidente Conte, come dice l'adagio inglese citato oggi dal «Corriere della Sera»: «Stai attento a quello che desideri, perché potresti averlo». Effettivamente adesso viene la fase forse più difficile: riuscirà l'Italia a spendere al meglio le risorse e a fare le riforme che si attendono da almeno vent'anni? Da qui a ottobre abbiamo bisogno di un piano che dovrà essere dettagliato e contenere per ogni singolo intervento studi di fattibilità e dettaglio dei costi. Bisognerà coinvolgere le Regioni e le Province autonome, sia nello sviluppo che nella gestione dei progetti. Allo stesso tempo, non dobbiamo illuderci che il superfreno che voleva Mark Rutte sia uscito di scena. Siamo il Paese che riceverà più aiuti e prestiti e, dunque, da come li gestiremo dipenderà la credibilità dell'intera operazione.

Abbiamo davvero la possibilità storica di diventare un modello per il rilancio dopo questa drammatica crisi e mi auguro che tutto questo avvenga con il contributo delle opposizioni responsabili, perché questo non è il momento delle polemiche e delle divisioni: è il momento di scrivere una pagina nuova, quella di un'Italia più giusta e più moderna.

definito sciocca, perché ha una sola risposta: noi stiamo dalla parte dell'Italia, di chi rappresenta l'Italia nei consessi internazionali, di chi ha l'onere *pro tempore* di rappresentare il Paese che è anche e soprattutto il mio, il nostro Paese. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo anche in questa occasione, perché per noi la difesa dell'interesse nazionale non è un espediente retorico, ma è il primo e principale motivo per cui abbiamo fondato il nostro partito e gli abbiamo dato il nome che ha, Fratelli d'Italia. Credo che abbiamo dimostrato in tante occasioni, anche anche con capacità di prevenire le posizioni politiche che si sono succedute nel tempo, che la difesa dell'interesse nazionale non è stata una moda. Noi abbiamo difeso l'interesse nazionale anche quando dicevano che il MES era uno strumento che serviva alle banche tedesche e non certamente a quelle italiane. Abbiamo difeso gli interessi nazionali quando l'Italia è stata lasciata per anni da sola ad affrontare l'emergenza di clandestini che arrivavano dall'Africa del Nord, abbandonata a se stessa: l'Europa quella volta non c'era o faceva semplicemente finta Abbiamo difeso i nostri interessi nazionali anche attaccando, facendo nomi e cognomi, i Paesi cosiddetti o sedicenti frugali, i quali però coltivano al proprio interno paradisi fiscali che hanno ben poco di frugale, se posso permettermi.

il nostro atteggiamento è oggi esattamente quello di ieri e dell'altro ieri; è semplicemente un fattore di coerenza e noi, sulla coerenza, abbiamo costruito il consenso di questo partito. C'è poi un altro motivo, molto più pratico, per cui noi abbiamo fatto il tifo per l'Italia, ed è un motivo

possa augurarsi che l'Italia subisca un tracollo politico, sociale ed economico dal quale non potremmo uscire se non come Paese ridotto in macerie. Nessuno - anche chi sta all'opposizione e si candida a governare questo Paese in futuro

una pandemia paurosa, a cui non serve aggiungere la scorribanda di fondi speculativi che vengono a rubarci i nostri gioielli di famiglia, né la volontà di qualcuno

se quello che oggi voi raccontate è la salvezza dell'Italia o, semplicemente, un rinvio di problemi purtroppo ineludibili. Ad ogni modo noi - lo dico io e gliel'ha già detto il presidente Meloni - le riconosciamo oggi che il nostro Paese, che rischiava di essere travolto da quella trattativa, ne è uscito in piedi. Certo, poteva andare molto meglio ed è anche un po' strano leggere le dichiarazioni di *leader* nazionali e internazionali che dicono che tutti hanno vinto e nessuno ha perso. È difficile capire da che parte stia la verità. Sicuramente si tratta di un compromesso che non modifica di un centimetro il nostro giudizio sull'azione politica del suo Governo e dei suoi Ministri, il quale rimane estremamente negativo estremamente negativo per quello che lei ha fatto - o, meglio, non ha fatto - nei mesi di pandemia e crisi economica. È un giudizio negativo dovuto ai troppi annunci, ai pochi fatti, agli scarsi risultati e alle troppe passerelle che ci giustificano nell'atteggiamento molto prudente rispetto

è assai giustificato dal comportamento di alcuni suoi Ministri. Faccio una breve parentesi. Mancano quaranta giorni all'inizio dell'anno scolastico e il Paese ancora non sa se le scuole apriranno. Anche questo ha molto a che fare con la capacità del nostro Paese di mostrarsi integralmente e veramente europeo. Con la scuola allo sbando, è difficile poter chiedere in Europa un trattamento degno di un Paese civile. Forse qualche Ministro dovrebbe pensare se non sia il caso di cambiare presto mestiere. Oltre a questa parentesi, che era doverosa, voglio fare sue le parole con cui ha invitato anche le opposizioni a ragionamenti ragionamenti che fuoriescano dalla logica della contrapposizione, delle trincee e delle posizioni dovute, per cui chi è all'opposizione parla male del Governo e chi è al Governo parla male dell'opposizione. Con la stessa onestà intellettuale le chiedo se è vero - io credo che non lo sia - che quello che lei ha affrontato

che i peggiori nemici dell'Italia li abbiamo incontrati tra i membri del Partito Popolare e dell'area liberale, coloro che sono amici del vostro Governo nei consessi europei? E non è vero

gravato su un Paese libero come la Grecia per molti anni. È stata la nostra attività che ha spinto l'Europa a svegliarsi e a capire che non poteva andare avanti su questa strada. fatto rilevare che circa 200 miliardi, tra quelli assegnati complessivamente al *recovery fund*, avranno come destinazione il nostro Paese. Mi lasci però dire che tra il dire e il fare c'è di mezzo un mare, un mare di guai, di trappole, di incognite, di cose che non sappiamo e di cose che non abbiamo capito; e chissà chi ha capito veramente come andranno le cose. Sulla prima vicenda a cui vorrei fare cenno credo non abbia ancora parlato nessuno: mi riferisco alle nuove alle nuove tasse introdotte per finanziare il *recovery fund*. Signor Presidente, ho letto - lei mi smentisca se dico una cosa inesatta - che dal 1° gennaio 2021 verrà introdotta la *plastic tax*, una tassa sulla plastica che colpirà pesantemente i nostri produttori. Sono 11.000 i produttori italiani di plastica che garantiscono 30 miliardi di fatturato ogni anno. C'è stata la volontà di introdurre la *plastic tax*, ma non c'è stata la volontà di introdurre la sacrosanta tassa sul *web*, sul *web*, in assenza della quale i giganti del *web* possono fare concorrenza sleale nei confronti delle imprese italiane ed europee che non appartengono alla ristretta cerchia dei giganti del *web*. C'è poi la questione dei modi e dei tempi, che è essenziale,

motivo e condizione per cui l'Olanda, la Germania o il Paese di turno potrà di nuovo imporci o tentare di imporci una condizionalità pesante sul regime fiscale, sulle pensioni, sulla sanità o su quello che abbiamo visto negli ultimi anni. stata una spaventosa pandemia in questo Paese e nell'intero continente. Soltanto a fronte di centinaia di migliaia di morti, finalmente l'Unione europea ha capito che era il caso di mettere in campo uno strumento straordinario. I 1.500 miliardi previsti dalla Banca centrale europea si sono ridotti a poco più della metà. Vorrei che fosse chiaro che la posizione di Fratelli d'Italia non è andare a chiedere una cortesia, un favore, una scorciatoia

non accetta lezioni da chi non è in grado di fornirne, perché non ha le condizioni etiche per poterlo fare, anche se si autodefinisce puritano e frugale. L'Italia, però, non può nemmeno ancora una volta per essere un cattivo esempio. Io difendo il mio Paese, ma non lo posso difendere di fronte a una realtà che parla un linguaggio diverso e a cui corrisponde, purtroppo, una realtà diversa. Mi riferisco al fatto che gli ultimi scostamenti di bilancio che il vostro Governo ha preteso in sede europea sono serviti non per gli investimenti, ma per la spesa corrente, per la spesa elettorale, per la spesa utilizzata per comprare il consenso. Questo non può più capitare, perché credo, signor lei, se è onesto, lo deve ammettere - che anche in Europa abbiano visto i filmati dei suoi Ministri festeggiare dal balcone di Palazzo Chigi la cancellazione per decreto della povertà con il reddito cittadinanza, il reddito d'emergenza, l'assunzione di *navigator* pagati per non fare nulla.

nutrono disprezzo nei confronti dei commercialisti, delle professioni e delle imprese, o perché questo Governo ha necessità persino degli otto miliardi subito, *cash*, e non può rinunciare nemmeno a quelli? Se questa è la verità, vuol dire che abbiamo necessità ora di soldi, e non di soldi promessi ma che possiamo veramente utilizzare. E vuol dire che la condizione del nostro Paese non permette sogni di gloria, ma impone scelte non solo lungimiranti, ma anche assolutamente veloci. ho concluso anche se c'erano altre cose che avrei voluto dire. Il tempo è galantuomo e come sempre farà chiarezza delle promesse, dei trionfalismi e degli annunci. C'è però un altro problema più grave: l'Italia tempo da attendere non ne ha più.

dico con molta chiarezza che non stiamo facendo trionfalismi: stiamo riconoscendo il risultato del vertice europeo. E dobbiamo dirle con forza che è un risultato di portata storica, perché può dare, per la prima volta, la possibilità di cambiare non solo il nostro Paese, ma anche l'Europa.

quali sono state le conseguenze. Altri Paesi in Europa sanno quali sono state le conseguenze dell'idea rigorista

più legata al sogno, al progetto europeo, a un'idea politica dell'Europa ed è stata ridotta semplicemente ad accordi intergovernativi.

si può fare un passo in avanti; si può superare la logica intergovernativa e dell'unanimità. Si può superare e bloccare l'idea dei veti; si può costruire davvero una forza delle istituzioni europee.

per rilanciare con forza il progetto di integrazione europea. Lo scontro con i cosiddetti Paesi frugali - i giovanotti biondi, come li chiamo io

perseguito di voler bloccare un progetto di integrazione europea. Questo è stato anche l'elemento dello scontro in Europa, un elemento politico molto forte. Per questa ragione, il risultato è importante; per questo il risultato segna - a nostro avviso - una svolta significativa. E abbiamo svolto fino in fondo e bene il nostro ruolo

sovranisti, avremmo ottenuto 209 miliardi? Questa è la domanda che rivolgo a tutti. Bisogna essere onesti dal punto di vista intellettuale per riconoscerlo.

EU che cosa ci dice? Gli assi fondamentali sono il *green new deal,* l'innovazione digitale. È su questo che dobbiamo assolutamente correre. È questa la vera modernizzazione del Paese. Non pensiamo - e lei, presidente Conte, so

Colleghi, non si deve tornare alla normalità, perché la normalità è stato il problema, è stato uno dei problemi. Dobbiamo guardare avanti e avere una grande capacità.

Ha rimesso in campo una fiducia in un momento difficile e complicato e anche di questo noi la ringraziamo.

Voglio dirlo anche rispetto ad alcuni interventi che ho ascoltato prima. Il risultato ci consegna uno strumento molto ambizioso. Sappiamo quanti miliardi vengono mobilitati, sia per i prestiti che per i sussidi, ma voglio aggiungere solo una riflessione al riguardo. Per il nostro Paese c'è un elemento in più in questa intesa, che è importante sottolineare. Per la prima volta, l'Italia passerà dalla posizione di contributore netto a quella di beneficiario netto del bilancio dell'Unione europea. Riceveremo, cioè, più soldi di quanti ne versiamo. Presidente Conte, solo per questo, da storica sindacalista, le dico grazie. Il miglior accordo possibile è esattamente Il Partito Democratico, non da oggi, ma da sempre, ha creduto all'Europa. Lo abbiamo sempre fatto: spesso, purtroppo, da soli. Ci abbiamo creduto anche quando, come molte volte negli ultimi anni, abbiamo criticato scelte, rigidità, posizioni che ovviamente stavano in campo. Abbiamo criticato, ma non abbiamo mai smesso di essere europeisti, perché noi continuiamo a credere e a lavorare per il sogno di Altiero Spinelli e di Delors - come qualcuno ha ricordato cioè di un'Europa comunità, umana e politica, oltre che economica. Crediamo nell'Europa solidale, coesa, attenta ai diritti, al lavoro, all'educazione, cioè ai fattori mobilitanti

degli italiani e degli europei. Lo siamo perché il risultato ottenuto dal nostro Paese è veramente importante, grazie alla coerenza, alla qualità, alla determinazione e alla capacità di convergenza che si è determinata

Siamo soddisfatti, però, anche per il segnale che tutta l'Europa ha saputo dare, con una inversione di prospettiva che da anni speravamo di raggiungere. Io voglio fare questa osservazione, anche per il lavoro che il Ministro degli affari esteri fa e sta cercando di fare. Questo è un accordo che si definisce storico. Io lo sottolineo che è storico. E poi ce lo diremo diversamente. Ma, se non si colgono i cambiamenti in campo, vuol dire che noi continuiamo a pensare che è come il giorno precedente. No: il cambiamento è storico, perché l'Europa ha dimostrato finalmente di esserci e di nuovo - secondo me - finalmente c'è l'Europa. Ha dimostrato di avere come soggetto, l'Europa, politico-unitario la consapevolezza, la responsabilità di scegliere politicamente che, uniti, riusciamo a determinare le scelte conseguenti. Come ha detto qualcuno prima di me, questo accordo è la vittoria della politica, di una capacità anche di metodo della politica, ossia quella di confrontarsi con gli altri Paesi e con gli altri soggetti.

noi invece siamo stati in grado, su un terreno di convergenza di interessi comuni, di determinare una svolta storica. Guardate che questo è un elemento serio e dovremmo, da questo punto di vista, tutti consapevoli che la svolta è in questa scelta politica, perché è ciò che consegna la responsabilità. Ma consegna anche la ragione per la quale stiamo in un Parlamento, sia nazionale che europeo, e la ragione per la quale noi corrispondiamo ovviamente a chi ci ha eletto e alle fasi storiche Io penso che questo sia davvero un punto importante. Perché dico che è anche una vittoria del metodo della politica? Lo dico perché hanno vinto il dialogo, la ricerca di punti di unità, il superamento di ogni oltranzismo verso l'attitudine costruttiva. Quando si costruisce con i negoziati, ovviamente si cercano i punti di incontro: un metodo della politica. Signor Presidente, penso che sia giusto in questa Assemblea - e lo voglio fare anch'io, per la mia storia politica di sinistra

Merkel, è stata determinante. Vi è stata anche una coincidenza nel legame verso la Germania, che lei ha esercitato nei nostri confronti; certo, anche dei francesi, degli spagnoli e dei portoghesi, ma io penso che la sua scelta,

occasioni, quando preparavamo la delegazione al negoziato - che noi non possiamo sbagliare. C'è un punto di serietà, di responsabilità e di attenzione che tutti dobbiamo avere. Non sbagliare vuol dire anche saper leggere la realtà complessa dell'oggi non non con gli occhi di ieri. Noi dobbiamo sapere che questa opportunità di riforme e di innovazione è l'occasione storica che - come dice Paolo Gentiloni Silveri - capita due volte nella storia della vita di tanti, non capita spesso.

e materiali; infrastruttura immateriale vuol dire la filiera della conoscenza, che è il più grande intreccio fondamentale per una occupazione e un lavoro di qualità. questa visione, anche i passi, uno dietro l'altro, che facciamo sono vecchi. Lo voglio dire anche a chi usa le parole del *made in Italy*: tutto il *made in Italy*, tutta la filiera ha bisogno della trasversalità di innovazione, ha bisogno di superare il *gap* digitale.

il divario nell'occupazione delle donne e dei giovani. *(Applausi)*. Questo è un asse trasversale: se si parla di moda, se si parla di digitale, si deve dire quali sono i soggetti verso i quali noi facciamo un investimento vero; altrimenti sono solo chiacchiere e non riusciremo a superare i *gap* veri, i differenziali di genere, di generazione generazione e anche di territorio. Questo è un punto decisivo per la sostenibilità e l'attuazione dell'Agenda 2030 dell'ONU.

perché la scelta sarà autentica; diversamente, rischiamo di vedere ancora il futuro di questo Paese per settori, senza comprendere invece che i *gap* da superare sono orizzontali a tutta la nostra Nazione. Siccome però fatto un buon negoziato, se mi posso permettere, sono fiduciosa e la fiducia in politica è la precondizione per un Paese.

Signor Presidente, illustri membri del Governo, colleghi senatori, per essere chiari ed evitare equivoci, da cittadino italiano, rappresentante di questo Parlamento ed esponente di un movimento politico, sono soddisfatto, e molto, dell'esito del vertice di Bruxelles. Per essere altrettanto chiari, però, signor presidente Conte, lei ha varcato la soglia di quest'Aula accompagnato da squilli di trombe e rulli di tamburi, col sorriso di chi ha vinto una guerra: duplice errore, signor presidente Conte. Intanto, la guerra deve ancora cominciare la guerra deve ancora cominciare - lo sottolineo - e lei deve ancora essere misurato nella sostanza sulle sue capacità politiche. Se, dopo quattro giorni e quattro notti di trattativa, il vertice dei Capi di Stato e di Governo si è concluso con un accordo che ha scontentato in buona parte i Paesi cosiddetti frugali, è stato merito non della sua esperienza nel condurre trattative in Europa né della particolare autorevolezza del Governo che lei guida, guida, ma della cancelliera tedesca Angela Merkel. Ella - non per virtù, ma per condizione generale, è a fine mandato e a fine carriera - si è potuta permettere il lusso

e toni diversi, per decenni abbiamo auspicato. L'Europa si è sempre presentata divisa di fronte a tutte le grandi crisi globali (che fossero l'11 settembre, i migranti

per la prima volta, la politica e la sua logica entrano nella dinamica europea. Questa è un'occasione da cogliere. A chi rimpiange una presunta età dell'oro nel sovranismo nazionale, ricordo che durante la prima Repubblica la sovranità italiana era qualificata da un aggettivo non edificante, ossia "limitata": la nostra era una sovranità limitata. La verità, colleghi - lo sapete e lo sappiamo bene - è che l'Italia, per tutto il periodo della cosiddetta prima Repubblica, è stata tenuta in forma dal sistema internazionale, non per

sistema politico, istituzionale ed economico non abbia più trovato un punto di equilibrio. Questa è quindi la grande sfida che abbiamo di fronte: vincere il pregiudizio, che non è nuovo, purtroppo, nei confronti dell'Italia. Il simpatico *premier* olandese Rutte Rutte pensa oggi quel che ieri pensava la Merkel, che poi è quello che hanno sempre pensato i grandi viaggiatori che tra il '600 e l'800 attraversavano il Belpaese per fare il *grand tour* e annotavano sui loro diari giudizi non edificanti sulle nostre capacità

Qualcosa del genere evidentemente pensava anche chi, fino a poco tempo fa, teorizzava la secessione, senza fiducia quindi nell'unità nazionale né nella capacità di autogoverno di almeno metà della Nazione. Noi dobbiamo guadagnare quella fiducia. Io stento a credere che lei possa, da solo e con una maggioranza così fragile, riuscire in questo compito che è titanico. Signor Presidente del Consiglio, noi stiamo facendo debiti ed è ragionevole immaginare che, nell'arco di un paio d'anni, il debito italiano arrivi al 180 per cento; se non si riuscirà, se chi governerà non riuscirà a fare in modo che cresca di pari passo anche il PIL, sarà la rovina dell'Italia. La grande quantità di denaro che prima o poi arriverà - perché arriverà, lo sappiamo bene - potrà essere una grande risorsa o potrà essere la nostra rovina definitiva, perché i tassi di interesse si alzeranno, la forbice dello *spread* si divaricherà, gli investitori internazionali scapperanno e a quel punto non ci sarà più

che ha fatto e - a maggior ragione - che farà questo Governo e dalle sue mancate scelte del passato, del presente e del futuro dipenderà il futuro della Nazione per i prossimi decenni. Non possiamo permetterci errori. Quindi, il mio e il nostro appello è quello di cambiare immediatamente metodo. metodo. Lei ha di fronte a sé a breve scadenza tre sfide: il voto sullo scostamento di bilancio, il voto sul MES - signor presidente Conte, chiamiamolo Ugo, risolviamo il problema, cadono tutte le pregiudiziali ideologiche: si tratta di un'occasione da cogliere -

*(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ho sentito il signor Presidente del Consiglio parlare di una risposta tempestiva dell'Europa ai nostri problemi. Io ho visto che, dopo sei mesi dall'inizio dell'emergenza, ci si è riuniti e si è trovato un accordo politico dai contorni ancora indefiniti per procurarci, fra una decina di mesi, delle somme di cui probabilmente avremo anche bisogno. Non è questa la mia definizione di «tempestivo», ma del resto anche la mia definizione di «poderoso» è un po' diversa da quella del signor Presidente del Consiglio, che ha un lessico tutto suo, ma comunque senz'altro coerente. Ciò che preoccupa questa opposizione, che vuole essere responsabile, è che noi vorremmo essere convinti di essere di fronte a un passo storico e di vedere un film diverso da quello del 2012.

perché la cifra di 209 miliardi di cui si sente tanto parlare nei documenti disponibili, in particolare nelle conclusioni adottate dal Consiglio, non sono riuscito a rinvenire. Quello che si può rinvenire lo si vede nelle analisi che hanno fatto economisti familiari con questo argomento; per esempio, penso alla dottoressa Silvia Merler, senz'altro non una leghista. Con una serie di stime dichiarate tali dalla Commissione europea si può arrivare alla ragionevole ipotesi che l'Italia potrebbe avere appunto un'ottantina di miliardi di sussidi, ma occorre fare anche un'operazione di verità. Dovremmo forse ricordare che il bilancio dell'Unione europea è un bilancio a saldo zero e che quindi se 750 miliardi escono, 750 miliardi entrano, quindi non si può parlare dei 209 miliardi che asseritamente arriverebbero all'Italia, senza che questo risulti *per tabulas*, senza chiarire in quanti anni e quanto ci mette l'Italia, perché quando si va a fare questo calcolo e si valuta nel complesso, come direbbe il nostro signor Presidente del Consiglio, in una logica di pacchetto quello che è successo a Bruxelles, si vede che in realtà l'Italia resta un contribuente netto del progetto e che quindi può anche darsi che questi prestiti aiutino a risolvere un problema di liquidità, ma sono comunque prestiti che paghiamo; nessuno ci sta regalando niente. niente. Un certo tono trionfalistico verso un'Europa che non sarà più come prima risulta, quindi, a mio parere, smentito: in realtà l'Europa risulta più di prima intergovernativa e lo si è visto nella dinamica delle trattative; risulta sempre meno federale, perché sarebbe federale un'Europa che potesse decidere di andare in *deficit* e di non fare mera redistribuzione, sarebbe federale un'ipotesi come quella che oggi auspica Wolfgang Münchau, un tedesco che non vorrebbe essere tedesco e scrive sul «Financial Times», uno dei più autorevoli commentatori

la capacità impositiva e per legittimarne, con una base nei trattati, le emissioni di debito comune, che finora sono destinate a restare *una tantum* dai contorni sufficientemente indefiniti. Abbiamo quindi un prestito che non risolve i nostri problemi di liquidità, ma questa è anche abbastanza normale, perché il piano che l'Europa propone è intitolato all'Europa della prossima generazione. Quello che noi vorremmo capire è come arriviamo alla prossima generazione nel quadro di disfacimento del tessuto socio-economico del Paese che tanti colleghi

dato di 209, perché non è una banalità. Quando gli italiani si accorgeranno che in realtà non abbiamo scoperto lo scrigno degli zecchini d'oro, credo che ci sarà un rimbalzo. A me sembra in realtà che il film sia esattamente lo stesso: abbiamo una maggioranza che è oggi, per caso, quella stessa che aveva sostenuto come un passo storico il completamento dell'Unione bancaria e che esultava per questo decisivo passo dell'Europa. Anche l'opposizione è la stessa: noi dicevamo di stare attenti perché c'era il *bail in*, che era una cosa pericolosa. Chi aveva ragione lo ha detto la Storia e noi ancora ne siamo addolorati, perché non abbiamo dimenticato le vittime di quella catastrofe, e chi ha ragione oggi lo dirà la Storia. Grazie, signor Presidente.

Presidente, vedo che anche oggi nessuno dei suoi detrattori, se così possiamo definirli, aspri critici della sua azione in Europa, sono stati disposti a riconoscerle alcunché. Ma va bene, va bene l'applauso che ha ricevuto e che l'ha accolta nell'Aula da parte della maggioranza,

chi la applaude riconosce che nella sua azione di Governo e nel modo in cui ha portato il Paese nella considerazione europea c'è un lavoro coraggioso, determinato e tra l'altro nell'interesse del Paese, ma questa cosa non è stata compresa, perché ci si focalizza sugli uomini, sulle persone, in questo caso tra l'altro si tratta del rappresentante di una delle più alte istituzioni che viene a riferire, quindi è stato sbagliato anche

Io ho una risposta per entrambe le cose; allora, nel primo caso, con l'approvazione del *recovery fund* - tra l'altro, se usiamo piano di ripresa, si fa capire anche alle persone il significato e il senso profondo di questa parola che racchiude, all'esito di quella che è stata una tragedia collettiva, l'intenzione e la programmazione di venirne fuori dando delle risposte - abbiamo anzitutto l'emissione di debito comune. Ciò significa una cosa molto semplice; quando si fanno dei debiti, come qualcuno ha detto, in una visione unitaria, si fanno

parla sempre di Paese e di patria dovrebbe anteporre; il fatto che siamo credibili, che dietro di noi c'è un Governo che ha reagito a fronte di una certa inerzia europea, almeno all'indomani della crisi,

come ho detto prima, ci si può domandare perché allora c'è tanta rabbia se i risultati sono così scontati e così a beneficio del sistema Italia Paese. Italia Paese. Alle persone, che l'hanno attaccata fino adesso, brucia riconoscere il principio molto semplice di avere ottenuto un risultato, se non altro perché si sono spesi tanto in opposizione, strumentalizzazione e dico anche insulti - se possiamo dirlo - che adesso se la cavano dicendo che lei ha combattuto per l'Italia e che almeno questo glielo riconoscono.

a vedere, nel 2011 quelli che adesso la attaccano, sono quelli che all'interno del governo Berlusconi - così fuori ci capiscono - sostennero l'approvazione del MES

sul Governo. C'è un governo Tremonti, ci sono tasse su tasse, lo scudo fiscale e tutti i provvedimenti che conosciamo.

Qualcuno di importante disse che la storia si ripete o in tragedia, purtroppo, o in farsa. Io credo che l'opposizione si stia veramente ripetendo in questa farsa. *(Applausi)*. E la bella fregatura l'hanno data loro, continuando a dare sempre falsi segnali e false informazioni

questa mattina è mancato a Roma Bruno Modugno. Era nato a Roma nel 1933. Giornalista, scrittore, regista e autore: una vita e una carriera intense. Ha lavorato per «Il Giornale d'Italia», è stato capocronista di «Telesera», diretto da Ugo Zatterin. Nel 1964 ha iniziato la sua esperienza alla Rai per più di trent'anni è stato autore e conduttore di programmi culturali, che chi ha i capelli bianchi ricorda ancora, come «Racconti dal vero», «Pianeta», «Due per sette», «La parola e l'immagine», «L'alba dell'uomo» insieme a Folco Quilici, «Giorno di festa», «Arcobaleno», «L'estate è un'avventura». È stato autore e conduttore del settimanale di Rai2 «Mattina 2» e della trasmissione «Avventura», che ha rivoluzionato la TV dei ragazzi, e chi a quell'epoca era un ragazzo come me lo ricorda. Vedo che una collega annuisce, quindi vuol dire che Ha condotto il TG1 negli anni di piombo, gli anni più difficili di questo Paese. Ha girato numerosi documentari dedicati alla ricerca etnologica, all'avventura, all'ambiente e anche alla caccia. Ha diretto ventuno telefilm per la Rai e ha diretto il film «Re di macchia», tratto da un suo romanzo. Era un grande appassionato di montagna e anche un grande appassionato della caccia. caccia. A fine carriera, fino ad oggi, finché non si è spento, era direttore editoriale del canale 235 di Sky Caccia TV, da lui voluto. Era un grande amico, un grande uomo, per me un collega cacciatore che, proprio per la sua ultima attività televisiva, mancherà in questo Paese al popolo dei seguaci di Diana e a quei veri ambientalisti che, come lui diceva, sono i veri tutori dell'ambiente naturale giorni all'anno. Alla moglie le più sentite condoglianze. Ciao Bruno, grazie per tutto quello che con orgoglio e passione hai fatto sempre, come dicevi tu, alla faccia di chi ci vuole male, come tu ci hai insegnato. Ti salutiamo in tanti e che la terra ti sia lieve.

accogliamo le riformulazioni per quanto riguarda i punti richiesti dal Governo. Per i punti 9) e 10)

Signor Presidente, colleghi senatori, la tematica del lavoro giovanile in Italia è di particolare sensibilità. Secondo alcune fonti istituzionali che si riferiscono ai mesi precedenti il coronavirus, il nostro Paese detiene in Europa il non invidiabile primato

è vero che vi è stato un lieve miglioramento negli ultimi anni, ma il *gap* tra Italia e Unione europea è ancora molto alto e per colmare questo vuoto bisogna ricorrere a politiche concrete e mirate.

La crisi causata dall'epidemia da coronavirus ha creato infatti un enorme buco nell'economia italiana

il peggior risultato dalla fine della Seconda guerra mondiale. Solo qualche mese fa, prima della pandemia, le industrie manifatturiere del Nord avevano a trovare personale altamente specializzato o ben formato. Purtroppo, ora lo scenario è completamente cambiato. Uno scenario che si concretizzerà il prossimo autunno e che vedrà il nostro Paese coinvolto in una congiura macroeconomica potenzialmente disastrosa, con conseguenze anche in questo negative sull'occupazione giovanile e in genere. Basti pensare, colleghi, che i lavoratori più giovani non riescono a tornare a lavorare perché occupati prevalentemente in settori particolarmente colpiti dalla crisi economica e in parte ancora coinvolti dal blocco, come quello del turismo; cruciale la situazione nel settore alberghiero, della ristorazione e dell'intrattenimento. Che fare, allora, colleghi? Serve un cambio di rotta, culturale e antropologico, ancor prima che politico; serve una politica del lavoro mirata a favorire l'incontro tra domanda e offerta. Serve un approccio diverso; serve favorire il dialogo con le imprese, che non devono essere demonizzate, come qualcuno tende troppo spesso a fare. Serve abbandonare la politica assistenzialista, tanto cara a questo Esecutivo, per applicare una politica lavorativa che premi il merito e la voglia di fare. Abbiamo assistito nei mesi scorsi a scelte inopportune e prive di alcuna logica concreta; scelte frutto della demagogia e del consenso elettorale, nate senza alcun preventivo confronto con le associazioni di categoria imprenditoriali. Abbiamo - anzi, avete - pensato di risolvere il problema della disoccupazione giovanile negandolo. Avete pensato che, attuando la politica del reddito di cittadinanza, tutto si sarebbe risolto: una imperdonabile miopia culturale, ancor prima che politica; una miopia che di certo non stupisce se si pensa che questo Esecutivo vanta Ministri che nei mesi scorsi festeggiavano l'abolizione della povertà. La verità, cari colleghi, è ben altra: il Paese è sempre più povero, la disoccupazione aumenta e quella giovanile è destinata a farlo ancora di più. Abbandonate, colleghi della maggioranza, per il bene - anzi, per la sopravvivenza - del nostro Paese, alcuni sterili preconcetti che nel tempo avete voluto applicare. Basta con il reddito di cittadinanza, che peraltro i vostri alleati europei in queste ore (proprio ieri) non apprezzavano, o con i navigator. Basta con la demonizzazione del lavoro. Si apra una nuova fase - se ne siete capaci in cui ai giovani venga data una prospettiva futura concreta. Si adottino misure volte a consentire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese, mantenendo intatta la forza-lavoro, avendo particolare attenzione per quella giovanile, tra quelle maggiormente a rischio, prevedendo iniziative normative volte alla riduzione del carico fiscale sui datori di lavoro che abbiano scelto o scelgano di non ricorrere alla cassa integrazione. altresì che si possano prevedere prospettive di sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro privati, dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, che mantengano almeno l'80 per cento dei livelli occupazionali, specie dei giovani. Queste proposte concrete, colleghi, contenute nella nostra mozione che voteremo a breve, sono fondamentali per il rilancio del lavoro, specie di quello giovanile. Sono proposte che servono alle future generazioni, che non vogliono assistenza, ma la speranza, anzi, la certezza che ognuno possa essere artefice del proprio destino. Un Paese come il nostro non può negarlo. Per questo, signor Presidente, visto anche il parziale accoglimento, da parte del Governo, di tutte le mozioni presentate, anche della nostra, il nostro voto sarà favorevole.

diceva il grande artista. Umilmente, io la interpreto nel senso che la giovinezza, nell'idea dell'artista, è un punto di approdo. È energia, è voglia di fare, è futuro, è cambiamento e costruzione. io penso che le decisioni che sta prendendo la Commissione europea, la comunicazione della Commissione al Consiglio, che citavamo stamattina, il sostegno all'occupazione giovanile come un ponte verso il lavoro per la prossima generazione, assumano il senso di aiutare i giovani a plasmare la ripresa dell'Europa. Se solo pensiamo agli investimenti previsti dalla Commissione su digitale e transizione ecologica, ci rendiamo conto che dobbiamo ripartire dalle energie e dalle competenze delle ragazze e dei ragazzi. Il mondo digitale segna un passaggio d'epoca. Noi ora ci troviamo ad affrontare, in questo passaggio d'epoca, anche la crisi del post-coronavirus. Naturalmente, tutti noi ci auguriamo che possiamo definirla epoca post-coronavirus,

Stanno soffrendo i giovani che andavano a fare i lavori stagionali. Non occorre leggere le statistiche. Abbiamo figli, amici, parenti. Conosciamo le esperienze che ci raccontano. Siamo rappresentanti politici. politici. Stanno soffrendo i lavoratori stagionali e stanno soffrendo gli apprendisti, perché, come dicevamo stamattina, con la chiusura di molti centri di formazione, quella bellissima esperienza di inclusione, anche in zone del Paese più difficili, che era l'alternanza tra scuola e lavoro, viene un po' negata in questo periodo. Noi di questo ci dobbiamo occupare da subito. Si prevede, appunto, un calo di immatricolazione di 35.000 studenti e, su questo, si possono aggravare le disuguaglianze.

Sappiamo che in Italia la crisi del post-coronavirus si inserisce in un quadro già difficile, con una disoccupazione giovanile molto alta, con tanti giovani che non lavorano e non studiano, con tanti ragazzi sottopagati al primo impiego e con cervelli in fuga.

Questa può essere la crisi di un Paese: non possiamo guardare ai giovani come categoria debole. Al contrario, dobbiamo cambiare il nostro pensiero sui giovani. Dobbiamo informare il nostro pensiero su opportunità, su accesso, su costruzione di un mondo nuovo, su energia della forza del lavoro giovanile. Poiché il pensiero forma il linguaggio, anche il nostro linguaggio deve cambiare: deve essere improntato su crescita, lavoro, opportunità, futuro; un linguaggio di vita e di speranza. Non si può opporre alcuna negazione, a mio avviso, al termine «lavoro», perché un'accezione negativa non mette al centro il lavoro. Certo, ci possono essere delle fasi della vita in cui le persone cadono in povertà quindi hanno bisogno di sussidi, ma non è la questione che ci riguarda; quello che ci riguarda è mettere al centro sempre lo sviluppo e la crescita. Il lavoro, quindi, deve essere la prospettiva di vita dei giovani e noi abbiamo il dovere di fare in modo che sia così. Come diceva il grande Troisi, il lavoro non è mai una parola da sola, è sempre accompagnato da qualcosa: il lavoro che non si trova, il lavoro nero. di mettere al centro delle nostre politiche il lavoro. Certo, non tutti i giovani sono uguali, quindi dobbiamo fare politiche differenti tra chi sta a scuola e chi ha bisogno di alternare scuola e lavoro, tra i giovani che devono scegliere percorsi universitari, i giovani che si affacciano al lavoro per la prima volta, i giovani che non studiano e lavorano e quelli che che mettono su famiglia e devono avere anche la possibilità di trovare un lavoro (soprattutto le giovani donne), di continuare a lavorare e di fare scelte di genitorialità, in un Paese a così basso livello di natalità. Noi abbiamo il dovere di compiere scelte decisive. È questo il senso della mozione che abbiamo presentato come Italia Viva, sulla quale esprimiamo il nostro voto determinatamente favorevole. Annunciamo anche il nostro fermo impegno per i prossimi mesi sull'occupazione giovanile. Ci sono stati anche dei punti di incontro e di contatto con le mozioni dell'opposizione e credo che questo sia un valore importantissimo: non dividersi su alcune questioni.

del Parlamento e del Governo. Naturalmente c'è tempo per approvare disegni di legge e per discutere le proposte

proponiamo di discutere - come è scritto nella mozione, nella riformulazione del Governo - la possibilità di renderlo obbligatorio. Non lo abbiamo deciso (con la mozione non si decide), però sappiamo che ci sono tanti disegni di legge parlamentari e c'è un dibattito esterno molto forte su questo argomento; dobbiamo far tesoro

Credo sia necessario un grandissimo lavoro di consapevolezza. Come diceva Moro: «nel profondo, è una nuova umanità che vuole farsi, è il moto irresistibile della storia». Riprendendo e parafrasando di nuovo il grande pittore «ci vuole molto tempo per diventare giovani»,

il tema di cui discutiamo è molto importante ed è anche molto difficile

occupano del tema dell'occupazione giovanile). Cercherò poi di dire anche qualcosa sulle definizioni che spesso usiamo. Abbiamo anche la responsabilità di andare molto oltre in questa discussione, perché ciò di cui ci stiamo occupando oggi dovrebbe essere il cuore dell'iniziativa politica di questo Parlamento e del Governo che la mia maggioranza sta sostenendo. Lo dico perché nei nostri discorsi abbiamo imparato, in queste settimane, ad argomentare i nostri ragionamenti e le nostre riflessioni come se ci fossero un mondo prima della pandemia e uno da costruire dopo l'evento, se così possiamo chiamarlo, che ha investito il nostro Paese e il mondo intero. Probabilmente questa è una suddivisione giusta, però

che ha attraversato il mondo come ciò a cui dobbiamo approdare, una normalità da riconquistare o una dimensione che gelosamente dobbiamo custodire e ricostruire dopo averla persa. Dobbiamo essere molto chiari su questo punto: il mondo prima della pandemia conteneva

drammatico le coorti anagraficamente più giovani, ossia le nuove generazioni. Quella di cui stiamo discutendo è una generazione che già molto prima del Covid-19 ha conosciuto la dimensione della precarietà dell'incertezza sul proprio futuro e non dobbiamo considerare quella fase come un'arcadia a cui approdare, perché non è così.

quando si parla di occupazione giovanile, lo si debba fare a partire da tre considerazioni (ma naturalmente questo è il mio punto di vista). La prima è che dobbiamo liberarci definitivamente dall'ossessione di pensare che il lavoro, tanto più

che quando abbiamo messo mano alle regole del mercato del lavoro, senza in realtà avere semplicemente l'obiettivo di ammodernarlo, ma di renderlo più flessibile, alla fine lo abbiamo precarizzato. e in questa partita a pagare il prezzo più alto sono stati innanzitutto i più giovani, che hanno conosciuto, appena entrati appena entrati nel mondo del lavoro, una dimensione fatta di incertezza e precarietà. Liberiamoci di questa ossessione e mettiamoci in testa che il lavoro si crea attraverso grandi investimenti, grandi politiche industriali. Penso ad esempio a quella espressione di cui spesso forse un po' abusiamo e di cui dovremmo capire più il contenuto (o meglio più come declinarla) che tutti usiamo, cioè la transizione ecologica, la trasformazione in senso ambientale dell'organizzazione produttiva e del lavoro. Vorrei dire che probabilmente questa è la chiave, a patto che non sia semplicemente un vessillo elitista che riguarda soltanto qualche operazione in qualche area metropolitana. La transizione ecologica, tuttavia, può diventare elemento di creazione di nuova e buona occupazione e innanzitutto per i più giovani, se ha questo aspetto pervasivo, se diventa realmente democratica, cioè se investe ogni aspetto della nostra materiale. In questo senso liberiamoci quindi dall'idea - lo dico anche ai colleghi a proposito di qualche tentazione rispetto alle cose da fare nel prosieguo di questa legislatura - che il lavoro si possa creare semplicemente flessibilizzandolo, tanto più nella fase in cui stiamo entrando. In secondo

perché bisogna che ci convinciamo di un elemento: non c'è produttività, né capacità d'investimento e neanche di rilancio da parte del tessuto produttivo, senza che questo passi attraverso una scommessa sul capitale umano e sulle persone, quindi sulle lavoratrici e sui lavoratori, che devono però essere messi nella condizione di poter svolgere al meglio il proprio lavoro e di legarlo fino in fondo alle competenze, a ciò che le donne e gli uomini hanno studiato, hanno imparato; soprattutto però devono avere la tranquillità di svolgerlo sapendo che quel lavoro ha una dimensione di certezza, di sicurezza, anche in relazione alla possibilità che se si dovesse creare un vuoto, c'è un sistema di protezione che sorregge questi lavoratori.

quella crisi economica che noi ovviamente dobbiamo fare di tutto per contrastare, proprio di fronte a questo scenario dobbiamo cedere alla tentazione che il lavoro lo si deve creare purchessia e che quindi ci possa essere uno scambio tra la possibilità di ricominciare a crescere e i diritti dei lavoratori, delle persone. Non possiamo immaginare il futuro, quello più lontano ma anche quello più prossimo, quello che sta arrivando nei prossimi mesi e nei prossimi anni, con questa formula; formula; anzi, esorto i colleghi della maggioranza a riprendere il filo di un ragionamento che ha che fare con alcune discussioni, con alcune iniziative legislative che vanno riprese in mano. Penso al tema della parità salariale,

pena il pagare un prezzo enorme, non solo in termini materiali, ma di dignità. Infine, c'è una questione gigantesca, legata al tema dell'occupazione giovanile: scuola, formazione, università. Questo grande vuoto che si è determinato nella scuola è un vuoto che le nostre ragazze e i nostri ragazzi pagheranno e quindi il nostro compito, la nostra responsabilità è permettere che a settembre si a regime, in presenza, e stiamo lavorando su questo terreno. C'è però il grande tema dell'istruzione superiore, della formazione universitaria, ci sono giovani che in queste ore stanno decidendo di abbandonare l'università o di non iniziarla. Se assecondiamo questa dinamica, nell'Italia del dopo Covid, stiamo assecondando la crescita di disuguaglianze già esistenti, ci sono famiglie che stanno discutendo del fatto che non possono più permettersi di pagare le tasse universitarie ai propri figli. Quando parliamo di giovani, anziché riempirci la bocca mettiamo sul tavolo proposte che hanno a che fare con il diritto allo studio, con l'abbassamento se non con la neutralizzazione, per alcune fasce di giovani, delle tasse universitarie e mettiamo nelle condizioni questi giovani di evitare che la condizione delle che la condizione delle famiglie di provenienza possa determinare il loro futuro. Se questo fosse vero, determinerebbe anche il futuro di questo Paese. Dicevo prima della definizione di giovani: forse usiamo questo termine con un approccio un po' troppo Dovremmo riferirci ai giovani non come ad una categoria tra le altre, ma come se fosse una classe sociale, se mi consente in senso gramsciano, cioè una classe da emancipare, perché se emancipiamo i giovani, vorrei dire se li politicizziamo, se diventano consapevoli anche della propria condizione, avremo emancipato anche un Paese che, in quel caso, avrebbe più chiaro il proprio destino e il proprio futuro. Per questo voteremo la mozione

è il fatto che questa mozione porta all'attenzione del Parlamento un problema di cui si parla troppo poco e soprattutto per cui si fa troppo poco e lo fa con una serie di impegni precisi che abbracciano una strategia a tutto campo, che va dagli investimenti agli ammortizzatori sociali, dal sistema di istruzione e formazione al terzo settore. Il secondo motivo è che lo fa all'interno di una dimensione europea, di una visione di Europa non come bancomat senza condizioni, dove andare a prendere un po' di soldi, ma come spazio politico in cui si decide insieme come realizzare un'economia più verde, digitale, sostenibile, inclusiva, un'economia che sia un moltiplicatore di opportunità e di equità per le future generazioni. L'occupazione giovanile è al centro delle raccomandazioni europee verso l'Italia da anni. Queste sono le condizioni dell'Europa che non dobbiamo né temere, né ignorare, ma abbracciare. Parto dal problema: metà dei lavori distrutti durante la crisi da Covid-19 coinvolgevano persone sotto i trentacinque anni, nonostante questa fascia di età sia un quarto soltanto degli occupati. Si tratta di un divario enorme. In due mesi abbiamo perso 400.000 occupati, nonostante gran parte degli occupati fossero in cassa integrazione e ci fossero vincoli ai licenziamenti collettivi. Per ora le fasce più colpite sono quelle del lavoro autonomo, dei lavori temporanei, che non vedono rinnovato il proprio contratto e dei giovani in ingresso nel mercato del lavoro. intere coorti Covid che si vedono private di quelle prime opportunità e di quel trampolino di formazione all'interno del mercato del lavoro.

e, nel decennio dal 2008 al 2018, la quota di lavoro stabile era scesa del 10 per cento nella fascia di età sotto i trentaquattro anni, mentre cresceva in tutte le altre fasce di età. A fronte di questi problemi, la nostra spesa sociale impegna solo il 4 per cento per politiche che raggiungono persone o famiglie sotto i quaranta riguarda anche gli interventi che ancora oggi dobbiamo mettere in campo. Ancora oggi la politica fa fatica a mettere come priorità, soprattutto quando c'è da trovare soldi, l'occupazione e le speranze delle giovani generazioni. i giovani sono sempre al centro dei nostri convegni, ma raramente al centro delle nostre leggi di bilancio o dei nostri decreti di spesa dopo qualche scostamento. infatti ci preoccupiamo dei timori di chi un lavoro ce l'ha e ha paura di perderlo, ma altrettanto giustamente dovremmo preoccuparci dei sogni di chi un lavoro non ce l'ha e lo sta cercando, investendo le proprie competenze e la propria fatica in quella ricerca. Spesso nella nostra discussione pubblica abbiamo una visione stereotipata e discriminante di giovani e persone in cerca di lavoro; bamboccioni, i primi, pigri o scarsamente qualificati, i secondi. Questa visione è un alibi per non vedere la loro fatica, il loro impegno, le loro speranze e le loro competenze, la loro voglia di trovare nel lavoro uno strumento di emancipazione, non di ricevere assistenza fine a se stessa, la loro richiesta di fiducia sulla capacità di inseguire i propri sogni e di realizzare i propri progetti di vita. Queste categorie - giovani, donne, persone in cerca di lavoro - non sono le categorie fragili del mercato del lavoro, sono i giacimenti di petrolio sul quale ci troviamo perché la ripresa dell'occupazione e della nostra economia avverrà solo se riattiviamo le speranze e le capacità di giovani le capacità di giovani donne e disoccupati. Il secondo motivo è la dimensione europea nella quale giustamente si inserisce la mozione richiamando la strategia, dalla Commissione soltanto un mese fa, di sostegno all'occupazione giovanile come ponte verso il lavoro per la prossima generazione. Non ci sono però solo le raccomandazioni europee. Se guardiamo al fondo sociale *plus*, al fondo *react* EU*,* al fondo ripresa e resilienza, l'Europa investe quasi 700 miliardi sul *target* dell'occupazione giovanile e il rilancio della crescita per aumentare le opportunità di lavoro delle giovani generazioni. la nostra capacità di spendere per rilanciare la crescita e nuove risorse si misurerà giustamente anche sulla capacità di spendere le risorse già esistenti e che spesso spendiamo poco o male. Spendiamo poco o male perché il nostro sistema di politica attiva e di formazione ancora sconta una confusione di ruoli istituzionali tra Stato e Regioni e un sistema di *governance* e di investimenti che non riesce a liberare soluzioni. Proprio perché il problema deve essere al centro dell'agenda di Governo e dell'azione del Parlamento e lo deve essere all'interno di questa dimensione europea, io penso siano importanti gli impegni che la mozione consegna all'attività di Governo. Mi limito a citarne tre. Il primo è un piano di investimenti verso una transizione ecologica e tecnologica che però non si limiti a indicare queste assi di sviluppo, ma ponga come condizione precisa la priorità dell'occupazione e della formazione dei nostri giovani. Dovremo mettere al centro l'occupazione giovanile quando parliamo di strategie di crescita e di sviluppo e non solo quando parliamo di un'area di politiche settoriali. Aggiungerei che lo dobbiamo fare anche quando pensiamo a strumenti difensivi, quando diamo liquidità alle imprese per non chiudere, pensiamo sempre alle condizioni da imporre per mantenere gli occupati, ma anche quando c'è da fare uno sforzo di riqualificazione per aumentare

Il secondo impegno importante della mozione è sugli investimenti nel sistema duale, nell'istruzione professionale e negli ITS, al fine di rilanciare il nostro sistema dell'istruzione e della formazione. Il terzo impegno è su una riforma organica degli ammortizzatori sociali. sociali. Io inviterei il Parlamento e il Governo ad andare oltre l'impegno preciso contenuto nella mozione e a individuare strumenti di solidarietà espansiva e di staffetta generazionale. Abbiamo bisogno di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, che metta al centro i disoccupati, le persone in cerca di lavoro e i giovani in ingresso nel mercato Il reddito di cittadinanza è uno strumento utile per contrastare la povertà, non è una politica attiva che può risolvere il problema dei disoccupati. Se perdi un lavoro, non devi aspettare di perdere la casa per ricevere una garanzia certa del reddito da parte dello Stato, ma devi ricevere un salario di formazione, che ti dia la garanzia di un reddito forte mentre accetti, con un patto individuale, di riformarti, di rimetterti in gioco e di investire sulle tue competenze. Dobbiamo riformare la Naspi, togliendo il *decalage* e la riduzione del reddito, per dare una garanzia forte ai disoccupati, e dobbiamo renderla più generosa per i giovani. È inutile che nei nostri convegni continuiamo a dire ai giovani di mettersi in gioco e di passare da esperienze diverse (perché non esiste più il posto fisso), quando poi per avere un sussidio di disoccupazione pieno si devono avere quattro anni di contribuzione continuativa; dobbiamo dare dei requisiti ridotti ai giovani in ingresso nel mercato del lavoro. Serve un salario di formazione che pensi ai disoccupati e a chi perderà un lavoro nel nostro mercato del lavoro e non solo a chi un lavoro ce l'ha già. Su questo l'azione del Parlamento e del Governo dovrebbe essere forte, perché queste sono le terapie intensive del *welfare* e delle politiche del lavoro sulle quali dobbiamo investire per non farci trovare impreparati dalla crisi occupazionale, che rischia di diventare una crisi sociale nell'autunno. Salario di formazione, politiche attive del lavoro e politiche della formazione: se non lo facciamo oggi, domani potrebbe essere troppo tardi. Su questo c'è bisogno di visione e coraggio da parte della politica. Non risolveranno il problema le commissioni senza mandato della politica, perché non abbiamo bisogno di commissioni per sapere quali sono purtroppo i buchi del nostro sistema di *welfare* e quali sono le proposte per coprire quei buchi; quello che serve è coraggio e visione, per fare una riforma che metta in sicurezza il *welfare* di fronte alle crisi e alle sfide che abbiamo davanti. Gli impegni di questa mozione non bastano per questa riforma, ma mi auguro che siano almeno un segnale nella giusta direzione, perché ci sia attenzione da parte di tutti noi sul fatto che queste scelte e queste decisioni vanno fatte oggi; in autunno

Signor Presidente, signor membro del Governo, colleghe e colleghi,

d'ostacolo alla crescita del Paese nel momento attuale, ma soprattutto ci fa vedere un futuro pieno di preoccupazioni per il sistema Italia. Troppo importante è la figura dei giovani per poterla trascurare e non metterla al centro della nostra attenzione; così facendo veramente correremmo un rischio di *default* nel breve periodo, cioè nel periodo di transizione in cui le vecchie leve lasceranno il mondo del lavoro e dell'occupazione (da cui dipende anche la crescita del nostro sistema Italia) ai giovani. Questa è la grande preoccupazione. A questa preoccupazione aggiungiamo quella a cui assistiamo o abbiamo assistito in questa legislatura e forse anche alla fine della legislatura precedente, ovvero

le energie necessarie per riportare l'occupazione al centro della propria attenzione. Mi piace riprendere ciò che ho sentito poc'anzi dai relatori intervenuti sul reddito di cittadinanza, reddito di cittadinanza, reddito che non può essere prodromico ad un'occupazione. Il reddito di cittadinanza vale per quello che è e noi di Forza Italia siamo

secondo le volontà del Governo, strettamente collegato alla riforma delle politiche attive sul lavoro. reddito di cittadinanza e le politiche attive sul lavoro sicuramente non attuano la necessaria formazione

da un momento all'altro, così come le esigenze del mondo del lavoro. Quelle di venti anni fa non sono quelle di oggi e quelle dei prossimi vent'anni saranno addirittura inimmaginabile per i cambiamenti che ci saranno.

di formazione, ma anche occasioni di lavoro e ciò fa sì che il bene sia nemico del meglio; si colpisce il bene, che è il lavoro in attesa del meglio che non arriverà e non arriverà sicuramente in tempi brevi. Toglietevi dalla testa che voi con decreto-legge possiate creare posti di lavoro. Li potete creare quando inserite nelle politiche attive del lavoro il *navigator*;

particolarmente interessante dedicato al mondo del lavoro. Mi riferisco a quel termine inglese che così poco mi piace del *mismatching*, nel quale si dimostra quanto siano inattive le politiche del lavoro che state ponendo in essere o perlomeno quanto siano insufficienti: se è vero se è vero che 220.000 lavoratori sono oggi richiesti dal mondo del lavoro

e il mondo del lavoro vada da un'altra. Che ci sia cioè un *mismatching* non già tra le richieste e le offerte di lavoro ma tra la politica e il lavoro.

si preoccupano più per i figli - forse ancora più per i nipoti - che per se stessi: manca una vera politica destinata al lavoro.

Siamo certi che servono strumenti che non possono dare risultati immediati ma occorre un atteggiamento diverso verso questa forma di disoccupazione, che è il vero dramma

Signor Presidente, vorrei soffermarmi sulla situazione dei giovani in Italia. L'Italia è all'ultimo posto in Europa per occupati giovanili, ma è anche al primo posto per quanto riguarda i ragazzi scoraggiati, che non lavorano e che non studiano più. Meglio di noi sono la Bulgaria e la Romania. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, già un ragazzo su sei

con le riformulazioni e l'eliminazione di cinque capoversi delle premesse si andava un po' a svuotare il senso della nostra mozione, l'idea che abbiamo noi di futuro e l'idea che abbiamo noi delle politiche giovanili. La Lega con la sua mozione non ha vincolato il Governo in punti stringenti, ma ha chiesto semplicemente al Governo che venga attuato, per quanto riguarda le politiche attive del lavoro dei nostri ragazzi, strutturato e operativo di politiche serie. Io mi rendo conto che il ministro Spadafora ha una grossa responsabilità, perché la sua delega è molto importante. Tutti noi parliamo

Bisogna ridurre i dati della disoccupazione che ci vedono ultimi. Bisogna ridurre la dispersione scolastica con progetti importanti e con una certa lungimiranza. Bisogna azzerare la fuga dei cervelli all'estero. futuro» che ha portato avanti il ministro Spadafora sulle politiche giovanili, quella che lui chiama una maratona digitale su cui si baseranno tutte le politiche che porterà avanti il Ministro con la sua delega alle politiche giovanili. Si è dove i ragazzi si sono confrontati su quattro macrotemi: pianeta, partecipazione, percorsi e incontro. Da questo convegno è scaturito un documento fatto proprio da questi ragazzi che parla chiaro:

I giovani - lo dico al Governo e ai colleghi della maggioranza e dell'opposizione - sono una ricchezza da preservare e tutelare, ma soprattutto da valorizzare. dunque al Governo e al ministro Spadafora quale idea di futuro hanno per i nostri figli. Ieri in 11a Commissione è passato anche il Piano nazionale di riforma (PNR) per il 2020. Da quello che ho capito, da come sono state riformulate tutte le mozioni e da ciò che è stato eliminato dalle mozioni, le politiche del Governo per quanto riguarda i nostri ragazzi - lo dice anche il PNR - sono l'assistenzialismo

Mi fa specie che i colleghi dei 5 Stelle siano silenti su questa situazione, perché quando quando dei colleghi, ora alla maggioranza, erano all'opposizione tanto si sono battuti contro il reddito di cittadinanza e tante critiche sono arrivate per i centri per l'impiego. Eppure adesso, anche con la riformulazione della nostra mozione, si chiedeva di rafforzare le iniziative che sta portando avanti questo Governo. Ma questo Governo vuole incrementare il reddito di cittadinanza e vuole portare avanti un piano straordinario per per i centri per l'impiego con ancora assunzioni di *navigator*, quando la Corte dei conti ha dichiarato che il reddito di cittadinanza e tutto ciò che ne consegue è un *flop*. osservazione non arriva solo dalla Lega, che ora è all'opposizione; lo dice la Corte dei conti e critiche importanti sono arrivate anche dall'ANPAL. Noi abbiamo un'altra idea di futuro per i nostri ragazzi e, come ha detto anche il senatore Salvini stamattina, in ogni provvedimento utile il MoVimento 5 Stelle porta avanti l'idea di voler legalizzare la *cannabis*, che è una droga.

Le politiche attive sul lavoro, che tanto avete sbandierato, non sono ancora partite perché i centri per l'impiego nei Comuni non sono ancora partiti e stanno ancora cercando gli immobili. (*Commenti*).

C'è tutta questa agitazione sulle droghe. Il MoVimento 5 Stelle ha anche depositato a settembre 2019 un disegno di legge sulla legalizzazione della *cannabis*. La droga uccide e c'è l'esempio di quei ragazzini minorenni

che si è salvato e ha iniziato a quattordici anni con una canna. Tanti ragazzi sono morti partendo da una canna e quel libro ne è la testimonianza perché è scritto da chi si è salvato. Il MoVimento 5 Stelle per i nostri ragazzi vuole assistenzialismo e droga leggera libera. Noi abbiamo un'altra idea di futuro per i nostri ragazzi e non lo veniamo a dire oggi con la mozione; l'abbiamo detto in tutti i provvedimenti portando avanti degli emendamenti. Ci vogliono delle risorse adeguate, a partire dalla scuola. Ci vogliono tante iniziative, che non sono queste, e politiche attive vere del lavoro. Ci vuole un piano strutturato e organico per politiche serie. Noi per questo non abbiamo inserito dei punti stringenti per il Governo perché volevamo su questo piano strutturato e organico portare avanti anche le nostre idee. Sono belle le parole della senatrice Parente, del senatore Laforgia e del senatore Nannicini quando, riferendosi alla condivisione e alle politiche giovanili, dicono che devono

degli emendamenti sui contributi ai canoni d'affitto per gli studenti fuori sede, proponendo una dote didattica digitale per le famiglie che sono in difficoltà, l'esenzione per le famiglie in difficoltà dal pagamento delle rette scolastiche e il taglio delle tasse universitarie. Abbiamo presentato tanti emendamenti per far sì che i giovani potessero intraprendere un'attività e, soprattutto, per sostenere le *startup* innovative. Questi emendamenti sono stati tutti bocciati; bene, ve li rimettiamo sul tavolo. Discutiamone insieme,

si legge di assistenzialismo e di centri per l'impiego, che non hanno funzionato e non funzioneranno mai perché i numeri sono evidenti. Però, prendo in parola quanto detto dalla senatrice Parente, ovvero che dobbiamo essere uniti in questo obiettivo. Noi voteremo con senso di responsabilità a favore di tutte le mozioni presentate per le politiche giovanili, perché è una responsabilità che ci prendiamo. A noi stanno a cuore i giovani, ci siamo sempre battuti, fanno parte del nostro essere, fanno parte delle nostre battaglie, della nostra lungimiranza. Smettiamola, però, di dire che i giovani sono il futuro: i giovani sono il presente! *(Applausi)*. Dobbiamo lavorare nel presente per dare loro modo di avere un futuro; grossi spiragli non ce ne sono, ma noi andremo avanti a combattere per i nostri ragazzi.

oggi quest'Assemblea si trova ad affrontare un tema cruciale per il futuro dell'Italia: le prospettive legate all'inserimento nel mercato del lavoro delle nuove generazioni, in un momento straordinario per il nostro Paese, piegato sul piano economico e sociale da una crisi globale indotta dalla pandemia. La sfida che abbiamo davanti è di portata epocale; in gioco c'è il futuro, non solo di una generazione chiamata a sperimentare e vivere una fase spartiacque della storia dell'Italia, dell'Europa e dell'intero pianeta, ma soprattutto il futuro di una Nazione che per decenni, al netto di dichiarazioni di principio, non è stata capace di guardare oltre se stessa e che oggi paga lo scotto di non essere stata in grado di investire sul ricambio generazionale e sui giovani. Le politiche legate al mondo del lavoro non sono state in grado di offrire la possibilità a migliaia di giovani lavoratori di costruirsi un futuro, condannandoli - quasi fosse una costante - alla condizione di precariato a tempo indeterminato. Eppure, è sulle nuove generazioni e sulla loro stabilità sul piano occupazionale che si regge soprattutto l'intero sistema di protezione sociale di questo Paese, messo a dura prova oggi dalla discontinuità di contratti atipici che hanno impedito a intere generazioni di immaginare e disegnare il loro domani, dopo dopo anni di sacrifici e duro lavoro. A intere generazioni è stato negato il futuro, quello stesso futuro che, al contrario, i loro padri e le loro madri - e prima ancora i loro nonni - avevano avuto il diritto e la possibilità di progettare e costruire. L'era pre-covid ci ha consegnato un Paese dove la compagine giovanile per troppi anni è stata ignorata, denigrata e sfruttata. Come in un paradosso, viviamo in un Paese dove i nostri giovani, sebbene più istruiti dei loro padri e dei loro nonni, sono di fatto più poveri. L'Italia è il Paese con il tasso di disoccupazione giovanile più alto a livello comunitario, con altrettanto elevati numeri di giovani cosiddetti NEET (quelli non impegnati nello studio, nel lavoro o nella formazione) o di ragazze e ragazzi sottopagati al primo impiego. Senza considerare il fenomeno che, per anni, qualcuno ha definito dei cervelli in fuga: le nostri menti più promettenti, i giovani più istruiti che l'Italia non solo non ha saputo valorizzare e riconoscere ma che ha mortificato offrendo loro una sola via, quella della migrazione per ragioni economiche da un Paese capace di offrire loro un futuro precario, negando di fatto loro quel diritto costituzionalmente garantito a una retribuzione proporzionata e sufficiente alla qualità e quantità del lavoro svolto. Se guardiamo i numeri, è proprio l'Istat che ci rivela che l'Italia è un Paese dal quale sono partiti 117.000 italiani, di cui 30.000 laureati, per un totale di emigrati - negli anni tra il 2013 e il 2018 - di circa 200.000. L'Italia deve tornare ad essere un Paese per giovani. Oggi è tempo di interrogarsi, ragionare e riflettere su qual è il modello di società che vogliamo. Lavoro e giovani: due parole con un significato importantissimo, e che per la politica devono avere un significato importantissimo, non soltanto in questo periodo. Queste due parole devono rappresentare le parole chiave per tracciare le linee guida della nostra azione politica. La parola «lavoro» è presente in maniera ricorrente nella nostra Costituzione: agli articoli 1, 4, 35, 37 e così via. qual è la parola che gli si abbina spesso? «Lavoretto», come se potessero aspirare soltanto a quello. Invece, alla parola «giovani» dovremmo abbinare i termini «formazione», «investimento», «incentivazione», «valorizzazione». parole alle quali devono però corrispondere delle azioni concrete, che si realizzino in politiche di sviluppo che favoriscano non solo l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro attraverso incentivi all'assunzione ma che permettano loro di restarci e, soprattutto, di restare nel nostro Paese. Il percorso di inserimento

Questo comporta, ovviamente, l'osservazione dell'evoluzione del mercato del lavoro. Ben venga, allora, l'osservatorio che viene ripristinato con il decreto rilancio. L'investimento in formazione, però, deve continuare anche in costanza di rapporto di lavoro. Ecco allora che arriva il concetto di *long life learning*, il costante allenamento formativo che permette lavoratori di arricchirsi e di aggiornarsi anche durante la loro carriera. Ma come si realizza? A questa domanda rispondiamo che si fa attraverso l'istituzione di *campus* interni, di progetti di *formal mentoring*, che diano la possibilità alle nuove generazioni di interagire nel mondo del lavoro con la generazione più saggia, che ha molto da trasferire ai giovani attraverso questi percorsi e che per questo non deve sentirsi messa da parte. Questo passaggio di competenze è fondamentale affinché le nostre aziende continuino ad esistere e continuino a mantenere in alcuni settori quel *know-how* tipico del *made in Italy*, che nessuno ci può copiare. *(Applausi)*. La formazione, accompagnata da digitalizzazione e innovazione, è la vera parola chiave, che ci deve accompagnare nel percorso di uscita dal *tunnel* nel quale ci ha introdotto il Covid. Dobbiamo fare in modo che la parola «giovani» non si abbini più alla parola «precari». Molto è stato fatto con il decreto dignità, che ha portato ad un *boom* di contratti a tempo indeterminato, facendo scendere il tasso di disoccupazione che da anni non invertiva il proprio *trend*. Abbiamo finalmente previsto delle tutele ad una categoria di giovani come i *raider*: perché è vero che il lavoro si trasforma e bisogna adeguarsi, ma non per questo si deve rinunciare alle tutele, ai diritti e alla sicurezza sul lavoro. Ben venga, allora, l'intenzione anche del ministro Catalfo di istituire un tavolo con le parti sociali per la creazione di un CCNL per questa categoria. Facciamo in modo che il concetto di giovane lavoratrice non si abbini più al concetto di disparità retributiva e che le retribuzioni partono da un salario minimo che dia piena attuazione all'articolo 36 della nostra Costituzione. Soprattutto, facciamo in modo che il passaggio di testimone tra una generazione ed un'altra avvenga con sistemi strutturali, come ad esempio la staffetta generazionale, che può permettere ad una persona prossima alla pensione, nei tre anni precedenti, di affiancare un giovane assunto, ricevendo in cambio una riduzione dell'orario dell'orario di lavoro ma a contributi pieni. Facciamo in modo che le parole che proferiamo in queste aule o quelle che scriviamo nelle nostre mozioni non restino lettera morta. Lavoriamo insieme perché diventino strumenti legislativi efficaci. Solo mettendo da parte gli interessi di partito e lavorando per raggiungere gli obiettivi che ci prefisseremo prefisseremo potremo acquistare credibilità agli occhi dei giovani. Non parole, ma esempi. Questo è il regalo più grande che la politica può fare alle nuove generazioni.

Si cerca sempre di dare la colpa ai giovani di qualsiasi cosa, come per la *movida*. In questo caso, oggi si parlava dell'utilizzo della *cannabis*, che, per quanto ne possano dire i colleghi della Lega e tutti quelli che la pensano come loro, non è una droga: è semplicemente un'erba medica. Chi lo dice? Lo dicono le statistiche.

non è vero che dalla *cannabis* si passa alle droghe pesanti, perché non è proprio una droga; è un erba medica. D'altronde la vendiamo in farmacia dal 2007.

Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

L'Italia è un vero e proprio giacimento culturale, un concentrato straordinario di beni culturali e di siti riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità: tesori storici, culturali, artistici e museali, ma anche architettonici, oltre ad aree archeologiche e ad un immenso patrimonio archivistico e bibliotecario. Tutto questo ci rende famosi nel mondo e con linguaggi culturali diversi concorre al racconto della nostra civiltà millenaria. Cultura, arte, storia, monumenti, ma anche i paesaggi contribuiscono a questa ricchezza italiana sterminata e unica nel mondo, cui si accompagnano le culture locali, quelle delle cosiddette piccole patrie, e più in generale la cultura immateriale, caratterizzata dalle tradizioni, dai linguaggi locali, dal folklore, dalla ritualità delle festività, dagli spettacoli tipici e anche dalla cultura enogastronomica, altrettanto famosa a livello internazionale. Insomma, nell'immaginario globale credo di poter dire che siamo la Nazione dei saperi e dei sapori tradizionali ed antichi, eppure ancora vivi e vitali in ogni borgo italiano, anche il più piccolo, ricco e fortemente identitario. La mozione di Fratelli d'Italia nasce anche da queste premesse e dalla consapevolezza che abbiamo la responsabilità culturale, politica - e vorrei dire anche etica e morale non solo di salvaguardare l'intero patrimonio ma anche di tutelarlo per tramandarlo alle future generazioni. Abbiamo inoltre il dovere di trasmetterne il significato, che definirei metastorico, e il senso simbolico (che, come suggerisce anche l'etimologia di questo aggettivo, significa mettere insieme, unire, armonizzare idea e rappresentazione, significante e significato, e più semplicemente portare dentro e contenere). È questo il senso della memoria e della storia che i simboli trasmettono.

intorno ai quali ruota parte della nostra mozione. La tutela non è solo un dovere morale, ma anche un richiamo costituzionale: mi riferisco all'articolo 9, che pone in capo alla Repubblica il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e quello di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Aggiungo che lo Stato ha legislazione esclusiva nel settore della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali a norma dell'articolo 117 della Costituzione, mentre la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e l'organizzazione di attività culturali è oggetto di legislazione concorrente. Complessivamente, la tutela del patrimonio culturale e artistico nazionale chiama in causa sia le attività amministrative di regolamentazione che gli interventi operativi di conservazione e di difesa tesi a garantire la protezione e la salvaguardia dei beni e la loro pubblica fruizione. Esiste anche la tutela penale dei beni culturali dettata dalle norme contenute sia nel codice dei beni culturali e del paesaggio, che naturalmente nel codice penale. I reati di tutela del patrimonio culturale nazionale sono definiti tanto di natura delittuosa quanto contravvenzionale e mirano a impedire il depauperamento del patrimonio e a punire danneggiamenti, deturpamenti, imbrattamenti eccetera, di beni di interesse storico e artistico. Complessivamente - questo è un punto della mozione - emerge una disciplina non organica e disomogenea. Manca un corpo di norme tese esclusivamente a tutelare il patrimonio culturale secondo una visione che sia adeguata alla peculiarità e straordinarietà del patrimonio stesso. Insomma, il complesso delle norme vigenti, il sistema di tutela del patrimonio culturale si rivela insufficiente e gli strumenti a disposizione appaiono quasi inadeguati rispetto all'entità degli atti di vandalismo, distruzione volontaria, furto e danneggiamento. Ci appare dunque necessario tentare di modificare il quadro sanzionatorio penale rispetto a chi deturpa, vandalizza e distrugge beni riconosciuti universalmente di valore storico, artistico e culturale. Dopo il concetto di tutela, vorrei passare all'aspetto della valorizzazione, sul quale insiste la nostra mozione, che sottolinea come la valorizzazione dei beni culturali presupponga prima di tutto la loro tutela, che sta nel loro riconoscimento, nella loro conservazione e protezione e nel loro restauro. La stessa definizione di patrimonio culturale come contenuta nel succitato codice dei beni culturali e del paesaggio è complessa e riguarda beni artistici, storici, archeologici etnoantropologici, archivistici e bibliografici, ma anche paesaggistici, naturali, morfologici; potrei continuare ma in buona sostanza si tutto ciò che è testimonianza di civiltà e di bellezza. Il concetto e l'azione di valorizzazione direi che è in guerra permanente con ogni forma di abbandono, trascuratezza, degrado del patrimonio, nonché evidentemente con ogni atto di danneggiamento, distruzione, furto e vandalismo. sottolineare che la valorizzazione richiede anche impegno di risorse adeguate e paradossalmente proprio l'Italia, concentrato straordinario di beni culturali, è tra i Paesi europei che stanzia meno fondi destinati alla cultura, trascurando questa immensa risorsa che potrebbe trasformarsi in ricchezza, opportunità, risorsa strategica, volano di turismo per il rilancio nel nostro Paese. Proprio la situazione di post-pandemia, la crisi economica che stiamo attraversando con la crisi del settore del turismo, ci dimostra ancora una volta e ancora di più quanto il turismo sia volano e asse portante dell'economia,

il turismo che potrebbe rappresentare, perché lo ha sempre fatto e deve tornare a farlo, un circolo virtuoso per l'indotto lavorativo e la produzione di ricchezza. In questa In questa illustrazione non mi soffermo sulle criticità e le doglianze che circondano la questione dei beni culturali, che sono comunque puntualmente evidenziate nella nostra mozione e riguardano non solo le condizioni di incuria e di abbandono, insomma quelle che vengono definite propriamente le ferite alla bellezza, ma anche la questione eterna ed irrisolta dell'incompleto censimento delle opere d'arte del patrimonio nazionale, nonché quella delle risorse dedicate al personale impiegato nel nel settore. Con la nostra mozione si intende porre l'accento più che altro sul fatto che il patrimonio culturale rappresenta la storia, la memoria e l'identità di una Nazione e a sua volta costituisce il presupposto sia materiale che ideale per trasmettere la consapevolezza delle proprie radici e il complesso delle tradizioni di un popolo.

patrimonio) chiede al Governo sostanzialmente tre impegni fondamentali: la predisposizione di un piano straordinario di interventi finalizzati alla messa in sicurezza, tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio; l'adozione di iniziative anche di carattere normativo finalizzate a garantire una adeguata difesa del patrimonio culturale, anche con una riforma organica della disciplina sanzionatoria; infine, la predisposizione e l'adozione di strumenti tecnologici tecnologici avanzati per un'adeguata azione di sorveglianza e salvaguardia quindi del patrimonio culturale italiano. Nella dichiarazione di voto mi riserverò poi di aggiungere alcuni elementi, sperando in un'azione condivisa dell'Assemblea che porti a una votazione congiunta di tutte le mozioni presentate in materia.

Signor Presidente, innanzitutto è giusto ricordare che all'articolo 9 la nostra Costituzione chiede allo Stato di farsi garante della tutela del nostro patrimonio artistico e paesaggistico e recita testualmente: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». In questo modo, la Costituzione ci ricorda qual è anche la missione dello Stato, ovvero garantire una una adeguata custodia e quindi una adeguata fruizione da parte dei cittadini del ricco patrimonio artistico e, più in generale, culturale. La cultura, dunque, come un bene comune della comunità ed essenziale, perché alla conoscenza del nostro patrimonio e alla sua fruizione è legato sicuramente il diritto al benessere e alla conoscenza più in generale. più in generale. Su tutto il nostro territorio si adagia un ricco tessuto culturale, un patrimonio materiale e immateriale. Nel patrimonio materiale, come giustamente ha ricordato la senatrice Rauti, è bene ricordare che rientrano anche gli archivi e le biblioteche, che svolgono un ruolo importantissimo per per la conservazione, la diffusione e la trasmissione della nostra memoria storica e quindi anche la conoscenza della nostra storia, che è fondamentale per poi *intellegere* i fatti del presente. Nel patrimonio Nel patrimonio immateriale ricordiamo tutte le lingue locali, i saperi, la cultura orale, ma anche l'opera, la musica sinfonica, il balletto, la poesia, la letteratura, il cinema. Si tratta, quindi, di un ricco tessuto che si adagia su tutto il territorio nazionale. necessario uscire dalla logica, come abbiamo già ribadito tante volte in quest'Aula, dei grandi poli meta di turismo di massa e iniziare a ragionare sui distretti culturali diffusi, perché solo così facendo, solo sostenendo e implementando il nostro patrimonio diffuso su tutto il territorio, possiamo pensare di far svolgere appieno la sua funzione sociale alla nostra cultura. Ci vuole un impegno costante per la salvaguardia e per la custodia di questo patrimonio e abbiamo anche l'obbligo di promuoverne la conoscenza, la consapevolezza e la sensibilità fra le nuove generazioni, perché solo così così potremo garantire che esso sia trasmesso, conservato e valorizzato. Ci vuole quindi una piena assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti, sia pubblici che privati, ma prima di tutto ci dobbiamo ricordare, proprio in virtù dell'articolo 9 della nostra Costituzione, che è lo Stato

del fatto che noi siamo sempre più sottoposti alle ricadute dei cambiamenti climatici e il nostro patrimonio artistico è sempre più esposto a questi fenomeni avversi e dunque noi dobbiamo ragionare anche in questa ottica. La crisi sanitaria, che è stata anche una crisi sociale ed sociale ed economica, ha colpito duramente il comparto culturale e ha fatto emergere drammaticamente delle criticità che ancora affliggono questo comparto e, in particolare, i suoi lavoratori, imponendo quindi una riflessione sul *welfare* di questi lavoratori. Sono allora molto lieta che sia stato avviato questo tavolo interministeriale tra il Mibact e il Ministero del lavoro proprio per dedicarsi alla revisione e alla costruzione di una normativa dedicata ai lavoratori dello spettacolo dal vivo e del cinema in particolare, tenendo conto delle tipicità di questi lavoratori. lavoratori. Oltre a questo comparto, per il quale - ribadisco - siamo lieti si sia avviato questo tavolo interministeriale, dobbiamo pensare anche ai lavoratori di tutti gli altri settori che compongono il vasto comparto della cultura in Italia. Italia. Se, come qualche anno fa è stato detto, la cultura è un servizio essenziale, vorrei proprio partire dal primo degli impegni della mozione, ovvero stabilire i livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere stabiliti in piena armonia con il con il diritto all'accesso, quindi alla fruizione del nostro patrimonio, ma anche in piena armonia con la tutela dei lavoratori. Quando parlo di tutela dei lavoratori, chiaramente parlo non solo di una giusta retribuzione, ma anche di un giusto riconoscimento e inquadramento professionale e, per tornare al *welfare*, di un sistema previdenziale e assistenziale che tenga conto della particolare tipicità di questi lavoratori.

speciali, perché solo ampliando e completando questo piano per la fruizione, raggiungeremo l'obiettivo di avere una più vasta conoscenza del nostro patrimonio e di assolvere al nostro dovere costituzionale. Abbiamo altresì l'obbligo di prevedere un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria perché questo si ricollega direttamente alla fruizione, ma anche alla conservazione, alla tutela, alla valorizzazione e dunque alla promozione del nostro patrimonio e di tutto il circuito turistico che ad esso è collegato, laddove però noi dovremo sicuramente ragionare in termini di turismo sostenibile, ricordandoci della necessità di distretti culturali diffusi, anche nell'ottica di alleggerire i grandi poli di attrazione e dare

il mondo. Per fare questo dovremo trovare un'armonia tra professionismo e volontariato e rilanciare l'occupazione attraverso questi piani di manutenzione ordinaria e straordinaria e valorizzare le professioni che sono legate alla tutela e alla conservazione. Non dobbiamo dimenticarci dimenticarci neanche della ricerca, perché essa è un punto fondamentale nel mondo della tutela, della conservazione, ma anche della fruizione del nostro patrimonio e spesso, quando si parla di patrimonio artistico e culturale da tutelare e da valorizzare, si dimentica la grande importanza che la ricerca campo. Dovremo anche impegnarci in un progetto, che il Governo si è impegnato a portare avanti approvando un emendamento nella legge di bilancio 2020, sulla mappatura dei nostri beni statali abbandonati, di interesse storico e culturale, proprio nell'ottica di un rilancio occupazionale, di un recupero dei luoghi, quindi di un contrasto al consumo di suolo e quindi alla creazione anche di nuovi poli di aggregazione e di sviluppo sociale e non solo economico del territorio. Sono necessari progetti virtuosi di recupero dei centri storici, laddove mi pare che questa emergenza abbia reso evidente che c'è bisogno di ripensare alla ricostruzione di un tessuto sociale residenziale all'interno dei nostri centri storici, che altrimenti

Concludo con un cenno al patrimonio immateriale. Parlando di patrimonio immateriale e della sua vastità, ho parlato dell'opera lirica e della musica sinfonica. Dobbiamo assolutamente cogliere questa occasione - è un impegno che chiediamo al Governo per risolvere le criticità che affliggono questo settore da troppo tempo e che stanno emergendo drammaticamente non solo in questa emergenza sanitaria, sociale ed economica, ma anche per fatti di cronaca che stiamo leggendo sui quotidiani in questo ultimo periodo. Dobbiamo ripensare tutti insieme a come selezionare la *governance* di queste fondazioni, alla natura che devono avere, a come far sì che operino in maggiore trasparenza, a come tutelare i lavoratori. [**Presidenza del vice alla danza e al balletto. L'Italia è la culla della danza e del balletto e non possiamo dimenticarci questi lavoratori. Per fare tutto questo, dunque, dovremo impiegare parte degli aiuti che ci verranno dall'Europa per questo comparto perché, come ha ricordato più volte il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l'Italia può ripartire se riparte anche dalla sua enorme bellezza. *(Applausi)*.

ci sia un modo, più degli altri, per tenere insieme un Paese, per contrastare divisioni e diseguaglianze, per rilanciare la consapevolezza piena delle nostre potenzialità, una visione e un'idea di futuro, specialmente in un momento di smarrimento e di crisi sociale come quello che stiamo vivendo. Questo strumento è il fattore culturale e questo è il significato politico di questa nostra mozione. Dare vitalità al nostro patrimonio culturale rafforza un sentire collettivo, il senso dell'appartenenza a una storia in divenire, il senso dell'appartenenza a una comunità di destino, che per noi non è solo nazionale, ma è pienamente europea e internazionale. Mettere la cultura al centro di un nuovo modello di sviluppo significa stare dalla parte dei diritti, della società aperta, del pensiero critico; significa voler investire - ed è quello che vogliamo fare sul patrimonio culturale, sul paesaggio, sul turismo culturale come *asset* economico e di sviluppo strategico del nostro Paese, come leva di di inclusione e di integrazione civile e sociale. La cultura è un potente moltiplicatore economico, capace di creare lavoro e imprenditoria, di creare prodotto interno lordo, di creare ricchezza e di redistribuirla, ma è al tempo stesso uno straordinario moltiplicatore sociale, capace di creare condivisione di valori, convivenza, rispetto reciproco, legami di comunità, inclusione e dunque più sicurezza,

Costituzione repubblicana: questi termini sono tenuti insieme indissolubilmente, nell'articolo 9, per volere dei nostri padri costituenti; sono nel patto di cittadinanza che è alla base della nostra rinascita dopo le macerie morali e materiali del fascismo e della guerra. Aver tenuto insieme, nella stessa concezione di patrimonio, beni culturali e paesaggio anticipa con eccezionale modernità quanto dopo molti decenni è stato codificato dalla Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa, quella che noi abbiamo approvato qualche mese fa e che rivoluziona l'idea del patrimonio culturale, ampliandolo fino a racchiudere il il portato di tutto il vissuto storico-antropologico delle nostre comunità, frutto dell'interazione incessante nel corso del tempo tra le popolazioni e i luoghi. Del resto, la politica che è il coronamento dell'etica - diceva Aristotele - è proprio l'arte di costruire la città e per questo la funzione della politica è fare cittadinanza, è fare società, è affermare l'idea di bene comune; è affermare il pubblico interesse, la *publica utilitas*; affermare la preminenza del pubblico sull'interesse privato. Ed è per questo che, sin dall'età dei Comuni, dell'Umanesimo e poi del Rinascimento, l'idea di conservare e abbellire i nostri borghi storici, il nostro paesaggio, anche quello agrario, è tutt'uno con la promozione della nostra cultura, con la definizione del nostro carattere nazionale e la nostra identità. Per questo sappiamo che una speculazione edilizia o la chiusura di un teatro sfregiano la nostra identità. Sappiamo oggi più che mai, in questo tempo che viviamo, che questo è un punto di verità. Non è un'urgenza che nasce oggi, perché è a partire dal 2014 che il Mibact ha messo in atto molteplici piani di finanziamento, finalizzati alla messa in sicurezza, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, destinando fondi consistenti e crescenti. Sappiamo che la riforma delle soprintendenze, il rafforzamento e l'ammodernamento del sistema museale ha dato nuova linfa, ha portato nei nostri musei molte più persone di quanto sia mai accaduto, ha ridato legittimazione ad un patrimonio culturale che ha senso solo se viene fruito e vissuto senza steccati, rinsaldando un senso di appartenenza popolare e collettivo, rinnovando anche il rapporto tra le opere d'arte, il territorio e il loro contesto originario, che per nessuna ragione va spezzato, perché rappresenta la memoria storica e la funzione sociale del patrimonio culturale. Presidente, al centro di questa nostra mozione non c'è una visione statica di patrimonio culturale, ma un'idea dinamica per cui da esso nascono distretti culturali che portano alla valorizzazione di territori, in particolare le aree interne del nostro entroterra. recuperi il patrimonio edilizio per finalità artistiche, culturali, e tra esse le residenze degli artisti; che rivitalizzi i quartieri delle nostre città, la qualità urbanistica e ambientale; che leghi le risorse europee al sostegno, al recupero e alla fruizione del nostro patrimonio culturale diffuso. Soprattutto, colleghi, al centro di questa nostra mozione c'è il lavoro, ci sono le lavoratrici e i lavoratori dei beni culturali, perché c'è una carenza di organico insostenibile di oltre 5.000 unità, che pregiudica le enormi potenzialità del nostro sistema culturale. *(Applausi)*. Per questo chiediamo con forza al nostro Governo un piano di assunzioni subito, da qui al 2022. Per questo chiediamo misure straordinarie di reclutamento. Per questo chiediamo di proseguire nell'attuazione dei piani di finanziamento e di implementarne di nuovi. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale hanno bisogno di una nuova generazione di studiosi e di ricercatori, di una nuova generazione di professionisti dei beni culturali. Ne ha bisogno più che mai il nostro Paese, per riconquistare fiducia

Ha facoltà di parlare la senatrice Borgonzoni per illustrare la mozione n. 266.

e anche per cercare di mitigare quelle tensioni sociali che magari, in situazioni come quelle che stiamo vivendo ora, rischiano di essere amplificate. Non a caso, sono

impegnare il Governo ad aumentare le risorse finanziarie per un piano straordinario di interventi, che è fondamentale per la messa in sicurezza,

Potete anche votare a favore: non è un'offesa tanto grande, se troviamo dei punti di unione sulla cultura, potrebbe essere anche un bel segnale verso chi ci ascolta e ci vede. La cultura unisce: qui lo diciamo, dimostriamolo ogni tanto nei fatti.

volta di Bologna con i suoi portici; ci abbiamo lavorato tanto e per questo ringrazio gli uffici del Ministero. A tale proposito, ci vuole una gestione e uno sviluppo ecosostenibile di tutti i siti per cercare di promuovere anche i

una dote che comunque abbiamo, perché abbiamo l'ingegno e la creatività, ma forse abbiamo investito meno in tale ambito. Si deve investire molto di più, soprattutto perché i siti UNESCO possono essere quel traino per riportare tantissimo turismo straniero nel nostro Paese. Non a caso, una delle proposte che avevo fatto era proprio quella di promuovere

A loro va fatto veramente un applauso, però bisogna dare loro anche gli strumenti, oltre ad aumentare il personale che lavora

mettere in un sistema unico all'interno dell'alveo del codice penale tutte quelle fattispecie di reati - che ora sono nel codice dei beni culturali o in altre normative

sono imbrattati di continuo. Abbiamo visto quello che succede principalmente in altri Stati, non da noi, però sull'imbrattamento delle statue sicuramente bisogna dare un un messaggio chiaro, perché non si può imbrattare un monumento, non si può andare a giocare dentro una fontana, non si può distruggere una statua. Ritengo infatti che il passato sia fondamentale averlo davanti, molte volte anche per non ripeterlo.

Ho fatto l'apertura del simposio che c'è stato al Colosseo. Noi abbiamo i dati satellitari su buona parte del nostro territorio dal 2009 ad oggi;

che possa controllare e prevenire le cadute, che possa indicare gli interventi che vanno fatti. Avendo i dati dal 2009 ad oggi, abbiamo anche la fortuna di poter capire quali sono i movimenti strutturali normali di un palazzo o di un'area archeologica dovuti al riempimento e allo svuotamento d'acqua e secondo le stagioni dell'anno, quali sono gli interventi che invece vanno fatti immediatamente perché c'è il rischio di crollo. La prima sperimentazione era stata fatta a Pompei ed Ercolano già nel 2015-2016:

va formato e va assunto del nuovo personale e su questo possiamo essere i primi. Quando è stato fatto questo simposio, sono andata anche in Brasile, a Rio de Janeiro, a parlare di questa cosa: possiamo avere un modello da riportare agli altri perché, quando abbiamo fatto il simposio all'area archeologica del Colosseo, sono venuti da tutto il mondo. Possiamo essere primi anche in una nuova visione della tutela del patrimonio artistico. Cerchiamo di farlo e per farlo c'è bisogno di investire dei soldi. Visto che oggi siamo intervenuti e sembra che siamo tutti d'accordo

Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi, la mozione che ci troviamo a illustrare in questa serata, nella quale abbiamo ascoltato con grande attenzione gli interventi delle altre forze politiche, che ci trovano, in larga parte, sintonici rispetto ai principi fondanti che le animano, mi consente di evidenziare un aspetto molto importante dal quale

siamo al centro del Mediterraneo; siamo un giardino al centro del Mediterraneo e siamo, altresì, un museo a cielo aperto. Abbiamo dato i natali a personaggi straordinari della letteratura, dell'arte e delle arti figurative. Siamo stati un popolo che geneticamente è stato vocato a questo, ma non per caso. È una cultura, è una religione che si è fatta molto spesso cultura e una cultura che si è fatta prassi. Questa è la verità e la ragione per la quale abbiamo anche il compito di trasferire alle nuove il patrimonio che ci è stato consegnato in un momento anche particolarmente difficile. Assistiamo, infatti, a una furia iconoclasta che ha colpito gli Stati Uniti d'America, ma che purtroppo colpisce e infetta anche l'Italia. Abbiamo sentito e visto, per esempio, la distruzione a Bergamo qui c'è la nostra collega Gallone - del monumento ai caduti della Folgore: un atto assolutamente vergognoso. C'è chi dice che dovremmo togliere addirittura dai nostri libri di testo Dante Alighieri, nel passaggio in cui dice «mentre che tutto in lui veder m'attacco, guardommi e con le man s'aperse il petto, dicendo: Or vedi com'io mi dilacco! Vedi come storpiato è Maometto! Dinanzi a me sen va piangendo Alì, fesso nel volto dal mento al ciuffetto. E tutti li altri che tu vedi qui, seminator di scandalo e di scisma fuor vivi, e però son fessi così». Questo passaggio di Dante, che è stato mirabilmente rappresentato in un quadro di Giovanni da Modena nella cattedrale di Bologna,

quando venne in Italia il presidente della Repubblica islamica Rouhani, addirittura si arrivò a coprire le statue al museo del Campidoglio perché rappresentavano rappresentavano una nudità. Ma noi siamo una cultura che si è fatta straordinaria e siamo eredi della cultura greco-romana; non possiamo dimenticarlo. Allora cosa dovremmo fare?

ricordi di una Roma antica, della quale qualcuno forse si vorrebbe dimenticare, ma che noi non possiamo inevitabilmente dimenticare. Per preservare tutto questo

del nostro codice penale. Quelli non sono più articoli adatti al momento, adatti alla bisogna. Non dobbiamo prevedere la la procedibilità solamente a querela di alcuni reati - che qualcuno definisce bagatellari, piccoli, di poco interesse - ma abbiamo la necessità di indicare una procedibilità d'ufficio, affinché le procure della Repubblica si occupino anche di questo tipo di reati. reati. È vergognoso pensare e mettere al centro la politica giudiziaria del benaltrismo: abbiamo ben altro a cui pensare e quindi non si riflette sulla distruzione che sta avvenendo lentamente. Non bastano, infatti, i terremoti, non bastano le alluvioni né i fenomeni di logorazione del tempo; abbiamo anche, purtroppo, dei fessi in servizio permanente effettivo, che passano il loro tempo la notte a dipingere le case, i muri, i monumenti, a distruggere. non può più essere possibile. Quindi: procedibilità d'ufficio, innalzamento delle pene pecuniarie e, soprattutto, lavori socialmente utili per coloro che vengono catturati a commettere questo tipo di reato. *(Applausi)*. In che modo? Preparandoli, Preparandoli, facendo imparare loro un mestiere: olio di gomito a ripulire ciò che hanno deturpato; mano al portafogli per risarcire i danni provocati. Dobbiamo avere il coraggio di andare in quella direzione e di far sì che anche i nostri ragazzi, la nostra gioventù sappia che questo patrimonio è proprietà di tutti, indipendentemente dall'appartenenza politica. È un patrimonio di tutti e come tale va difeso e preservato. Noi in questa direzione vogliamo andare; vogliamo soprattutto che ci sia il coraggio anche da parte dell'Assemblea, in questa situazione, di porre mano a una riforma, che sarà importante, dei citati articoli 635 e 639, che ci consentirebbe di mettere tanti giovani nelle condizioni di imparare un mestiere, quello di ripulire i monumenti; di mettergli una bella pettorina tricolore - o scegliete voi il colore che volete - con scritto «Amo l'Italia», e metterli lì a lavorare nell'interesse della nostra Nazione. *(Applausi).* Questo è ciò che dobbiamo fare. Ci sono interessi straordinari, economici, che gravitano intorno alla difesa e alla preservazione dei monumenti. Proprio noi, che siamo il primo Paese al mondo come detenzione di patrimonio artistico - secondo qualcuno, fino al 75 per cento - dovremmo essere veramente orgogliosi di questo. E a coloro che si permettono dissentire, di essere in sintonia con una certa "creatività" che distrugge, dobbiamo dire che il momento è finito: dobbiamo dire loro che dobbiamo amare veramente la nostra Patria Italia; dobbiamo amare questo Paese e incominciare a farlo dalle piccole cose. Quindi, non si deturpano più muri e monumenti, ma si devono riconvertire. Coloro che fanno questi corsi, quindi imparano un mestiere,

una ragione tipicamente italiana, quella del contrappasso. Ebbene, mandiamoli a ripulire i monumenti perché è la cosa, secondo me, più importante che potremmo davvero fare, anche per la gioia dei

particolare e un'elevazione d'animo, che è estremamente importante in un momento di decadenza anche culturale e politica. Riprendiamoci gli spazi che ci meritiamo. Portiamo la politica a quell'altezza che essa stessa

nostra mozione, abbia visto la presentazione di altre quattro mozioni, tutte animate dalla medesima volontà di valorizzazione e tutela del patrimonio artistico nazionale. È stato bello il dibattito che abbiamo ascoltato in Aula, perché sono stati molti gli spunti, che ho apprezzato, anche delle mozioni altrui. Mi ha colpito molto l'intervento del collega Aimi, con il quale condivido la preoccupazione per i recenti attentati operati ad opere simbolo di storia e cultura, episodi che la cronaca ci ha restituito; una sorta di furore neoiconoclasta, che viene ricondotto da taluni analisti alla cosiddetta categoria della *cancel culture*, ovvero la cultura della cancellazione, dettata dalla volontà di rimuovere la storia e la memoria, attaccando statue, monumenti simbolici e i valori che rappresentano. Ci preoccupa il fenomeno di cancellazione e di rimozione del passato, che ha nei *social* - come è noto - il suo megafono e che, dal nostro punto di vista, rappresenta una deriva pericolosa anticulturale. Anche noi, collega Aimi, abbiamo presentato un disegno di legge, che, senza entrare nell'articolato, concettualmente punta a inasprire confronti di chi compie atti vandalici, deturpa e distrugge beni storici e artistici. È anche in virtù del disegno di legge che abbiamo presentato che mi sento - come ho già dichiarato - di accettare quanto è stato proposto dal Governo rispetto alla nostra mozione, ovvero espungere due parti e riformularne alcune.

anche per quello che ho ascoltato, che vi sia un filo rosso che le attraversa e le accomuna tutte; sia pure con diversi accenti e sfumature, tutte nascono dall'esigenza condivisa di difesa del patrimonio nazionale, della storia che esso rappresenta e della memoria che ci tramanda. È quindi qualcosa di collettivo, di condiviso, di comunitario, di comune senso di appartenenza e di orgoglio. Aggiungo che in tutte le mozioni c'è - a mio avviso - il desiderio - forse, lasciatemelo dire, anche accentuato dalla crisi che stiamo attraversando - di restituzione di restituzione di senso e di valore a tutto ciò che ci circonda, a tutto ciò che abbiamo ricevuto e che troppo spesso non abbiamo saputo rispettare abbastanza, dall'ambiente al patrimonio artistico. È allora forse il momento di rovesciare

perché è bello constatare che su alcuni temi si riescano a trovare convergenze e trasversalità nell'Assemblea. Penso che, su un tema così caratterizzante l'identità italiana, come il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale del nostro Paese, sia bello vedere che nelle diverse mozioni ci sono punti che ritornano e questioni che si riaffacciano. C'è quindi una volontà politica trasversale di potenziare questo ambito, questo settore, per

ma anche estremamente ricco di borghi, di quella che viene definita l'Italia minore, che sa offrire comunque grandi opportunità ai turisti oltre che, ovviamente, ai residenti; un'Italia minore

e della musica sinfonica: un grandissimo patrimonio del nostro Paese che, proprio nell'attuale fase così difficile, rischia di uscire pesantemente colpito

è rimasto arenato e meriterebbe di essere ripreso e, proprio per le condizioni che stiamo vivendo, rilanciato. C'è poi il tema dell'educazione. Abbiamo bisogno di educare i nostri giovani, a partire dalle scuole, allo straordinario valore del nostro patrimonio storico-artistico, che - come dicevo all'inizio di quest'intervento - contribuisce costruire l'identità del nostro Paese. Infine, le risorse: ovviamente tutte queste cose importanti e interessanti non si possono porre in essere se non abbiamo a disposizione nuove e anche rilevanti risorse. Spiace registrare come nel nostro Paese le amministrazioni regionali e comunali fatichino a operare in modo da fruire pienamente delle risorse che l'Europa già ci mette a disposizione. I fondi europei destinati alla cultura spesso restano inattivi per l'incapacità di attingervi attraverso

specifici dedicati proprio all'attingimento delle risorse che i bandi europei mettono a disposizione. In questo modo potremmo aiutare le amministrazioni locali a spingere spingere su progetti dedicati alla cultura e al patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale del nostro Paese. Italia Viva voterà a favore delle mozioni che ha sottoscritto e ovviamente di quelle che hanno ricevuto il parere favorevole del Governo.

è centrale sulla questione che ci troviamo ad affrontare. Sono contenta che il Governo si prenda la responsabilità di rispondere favorevolmente alle mozioni che con esso voteremo concordemente, perché sono tutte importanti e portatrici di valori fondamentali, che, proprio in questa fase di ripresa e sviluppo economico, non dobbiamo dimenticare. Chi siamo noi italiani? Quando pensiamo agli italiani, all'Italia, al Belpaese, cos'è che ci viene in mente? Sicuramente molti di noi pensano allo sviluppo scientifico e alla tecnica, ma soprattutto quello che abbiamo in mente è un'immagine: il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nostra Nazione. Così avviene per tutti

anche diffuso, com'è stato detto più volte. Il presidente Ciampi, nel maggio del 2003, legò l'articolo 9 della Costituzione all'identità: questo è fondamentale, perché da quell'articolo 9 della Costituzione, che mette lo Stato a tutela di questi beni, traiamo il concetto d'identità e di quello che siamo nel profondo e che conserviamo conserviamo della nostra immagine. Tutti i beni immateriali necessitano di un tessuto visivo locale, un *genius loci* in cui insediarsi e mettere radici e a cui ancorarsi. Tutti i nostri piccoli piccoli comparti diffusi, i centri storici consolidati (non solo quelli grandi e vincolati o le bellezze monumentali, ma anche i piccoli insediamenti) sono fondamentali per la nostra identità.

della Costituzione, perché la Repubblica ne deve promuovere lo sviluppo e deve tutelare il paesaggio. Nello stesso momento in cui spinge per dargli vigore, lo deve conservare e tutelare, ma non è una conservazione statica nel passato, bensì una conservazione attiva, di identità e di valore.

un disegno di legge sullo stop al consumo del suolo agricolo e sulla tutela del paesaggio. Sono tre tasselli fondamentali

che tende a livellare tutto, a uniformare tutto, a renderci tutti uguali e più poveri. Dobbiamo infatti ricordare che questo è il patrimonio collettivo, è ciò che ci rende ricchi, e l'unica cosa che ci rende ricchi è il bene comune.

tutelati non si può subordinare a nessun altro valore, neanche a quello economico. Eppure, le Regioni continuano a legiferare senza che lo Stato si prenda cura di quei territori; così avviene che il

poiché non aveva vincolo, per far posto ad un centro residenziale privato; così come avvenuto per i villini *liberty* di Roma. Noi non lo possiamo permettere, perché noi siamo lì, noi siamo quello;

punto - non può essere nell'assalto e nella mercificazione del patrimonio collettivo.

rilanciare questo patrimonio collettivo con la manutenzione, la tutela, il recupero, la fruizione. E dobbiamo fare in modo che provvedimenti come semplificazione o quello sull'Italia veloce non vadano in altra direzione, perché andrebbero a contraddire tutto quanto detto e tutti gli impegni presi dal nostro Governo anche in sede europea prima della crisi Covid. Mi riferisco a quelle dichiarazioni che non erano piaciute a Confindustria quando furono fatte, fino al gennaio di quest'anno. Non vorremmo che adesso la paura di non farcela da un punto di vista economico ci facesse fare degli errori come nel Dopoguerra, quando andammo, con i piani di ricostruzione, a distruggere gran parte del nostro patrimonio. Ben vengano, quindi, i livelli essenziali delle prestazioni, i piani di fruizione, i piani di manutenzione, le misure per il recupero, l'incentivazione della conoscenza nelle scuole. ben venga la richiesta di più fondi per le professionalità, per rafforzare le sovrintendenze, per dare alle professionalità del settore più forza e competenza, da inserire anche negli uffici tecnici. Possiamo velocizzare solo se le sovrintendenze, gli uffici tecnici e i geni civili saranno competenti. Dovranno essere fatte assunzioni di livello affinché

Signor Presidente, al centro della nostra mozione c'è innanzitutto il lavoro, c'è il destino di migliaia di lavoratrici e di lavoratori della cultura, che non è un loro fatto personale, ma riguarda tutti noi, il nostro Paese. Riguarda l'ambizione che abbiamo per il nostro futuro e per quello delle nuove generazioni; quale posto vogliamo occupare nel mondo, se quello di un Paese

artigianato, che ne fanno valore aggiunto fondamentale per le nostre manifatture, per la moda, per il nostro *made in Italy*; un Paese riconosciuto, rispettato, ambito, appunto, per l'enormità del suo patrimonio artistico e culturale. È per questo che diciamo con forza che non è più ammissibile che migliaia di lavoratori della cultura siano invisibili, costretti a vivere la propria passione, la propria speranza senza alcuna certezza, tra mille impedimenti e frustrazioni; costretti ad inseguire continuamente un progetto di vita che non si realizza mai, tra lavoro in nero, contratti atipici da *freelance*, intermittenti, da partite IVA, da prestatori d'opera occasionali o alla giornata, in un tempo che passa inesorabile e poi butta fuori, dopo anni di investimenti sprecati e mortifica talenti di cui invece il nostro Paese e la nostra società hanno estremo bisogno. In questo disagio dei lavoratori della cultura c'è l'immagine di un Paese che non crede in sé stesso o forse non ci ha mai creduto. E non possiamo fare finta di nulla, soprattutto nel momento in cui l'emergenza Covid squaderna in tutta la sua evidenza verità irriducibili. E queste storture c'erano anche prima dell'arrivo del virus e, del resto, gli sforzi assolutamente importanti fatti dal Governo per non lasciare solo nessuno sono stati così enormi e complicati proprio per la difficoltà addirittura di mappare in tanti ambiti i lavoratori della cultura. Per questo la crisi ci impone di ripensare, di ridefinire il nostro sistema culturale, correggendo devianze, scardinando posizioni dominanti che condizionano, soffocano; abbattendo muri che impediscono l'accesso a tante energie innovative e vitali; superando i limiti strutturali di un sistema che è troppo chiuso, troppo escludente. Fare cultura è innanzitutto un lavoro e deve essere un lavoro con piena dignità, deve essere sicuro e giusto. chiediamo uno statuto del lavoro culturale e creativo, che parta dal riconoscimento dello *status* delle professioni artistiche e sia in grado di disegnare un sistema di diritti, di protezioni sociali, costruendo una rete universale di *welfare* che sia specifica, definendo - lo chiediamo in questa mozione - livelli essenziali delle prestazioni omogenei tra le Regioni; è quello che ci hanno chiesto nelle audizioni con forza in questi giorni in Senato. Senato. La crisi innescata dal Covid moltiplica disparità e diseguaglianze territoriali e sociali; colpisce soprattutto i non garantiti, i lavoratori autonomi e le piccole imprese culturali, con storture del mercato già prima esistenti ma adesso amplificate e drammatiche. Per questo c'è bisogno di un intervento a sostegno delle produzioni indipendenti, riconoscendone la specificità.

è capacità di costruire *civitas* e c'è, in tale capacità, un nesso molto forte tra bene culturale e comunità territoriale, che sta proprio nella capacità di prendersi cura del patrimonio culturale attraverso la partecipazione diffusa dei cittadini del volontariato. La tutela non è solo riservata agli addetti, ma si fonda anche sul protagonismo di tantissimi cittadini e questo è un bene, è civismo che alimenta memoria, consapevolezza, senso d'identità, che fa dei beni culturali un grande bene comune. È un'idea della cultura aperta e non elitaria. C'è però un tema che richiamiamo nella mozione: è fondamentale che ci sia una gestione virtuosa del volontariato e non un abuso, un abuso, non un uso surrettizio a scapito dei compiti e del riconoscimento delle figure professionali dei beni culturali, che invece va rafforzato. Per tale ragione chiediamo al Governo di avviare un processo di regolamentazione del volontariato dei beni culturali, garantendo il rispetto dei ruoli tra professionisti e volontari ed escludendo, una volta per tutte, il ricorso al volontariato culturale in sostituzione e come soluzione alla carenza di personale, garantendo la tutela degli organici lavorativi, la qualità e l'offerta dei servizi culturali. Signor Presidente, in conclusione, tutte le mozioni noi le voteremo con le riformulazioni proposte - seppur diverse tra loro, sono molto importanti perché hanno il merito di politicizzare e parlamentarizzare un dibattito sulla cultura che stenta a crescere tra gli addetti ai lavori e nell'opinione pubblica, ma che pure è fondamentale perché riguarda il nostro patrimonio inalienabile, che è la nostra idea di società, la nostra idea di democrazia, quella che da un archivio o da un museo vive in un teatro, in un cinema, in una lettura in piazza, nella musica che suona in un cortile ed esprime e racchiude il significato della nostra civiltà: libertà ed emancipazione, quello che noi siamo e non possiamo perdere per alcuna ragione. *(Applausi)*.

deprecare il fatto che l'Italia, pur avendo il patrimonio culturale e artistico più ricco del mondo; pur avendo il maggior numero di siti dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, è in Europa, dopo la Grecia, il Paese che meno spende per la cultura. È un danno non soltanto ad un comparto industriale, perché la cultura è un comparto industriale; industriale; non soltanto al turismo, perché la cultura è il naturale volano del turismo; ma è un danno all'identità, parola che ho sentito citare prima dalla collega Nugnes e che - a mio avviso - è centrale in questo nostro dibattito. Chi avesse letto l'ultimo libro, tradotto da poco, di Francis Fukuyama i nuovi populismi» sa quanto l'identità culturale del singolo, delle Nazioni, dei popoli e delle comunità sia centrale per la buona crescita del singolo come delle comunità e sa anche quanto questa parola sia ormai proscritta per una serie di questioni che sarebbe lungo qui affrontare. Ma questo, colleghi, è un problema, perché, così come l'alternativa alla religione non è il trionfo della dea ragione - come qualche disperato illuminista ritiene - ma è la superstizione, allo stesso modo l'alternativa al patriottismo non è la pace e l'armonia tra i popoli, ma è il nazionalismo sfrenato. Si tratta quindi di riappropriarci di quegli elementi che costituiscono la nostra identità, in primo luogo tutto quello che ha a che fare con la cultura, la storia e il passato, e di esserne legittimamente orgogliosi. Non è un discorso di destra; potrei citare decine di intellettuali reazionari o conservatori a sostegno della tesi, ma citerò Simone Weil e Antonio Gramsci. Ne «La prima radice» Simone Weil scrive che il radicamento è forse il bisogno più importante e più misconosciuto dell'animo umano; quando parla di radicamento, intende proprio la prossimità con l'identità culturale di un popolo. Antonio Gramsci scriveva che nella svalutazione del passato è implicita una giustificazione della nullità del presente. le nostre radici le stiamo tagliando una dopo l'altra; il passato lo stiamo sistematicamente svalutando; siamo calati in un eterno presente fatto di vuoto e di nulla. Tutto questo allude a una sottocultura nichilista che non porta nulla di buono per nessuno. Come siamo arrivati a tutto questo? Ci siamo arrivati nel corso dei decenni, perché ne parliamo da poco, ma il fenomeno del politicamente corretto è antico. Ricordo uno splendido libro di uno storico dell'arte, oltre che della letteratura,

statunitense, fatta di tabù e di conformismi che annullavano l'essenza della cultura (in quel caso statunitense, ma forse della cultura in generale). Quel fenomeno si incrocia oggi con con le istanze di movimenti per i diritti civili che in sé sono più che legittime e più che condivisibili. È evidente che qualsiasi persona perbene, di cultura liberale e democratica, non può che auspicare che i diritti di ciascuno siano riconosciuti come tali indipendentemente dalle diversità di razza, di religione e di cultura. Questi movimenti però stanno travalicando se stessi e stanno assumendo una forza e un impulso nichilista (nel senso letterale), con la pretesa non di di creare le condizioni per una civile convivenza, ma di cancellare la storia. Noi ridiamo, guardiamo con distacco e con sufficienza quel che accade dall'altra parte dell'oceano, ma questa sottocultura si sta facendo largo e si è già anche nella società italiana, perché la stupidità è contagiosa e si diffonde con grande facilità. Io ricordo con raccapriccio di aver ascoltato con le mie orecchie il coro che inaugurò l'Expo di Milano. Era il 2015 si cantava l'inno nazionale, niente meno che l'inno nazionale. Qualche illuminato benpensante ritenne di rivederlo in chiave pacifista (che allude la tragedia) divenne un ignobile e mortifero (quello sì) «siam pronti alla vita». Ricordo che nella Firenze del sindaco Nardella, nella pur nobile e autorevole cornice del Maggio fiorentino, si è pensato bene di riscrivere in chiave anti femminicidio la «Carmen» di Bizet; quindi la povera Carmen in quel caso non muore, perché si sarebbe lanciato un messaggio sbagliato alla società, come se uno andasse a vedere la «Carmen» di Bizet e poi ammazzasse la moglie, la fidanzata o una qualsiasi donna incontrata per strada. C'è chi vorrebbe mettere al bando Dante Alighieri perché islamofobo. Si parla periodicamente della necessità, secondo alcuni, di rimuovere i simboli e le tracce del regime fascista: monumenti, statue, obelischi persino l'architettura razionalista, secondo alcuni - è in contrasto con la sensibilità del presente - fino alla deturpazione della statua di Montanelli a Milano. Pare che che Montanelli, da giovane ufficiale dell'esercito italiano coloniale in Eritrea, abbia preso in moglie una minorenne eritrea; cosa che naturalmente, con la nostra sensibilità di oggi, ci fa più o meno orrore. Ma, nella sensibilità di oggi, giudicare il passato con le categorie etiche del presente è un errore, perché impedisce di capire e di comprendere il passato e porta a delle vere mostruosità rispetto alla storia e rispetto all'identità. È questo che io credo dovremmo combattere, perché questo modo di fare è tipico dei regimi dittatoriali e dei sistemi fondamentalisti religiosi. E noi, che non abbiamo particolare simpatia per le dittature del Novecento, né particolare affinità con le teocrazie contemporanee, dovremmo avere la forza morale e il coraggio civile di opporci, in nome della nostra storia, perché la storia si disincanta e si rivede, ma non si cancella se si ha rispetto di se stessi perché - come diceva il cantante - in fondo «la storia siamo noi». Quindi, la richiesta al Governo è di fare il possibile affinché in questi anni di legislatura la spesa pubblica per la cultura legislatura la spesa pubblica per la cultura italiana si allinei quantomeno alla media europea e perché tutto quello che appartiene alla nostra identità storica, culturale, artistica e monumentale venga tutelato, ricordando anche l'opportunità - lo ha detto il collega Aimi di occuparci di un aspetto che mi sembra sgradevole, ma necessario: il codice penale. La Convenzione dell'Aja classifica come reati di guerra e crimini contro l'umanità l'abbattimento di simboli o di opere dell'ingegno e d'arte disposizione è stata scritta nel 1954, quando non si arrivava proprio a concepire che la minaccia a un monumento nazionale potesse venire da altri, se non da un esercito straniero.

rappresentanti del Governo, colleghi, una tutela realmente efficace del nostro patrimonio culturale passa attraverso due aspetti fondamentali: da un lato, la protezione delle opere d'arte dagli atti vandalici e dalle altre numerose condotte criminali posti in essere contro i nostri beni artistici, attraverso un complesso di norme *ad hoc* che puniscano gravemente gli autori; dall'altro lato, l'utilizzo delle tecnologie più avanzate in grado di supportare i processi di monitoraggio diagnostico e fruizione sostenibile dei beni culturali, ovvero che tengano conto sia delle mutazioni dell'ambiente circostante, sia delle caratteristiche degli utenti, al fine di ottimizzare la fruizione di un ambiente culturale. Riguardo al primo aspetto, tutti ricordiamo lo spiacevole episodio dell'agosto 2015: l'orrendo atto di vandalismo perpetrato ai danni della fontana della Barcaccia del Bernini in piazza di Spagna a Roma. Non credo ci sia stato un solo cittadino italiano che non si sia sentito ferito personalmente da quell'atto dissennato, perpetrato gratuitamente da alcuni tifosi stranieri, i quali non hanno pagato quasi niente perché il giudice italiano non li ha potuti processare in quanto erano già stati processati in Olanda. Tuttavia, se anche fossero stati condannati, in base alle normative vigenti, avrebbero rischiato al massimo fino a un anno di reclusione per danneggiamento e un'ammenda non inferiore a circa 2.000 euro. Tutto ciò è ridicolo e svilente e questo non è sicuramente l'unico caso. Purtroppo non sono così rari i momenti in cui assistiamo a episodi di maleducazione, ignoranza e inciviltà: chi si fa il bagno nelle fontane, chi si arrampica sui monumenti, chi deturpa gravemente un patrimonio inestimabile per il nostro Paese. Tutto ciò è ridicolo. Noi chiediamo di inasprire le sanzioni e anche le pene pecuniarie, se vogliamo che funzionino davvero come deterrente per evitare che atti simili si ripetano. Si sa che il mercato abusivo di scavi e beni archeologici e pittorici trafugati non di rado finisce nel circuito clandestino. Alcune volte dei reperti vengono addirittura posti in vendita nelle aste ufficiali di importanti case, generalmente straniere. A nostro avviso, sarebbe necessario applicare delle sanzioni anche alle persone giuridiche che fanno mercato di queste opere indebitamente sottratte al patrimonio nazionale. Lo Stato d'altra parte - noi puntiamo molto su questo, perché abbiamo fatto anche delle audizioni al riguardo - dovrebbe stare al fianco di quelle associazioni e fondazioni che, al contrario, tutelano e valorizzano le opere d'arte, dando anche un grande supporto a tutti i tessuti territoriali. Il nostro patrimonio artistico è minacciato dalla criminalità organizzata che ha fatto dello scavo e della ricettazione un importante *business* della propria attività.

La banca dati dei beni culturali sottratti illecitamente ci riporta dei dati davvero preoccupanti: nel 2018, quasi 800.000 opere d'arte trafugate, 1.200.000 sequestri di reperti archeologici e quasi 300.000 beni falsificati, con 1.200 arresti e 36.000 denunce. Oltre ad intervenire con norme interne in materia, è necessario ratificare la Convenzione di Nicosia del 2017, che è stata sottoscritta anche dall'Italia insieme ad altri otto Paesi, al fine di adeguare il nostro ordinamento ai principi in essa indicati e che mirano ad inasprire l'apparato sanzionatorio in materia di reati contro il patrimonio culturale. Inoltre, l'attuale tutela penale del patrimonio storico e culturale italiano presenta alcune lacune. In particolare, risulta priva di coerenza, divisa tra codice penale e codice dei beni culturali. È di fondamentale importanza che nell'ipotesi in cui vi sia condanna per una delle fattispecie come il furto, la ricettazione, l'illecita esportazione, il danneggiamento o l'imbrattamento, venga irrogata la misura della confisca obbligatoria sia dei beni che sono prodotto o profitto del reato, del reato, sia delle cose servite per commetterlo. Anch'io sono una appassionata di patrimonio artistico e culturale e credo che la tutela delle opere d'arte in genere non debba dipendere da un periodo storico. Il punto di partenza è il momento del riconoscimento dell'opera d'arte come tale. Un'opera d'arte non è solo un oggetto di importanza storica, ma un momento storico che si fa materia e in cui una cultura nazionale si riconosce. Occorre parlarne di più, occorre iniziare a formare gli studenti, perché il nostro patrimonio artistico non deve essere patrimonio di pochi cultori. Il nostro patrimonio artistico è lo specchio e il ritratto della nostra Nazione, della sua storia, del suo presente e del suo futuro. La cura e l'attenzione che noi mettiamo nei confronti del nostro patrimonio culturale è il termometro del nostro livello civico e culturale, quindi occorrono regole e sanzioni certe.

Tutti ci dobbiamo impegnare nel preservare i nostri tesori storico-artistici, che sono messi a dura prova non solo dal tempo, ma sempre più spesso dalla mano dell'uomo. E solo in tal modo, tutelando il nostro passato e le nostre tradizioni, preserveremo il nostro futuro. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi senatori, prendo la parola per condividere con quest'Aula qualche considerazione di ordine generale, prima di esprimere l'intenzione di voto favorevole del mio Gruppo alla mozione sul patrimonio artistico illustrata dalla senatrice Montevecchi. Vorrei cominciare richiamando alla vostra memoria i punti 20 e 27 del programma di questo Governo, presentato appena una decina di mesi fa, anche se sembrano trascorsi secoli dopo l'esperienza straniante della pandemia. In tali punti si trattavano i temi afferenti in modo diretto o indiretto al patrimonio culturale. Al punto 27 se ne parlava in relazione alla promozione di multiformi percorsi del turismo che valorizzino - cito alla lettera - «la ricchezza del nostro patrimonio naturale, storico, artistico e culturale, anche attraverso il recupero delle più antiche identità e delle tradizioni locali». Il riferimento si chiudeva con la considerazione inoppugnabile, ma per verità generica, secondo cui la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese sono obiettivi prioritari dell'azione di Governo. Governo. L'ho definita una considerazione generica per l'assenza di qualunque riferimento alla conservazione del patrimonio in funzione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, come invece plasticamente rilevabile dalla lettura coordinata del comma 2 dell'articolo 9 della Costituzione, che individua la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione quali doveri ineludibili dello Stato repubblicano, con il comma 1 dello stesso articolo, che finalizza la tutela alla promozione e allo sviluppo della cultura e della ricerca. Questa lacuna, a così alto livello, era il frutto, a mio avviso, dell'imporsi nella società italiana degli ultimi decenni di una visione strumentale del patrimonio, inteso in funzione puramente economicistica e - oserei dire - mercantile. Vogliamo imputarla al berlusconismo che ci ha modificati tutti geneticamente? Ciascuno avrà la sua spiegazione, ma la caduta della tensione morale e l'impoverimento culturale del Paese sono dati oggettivi e la crisi della scuola pubblica vi ha molto a che fare. Quella lacuna non poteva non destare perplessità in termini assoluti e in rapporto al programma di Governo medesimo, soprattutto di fronte a un discorso del Presidente incaricato che, lo ricorderete, infiammando i cuori degli umanisti, aveva fatto riferimento esplicito alla necessità per questo Paese di un nuovo Rinascimento. Ebbene, lo ricordo a me stessa, il Rinascimento è stato il risultato e - direi - il fiorire, in termini creativi e di sensibilità, dell'Umanesimo, connotato dalla riscoperta del mondo classico attraverso lo studio e l'indagine dei testi. Destava sconcerto, perciò, che il prefigurarsi come obiettivo di questo Governo l'impulso verso un nuovo Rinascimento non prevedesse alcun passaggio programmatico incentrato su un nuovo Umanesimo, cioè sulla tutela del patrimonio intesa non come mera conservazione, ma come studio e fruizione del patrimonio stesso per finalità eminentemente di conoscenza e di crescita culturale. Queste sono le ragioni per cui a tanti oggi piange il cuore vedendo ancora chiusi archivi e biblioteche e un terzo dei musei. Era assai spiacevole non solo per me, avendo il MoVimento da sempre un approccio diverso, cogliere nel ripetuto riferimento a tale patrimonio solo in chiave strumentale e quale attrattore di flussi turistici, possibilmente a sette cifre, antichi riverberi dell'idea di patrimonio culturale come petrolio d'Italia, la scorciatoia per un arricchimento facile alla portata di tutti e garantito dalla mera offerta commerciale delle nostre memorie e del nostro passato, secondo un'impostazione che rischiava di vederci proni ai desiderata turistici, invece che artefici del nostro futuro attraverso e grazie agli stimoli creativi derivanti dall'approfondita conoscenza di ciò che è stato e delle straordinarie testimonianze per numero e qualità che il passato ha lasciato sul nostro territorio. Queste sono le ragioni stesse, peraltro, della preferenza del turismo internazionale per il nostro Paese. Non starò qui a dare numeri o, meglio, le percentuali, come hanno fatto alcuni colleghi più temerari. Semplicemente non è calcolabile a quanto ammonti il patrimonio artistico e culturale italiano sia in assoluto sia in confronto agli altri Paesi. Chi si avventura nella pseudo statistica, accetta di partire da presupposti inconsistenti e, cioè, dal numero dei beni immobili censiti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Per la cronaca, siamo ancora primi con 54, ma la Cina ci tallona con 53. un criterio talmente inaffidabile che, se lo adottassimo per i beni culturali immateriali, saremmo costretti ad ammettere una sorprendente minorità rispetto a moltissimi altri Stati per la semplice ragione che abbiamo iniziato tardi a riconoscere valore ai beni culturali immateriali. Dal 2011 poi, ciascun Paese può candidare solo un nuovo bene immateriale ogni anno. Sicché, Achille non supera la tartaruga. Personalmente mi ero ripromessa di vigilare per scongiurare la deriva paventata lo scorso autunno e denunciarne, come poi ho fatto, ogni avvisaglia. I timori della vigilia si sono in effetti rivelati fondati: il patrimonio come strumento per altri fini e come petrolio continua ad avere, persino nel vertice ministeriale, il suo campione, ma il caso ci ha messo lo zampino e la pandemia da Covid-19 ha rimescolato le carte. Quella deriva oggi può essere fermata. La crisi dolorosissima del turismo, lo stesso turismo però che ha azzannato le nostre principali città d'arte e ha divorato Venezia, può e deve imporci un salutare ripensamento delle ragioni per le quali in questo Paese per almeno duecento anni si è fatta realmente tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. La tutela e la valorizzazione vanno solo in questo ordine, ma entrambe hanno l'obiettivo di assicurare la fruizione dei beni culturali a tutti i cittadini, ormai riconosciuta servizio essenziale. Perché garantire la fruizione? Perché, alimentando il senso di appartenenza e il sentimento dell'identità nazionale, le dinamiche culturali generino nuova cultura. Nel frangente odierno, colleghi, noi tutti siamo chiamati a dare un segnale in rapporto a una decisione cruciale: o continuare su quella strada, appostando, però, risorse adeguate, o ammettere senza ipocrisie che non ci riconosciamo più in tali obiettivi e rinunciare a perseguirli solo sulla carta, svuotati di senso, come ci stiamo, purtroppo, abituando a fare. a fare. Volendo fare un esempio concreto e attuale, penso al PNR 2020, in cui, tra le priorità enunciate in tema di patrimonio culturale, la tutela praticamente non c'è. Almeno duecento anni, ho detto poco fa, riferendomi all'editto Pacca del 1820, antenato comune delle legislazioni di tutela pre-unitaria e post-unitaria. Troppo spesso, infatti, dimentichiamo che è stata la cultura a fare l'Italia, in concorso con la geografia, ma ben prima della storia e della politica. E dimentichiamo che Roma ha giustamente un ruolo prioritario da sempre in questo processo. Definire una politica di tutela del patrimonio culturale di Roma, considerato nel suo stratificarsi storico obiettivo adombrato al punto 20) del programma di Governo - è una necessità assoluta. Nella Capitale bisogna, infatti, porre un argine alle trasformazioni dell'edilizia di fine Ottocento-inizio Novecento, ma le stesse testimonianze archeologiche di Roma sono sottoposte ad aggressioni continue. Si impone, insomma, una rigorosa azione di vigilanza. Occorre che il Ministero doti la Capitale di una soprintendenza di livello dirigenziale generale e ne affidi la guida a persona inflessibile nel perseguire l'interesse pubblico. Roma, però, è anche lo specchio del Paese, dove una scellerata politica di tagli ha quasi azzerato negli anni le assunzioni nel Ministero dei beni e delle attività culturali, al quale mancano oggi quasi 10.000 unità, e non può certo sostituirle il volontariato, togliendo di fatto al personale degli uffici territoriali unificati - replicando l'errore già commesso negli anni Venti del Novecento - la possibilità di lavorare con la dovuta diligenza su un patrimonio diffuso capillarmente, che richiede senso di responsabilità individuale e collettivo, cure amorevoli quanto continue, minacciato e depredato com'è - soprattutto se parliamo di beni mobili - anche da criminali che fanno capo a organizzazioni malavitose alle quali il traffico internazionale di opere d'arte frutta ormai quasi quanto quello delle armi. È sotto gli occhi di tutti che l'edilizia storica, urbana e rurale, in mancanza di un piano strategico che la preservi, incentivando, o almeno rendendo più conveniente il recupero rispetto alla sostituzione, rischia di scomparire in pochi anni. La insidiano persino i solerti - quanto ignari - Vigili del fuoco, chiamati a scongiurare i pericoli per la pubblica incolumità causati dalla ruderizzazione conseguente ai mancati restauri (avrete visto cosa è accaduto due giorni fa a Casaletto Lodigiano, ma accade ovunque) e, d'altro canto, i palazzinari pronti a sfruttare le lacune della vincolistica sia nei centri storici sia fuori dagli abitati. L'assalto portato oggi al paesaggio, poi, soprattutto nel Sud Italia, nasce dalla stessa povertà spirituale che stenta a riconoscere dignità ai beni artistici, se non in proporzione alla loro capacità di attrarre flussi turistici, dunque di generare profitti. La pandemia, che, però, ha azzerato i flussi turistici esteri, ci costringe oggi a cercare nuove ragioni per agire, a decidere cosa vogliamo fare della nostra blasonata eredità culturale e a farlo in concreto nel quotidiano, a Roma come nell'ultimo degli altri 8.000 Comuni italiani. L'aspirazione a un nuovo Umanesimo - asserito a suo tempo dal Presidente del Consiglio - va, dunque, posta realmente al centro dell'azione di Governo. Deve essere un obiettivo condiviso e trasversale; deve farsi opportunità concreta che impegna l'Esecutivo, ma vorrei dire tutta l'Assemblea, a votare la mozione a prima firma della collega Montevecchi per dare il segnale di un'inversione di tendenza, e subito dopo agire nella direzione che tutti auspichiamo, riconoscendo, cioè, nel patrimonio artistico e nella sua conservazione una componente imprescindibile del nostro DNA di italiani. Dichiaro, quindi, il voto favorevole alla mozione n. 263

Signor Presidente, chiediamo la votazione per parti separate del terzo punto delle premesse della mozione n. 264, che fa riferimento alla Convenzione di Faro. Com'è noto, noi, come Lega, abbiamo votato contro la ratifica e la consideriamo

dopo una giornata campale come quella di oggi, l'argomento di cui vi voglio parlare vi potrà apparire banale. Io voglio parlare di cinghiali e di lupi. Se incontraste un cinghiale o un lupo testa a testa forse chi è contrario al loro abbattimento cambierebbe idea. Sono pericolosi per le persone. Troppi fatti hanno coinvolto le persone, gli animali, i greggi, i beni privati. Se penso alla manifestazione del novembre-dicembre scorso in piazza Montecitorio, in cui il Ministro dell'agricoltura - lo dico alla maniera della Prima Repubblica - e parecchi senatori fecero delle dichiarazioni di impegno, mi vien voglia di dire che ci siamo dimenticati della questione troppo in fretta rispetto alla gravità Quando la politica dice che dobbiamo monitorare, che dobbiamo vedere, che vedremo, che faremo, non arriva nessun risultato. Ora, io credo che i cinghiali in Italia siano almeno un milione (ma mi sbaglio per difetto) e che i lupi siano parecchie migliaia, che siano stati inseriti dall'uomo con finalità positive, ma che poi si siano moltiplicati troppo,

Aggiungo ancora una premessa, anche se sono alla fine: non si tratta di un argomento di centrodestra o di centrosinistra; è un argomento di sensibilità personale,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, il mio intervento di oggi è per portare a conoscenza di quest'Assemblea quanto accaduto nei giorni scorsi in Val di Susa. Quest'area del Piemonte, a forte vocazione turistica e con il merito di aver fatto conoscere Torino e le sue valli al mondo intero, grazie alle Olimpiadi invernali del 2006, da due lustri ormai è alla ribalta delle cronache solo ed esclusivamente per le contestazioni al cantiere di Chiomonte. Manifestare democraticamente per ciò in cui si crede è un dogma per noi della Lega, ma nel corso degli anni i pacifici manifestanti residenti sono stati sostituiti dagli anarco-insurrezionalisti. Il mio intervento di fine seduta a luglio ormai è un appuntamento fisso, perché a luglio si svolge il No TAV Camp, che puntualmente si conclude con l'attacco al cantiere. Tra i partecipanti all'evento, vi sono componenti dei centri sociali di Torino, Milano, Bologna, Oltralpe, ma anche ex terroristi di prima linea e brigate rosse. Nel corso degli anni la procura della Repubblica di Torino ha emesso più di mille avvisi di garanzia per i reati che vanno dagli atti vandalici al tentato omicidio. Il 2020, però, ha evidenziato una *escalation* violenta di una gravità inaudita e inaspettata: la tentata strage. Tentata strage, perché disseminare le corsie di emergenza dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia di chiodi a tribolo romano per provocare incidenti è da assassini *in pectore* o da dementi. Solo per un caso fortuito e per la professionalità delle Forze dell'ordine non si è verificato un incidente mortale. Tuttavia più di un mezzo della polizia è stato accidentato e alcuni sono andati a sbattere contro il *guard rail*. Diverse auto di cittadini, famiglie in vacanza, moto hanno forato le gomme sbandando e rischiando la tragedia. Quanta pazienza dovranno ancora avere i valsusini? Il tutto con il rumorosissimo silenzio del Governo e del ministro Lamorgese, come dimostrato dai comunicati stampa della quasi totalità dei sindacati di Polizia. Si rende, quindi, necessario intervenire prontamente in modo drastico, per evitare che questi episodi si ripetano. Non è più accettabile consentire l'organizzazione di raduni e *camp* finalizzati solo all'attacco al cantiere e alle Forze di polizia; non è più ammissibile permettere che componenti di questa maggioranza sostengano l'operato di queste frange violente, giustificandole e criticando le Forze dell'ordine. Ogni forma di giustificazione legittima e fomenta ulteriori violenze. Mai come ora è necessario e auspicabile far sentire alle Forze dell'ordine la vicinanza dello Stato (quella della popolazione per bene ce l'hanno già). Pugno duro e pene certe contro chi usa come *totem* l'Alta velocità e i suoi cantieri, ma che in realtà vuole attaccare lo Stato attraverso le sue istituzioni. Denuncia per tentata strage agli autori del folle gesto della A32 e per il lancio di bombe carta contro gli agenti di polizia a presidio dei Denuncia per tentata strage agli autori del folle gesto della A32 e per il lancio di bombe carta contro gli agenti di polizia a presidio dei cantieri. Il tutto perché la vita di un poliziotto o di un militare non vale meno della nostra, anzi. E il messaggio deve arrivare a tutti forte e chiaro.

La piccola è prigioniera delle norme sanitarie per il contenimento del contagio: le autorità sanitarie ritengono che non sia più un pericolo per gli altri, ma, come dichiarato dalla madre, serve un doppio tampone negativo per liberarla. Questa bambina quindi, che da quattro mesi è prigioniera, ha avuto all'inizio sintomi riconducibili al Covid: il 24 marzo aveva la febbre alta e i medici avevano accertato però che non aveva disturbi polmonari e l'hanno rimandata a casa senza *test*; successivamente

che la figlia è tormentata dagli incubi, si sveglia urlando, parla di mostri e dottori cattivi, comincia a manifestare disturbi comportamentali, non vuole farsi toccare o salire in auto. Tutti le hanno confermato che la bambina non è più contagiosa, ma nessuno si è assunto la responsabilità di liberarla. La mamma chiede che si valutino altri elementi per la fine della quarantena. Ne approfitto in conclusione per ricordare che in Olanda, dall'inizio del *lockdown*, che è stato diverso in Italia (perché noi ne abbiamo avuto uno tutto italiano) sul sito del Ministero della salute c'è scritto: pensi di avere il coronavirus? Le autorità rispondono: se ti senti meglio e non hai sintomi per ventiquattr'ore sei guarito, allora non puoi più infettare gli altri. Siccome in Olanda - dove, se non avevi sintomi, eri guarito - i morti per 1.000 abitanti sono meno della metà di quelli italiani, penso che la versione giusta sia proprio quella e quindi, se non hai sintomi, puoi uscire e non

spero che questa vicenda si risolva presto.

ma anche per lo stravolgimento del vivere sociale in cui le problematiche generali, le difficoltà economiche e i contrasti culturali creano purtroppo l'ambiente e le condizioni favorevoli al verificarsi di fatti come quello citato, che non sarà certamente l'ultimo. Quanto ricordato riporta alla mente le tristi immagini, purtroppo abbastanza frequenti, di neonati abbandonati, spesso con il cordone ombelicale ancora attaccato, nei cassonetti dei rifiuti o su una panchina dei giardinetti pubblici, esposti al freddo, alla pioggia, al caldo o a possibili infezioni per la scarsa igiene, in un momento particolare della loro vita. Tutto ciò spesso mette a rischio la loro stessa incolumità. Allora ben vengano queste iniziative delle culle termiche, che potremmo definire culle per la vita o culle sociali, in cui il neonato può essere lasciato in sicurezza e nell'anonimato e da lì ricevere l'opportuna assistenza e le giuste cure, non solo mediche, con farmaci e latte, ma soprattutto un supporto psicologico, una carezza amorevole, un sorriso amichevole, un gesto d'amore. Ricordo quasi con nostalgia la ruota degli esposti dell'ospedale Annunziata di Napoli (dove lavoro), oggi un cimelio storico che però tante storie più o meno a lieto fine ha vissuto e potrebbe raccontare. Nella ruota i tanti piccoli Esposito sono stati lasciati con tanto amore e speranza per ricevere quelle cure e quegli aiuti concreti necessari per sopravvivere che i loro genitori erano impossibilitati a dar loro. Secondo me la possibilità di offrire una culla termica, un riparo concreto nei vari punti nascita o in strutture che si offrono volontariamente come le chiese, in cui, quando le condizioni familiari sono così gravemente compromesse e sconvolte, i genitori possono lasciare queste piccole creature innocenti, salvando loro la vita, può e deve essere una soluzione e una risposta concreta e attuabile. Queste culle supertecnologiche, che potremmo definire moderne ruote degli esposti, sono già circa 50 su tutto il territorio nazionale, ubicate presso diverse strutture sanitarie o ospedaliere. Occorre solo un'informazione più diffusa e capillare. Certamente il supporto economico, psicologico e di guida delle strutture pubbliche a ciò preposte rappresenta la soluzione che dovrebbe essere perseguita, però necessita ovviamente di una programmazione attenta, capace di riconoscere situazioni familiari a rischio e di dare un supporto efficace e concreto per risollevarle. Quando ciò non è possibile a causa di pastoie burocratiche, di cattiva organizzazione o di complessità del quadro familiare, offrire un rifugio temporaneo al piccolo neonato è da prendere in seria considerazione, al fine di evitare le piccole grandi tragedie che si verificano non solo nel nostro nostro Paese. Non facciamo solo discorsi o sermoni che lasciano il tempo che trovano. La vita di ogni giorno ci pone spesso di fronte a scelte difficili. Non dimentichiamo mai però che al centro di ogni decisione e di ogni presa in carico si deve anteporre l'interesse del bambino, neonato o lattante che sia *(Applausi)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la diffusione dell'infezione da Covid-19 resta un problema molto grave ed è notizia di questi giorni che ci sono stati oltre 250.000 nuovi casi di Covid a livello mondiale: è il nuovo *record* di contagi in un solo giorno. I dati generali parlano di oltre 15 milioni di casi positivi e di oltre 600.000 morti nel mondo; nei Paesi molto popolosi l'incidenza della diffusione pandemica è elevata e ricordiamo che c'è stata un'impennata della diffusione nelle popolazioni del continente africano, negli Stati Uniti, in Brasile, India e Perù. L'evento pandemico ha colpito anche il nostro Paese, ma grazie alle misure adottate si è potuto arginare il problema, anche se resta aperta la potenzialità della ripresa dei focolai nel caso in cui non venissero rispettate le norme comportamentali. Questo ci dice che siamo nel pieno della battaglia contro il virus, quindi è fondamentale continuare a tenere comportamenti corretti: uso della mascherina, distanziamento di almeno un metro e lavaggio frequente delle mani. mentre vengono regolamentati i controlli dei passeggeri in aeroporti, porti e nelle stazioni ferroviarie, resta il grave problema dei confini Sud dell'Europa, in special modo lungo le coste del Mediterraneo che si affacciano sul continente africano. In questi Paesi le misure di contenimento possono essere applicate con molta difficoltà rispetto ai Paesi europei, americani o asiatici. Le motivazioni sono riconducibili alle problematiche politiche (che rendono molte volte impossibili le azioni dei Governi o

l'assenza in molti Paesi africani di dati e di statistiche attendibili non permette di avere il quadro reale della diffusione del virus, così da rendere ancora più difficoltosa la possibilità di un intervento sanitario basato sulla corretta ed efficace prevenzione. A fronte di questa situazione così gravosa, purtroppo, con mezzi di ventura e mettendo a rischio la propria vita, i migranti, sperando in una vita migliore, fuggono da aree con carestie e guerre dove la morte è certa e imboccano la porta del Sud dell'Europa per arrivare nel nostro continente con barconi fatiscenti e, soccorsi in mare, approdano nelle isole Pelagie, Lampedusa e Linosa. Questi migranti vengono alloggiati in *hotspot* stracolmi e riescono spesso ad eludere la sorveglianza fuggendo. È notizia di queste ore che solo nell'*hotspot* di Lampedusa sono presenti oltre 500 migranti, con conseguenti possibili serie problematiche sanitarie. Peraltro, risulta che dalle località sopra citate i migranti vengono trasferiti presso la città di Porto Empedocle, con evidenti problematiche relative all'accoglimento e alla forte preoccupazione degli esercenti e della popolazione in generale. A tal proposito si fa presente che il sindaco Ida Carmina ha più volte evidenziato le problematiche sopra citate che generano negative ripercussioni anche sul flusso turistico e quindi sull'andamento economico dell'area in questione. La Sicilia, quindi, ancora una volta è la frontiera dell'Europa e, a quanto sopra elencato, si aggiunge anche il problema degli sbarchi fantasma, con piccole imbarcazioni che, riuscendo ad eludere i controlli in mare aperto, possono sbarcare sulle coste siciliane senza il minimo controllo e contenimento. Ferma restando l'accoglienza ai migranti, specie di chi fugge da guerre e carestie, è assolutamente necessario mettere in atto tutte quelle misure di controllo sanitario con tampone per mettere in quarantena i positivi e prendere le misure necessarie per evitare che si possano verificare focolai diffusivi che potrebbero vanificare tutti gli sforzi che gli italiani hanno compiuto. Per questo è necessario un fermo richiamo del Parlamento ai competenti organi affinché non si abbassino assolutamente la tensione e